una nuova finestra"). Comunico che in data 4 marzo è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7» (1056). **Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel

la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di dieci minuti per Gruppo, con cinque minuti aggiuntivi in via eccezionale per il Gruppo Misto. Ha facoltà di parlareil Ministro degli affari esteri e della cooperazione

Considero giusto e urgente condividere con il Senato della Repubblica le motivazioni che hanno indotto il Governo a promuovere due nuove missioni. Si tratta dell'operazione Levante in Medio Oriente e del dispositivo multi-dominio nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, in cui è compresa anche la missione europea Aspides. Sabato scorso, come sapete, il cacciatorpediniere Caio Duilio ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi nello stretto di Bab El Mandeb e sono certo che tutta l'Assemblea del Senato vorrà rinnovare all'equipaggio del Caio Duilio e a tutte le Forze armate la profonda gratitudine per il loro costante e prezioso operato. L'attacco al nostro cacciatorpediniere conferma ancora una volta la gravità della minaccia terroristica degli Houthi e la tempestività delle iniziative che il Governo ha deciso di intraprendere. attaccata la nave Sky II battente bandiera liberiana, di proprietà svizzera, e diretta a Gibuti. La situazione nel Mar Rosso va inquadrata nella più ampia crisi in Medio Oriente scatenata dai brutali attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Come ho già avuto modo di riferire in Parlamento in diverse occasioni, il Governo italiano ha operato perseguendo alcuni obiettivi fondamentali: innanzitutto favorire il rilascio incondizionato degli ostaggi e consentire l'accesso umanitario; evitare un'*escalation* nella Regione; promuovere un cessate il fuoco; creare le condizioni minime per far prevalere la via della diplomazia e della politica su quella delle armi e della Abbiamo appreso con sgomento della strage di giovedì scorso a Gaza: un massacro di civili inermi che ha complicato, purtroppo, anche i negoziati in corso per il raggiungimento di una tregua. Nessuno può cancellare i fatti del 7 ottobre: è stata la spietata caccia all'ebreo scatenata da Hamas ad innescare il conflitto. Tuttavia sono troppe le vittime palestinesi che non hanno nulla a che vedere con i terroristi. La strage del pane impone di intensificare gli sforzi per giungere al più presto ad un cessate il fuoco. Abbiamo chiesto ad Israele di accertare con rigore la dinamica dei fatti e le responsabilità. È fondamentale, onorevoli senatori, continuare a lavorare per un rapido rilascio degli ostaggi, ma anche per incrementare gli aiuti nella Striscia di Gaza, altrimenti corriamo il rischio di una catastrofe umanitaria ancor più devastante. Dobbiamo far arrivare alla Striscia tutti gli aiuti alimentari di cui c'è bisogno. Desidero promuovere un'iniziativa umanitaria coordinata, che ho chiamato «Pane per Gaza», in inglese «Food for Gaza». *(Applausi)*. Ne ho parlato qualche istante fa con il direttore generale della FAO e poi ne parlerò con la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale. Intendo riunire la prossima settimana, probabilmente lunedì, al Ministero degli affari esteri un primo tavolo anche con la Mezzaluna Rossa e con altre organizzazioni. L'obiettivo è quello di fare sistema per agevolare l'accesso degli aiuti e alleviare le sofferenze della popolazione. Il momento è ora, nella prospettiva di un auspicato cessate il fuoco. Noi sosteniamo il dialogo degli americani di queste ore con i Paesi arabi moderati. Il successo di un intervento umanitario coordinato potrà a sua volta facilitare le condizioni di uno sbocco politico cui tutti lavoriamo. lo sapete, non nasce certamente oggi: fin dall'inizio della crisi, il Governo italiano ha trasmesso beni di prima necessità per un totale di 16 tonnellate, con velivoli dell'Aeronautica militare. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per interventi umanitari nella Striscia, con particolare attenzione all'emergenza sanitaria ed alimentare. Con i primi 10 milioni abbiamo finanziato, a inizio dicembre, la Croce Rossa internazionale, la Mezzaluna Rossa e le agenzie delle Nazioni Unite. ho subito riferito in Parlamento, abbiamo stanziato altri 10 milioni di euro, destinati appunto alle agenzie del polo ONU di Roma, all'Organizzazione mondiale della sanità, all'Agenzia umanitaria dell'Unione europea, ad organizzazioni della società civile italiana. Tra le attività previste ci sono anche lo sminamento e la rimozione degli ordigni inesplosi a Gaza. Abbiamo altresì, come sapete, inviato una nave della Marina militare, la nave Vulcano, con a bordo un ospedale con TAC, capacità chirurgica e di rianimazione. La nave è rimasta nel porto di Al-Arish, in Egitto, per due mesi, fino al 31 gennaio, prestando supporto medico a pazienti provenienti da Gaza. La nave Vulcano è rientrata in Italia il 5 febbraio con a bordo minori palestinesi e i loro familiari; i piccoli stanno ricevendo cure mediche specialistiche nei migliori ospedali pediatrici del nostro Paese. Altri erano stati trasportati in Italia con due voli dell'Aeronautica militare, sempre nell'ambito dell'iniziativa volta a prestare cure mediche indispensabili a 100 bambini bambini palestinesi. Il Governo è pronto a ripetere questa operazione, se sarà possibile farlo, abbiamo già dato la nostra disponibilità a trasportare nel nostro Paese altri 100 bambini feriti nella Striscia di Gaza. Si è trattato di un'iniziativa unica in Europa, resa possibile dal grande lavoro di squadra che coinvolge tutti gli attori del sistema Italia e il terzo settore: la Caritas, la Federazione delle chiese evangeliche, la Comunità di Sant'Egidio e l'ARCI. l'ARCI. L'operazione nazionale Levante in Medio Oriente si inserisce nella stessa linea di azione e ha fra i suoi obiettivi quello di aderire all'iniziativa multinazionale *Maritime Aid to Gaza*, volta all'apertura di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari con approdo diretto nella Striscia di Gaza, a partire da un polo logistico da costruire a Cipro. Devo dire che durante le riunioni del Consiglio affari esteri l'Italia è stata la prima ad accettare e a sostenere la proposta del Governo cipriota. Altro obiettivo è quello di paracadutare materiale umanitario sulla Striscia, alla stregua di quanto stanno già facendo altri *partner* come la Francia e la Giordania. Vogliamo fornire ulteriore supporto sanitario a favore della popolazione palestinese tramite lo schieramento di un ospedale militare da campo. A tutto ciò si aggiunge anche la necessità di salvaguardare l'incolumità dei nostri connazionali, civili e militari, presenti nell'area mediorientale. Ricordo che in Libano, tra la missione UNIFIL delle Nazioni Unite e la missione bilaterale MIBIL a favore delle Forze armate libanesi, abbiamo oltre 1.000 militari italiani schierati. Per questo il nostro sforzo è sempre stato orientato anche alla protezione dei contingenti nazionali, prevedendo l'innalzamento delle misure di sicurezza e la predisposizione di eventuali operazioni di evacuazione. Sul piano politico-diplomatico, resta essenziale raggiungere un cessate il fuoco sostenibile a Gaza, anche per attenuare le tensioni regionali. L'Italia chiede una pausa prolungata e duratura delle ostilità che porti a un cessate il fuoco sostenibile, come richiesto anche dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Il conflitto tra Israele e Hamas ha già avuto un impatto devastante sulla regione, dove sono attivi diversi focolai di tensione: all'allargamento degli scontri in Cisgiordania e l'incremento di intensità nel confronto tra Forze armate israeliane ed Hezbollah lungo il confine libanese, le recenti tensioni in Siria, Iraq e, in parte, anche tra Iran e Pakistan, per non parlare degli attacchi degli Houthi. L'Italia partecipa attivamente, insieme ai suoi principali alleati e ai Paesi arabi moderati, ad ogni sforzo utile a contenere l'incendio. Durante la mia ultima missione in Libano, Israele e Palestina, a fine gennaio, ho ribadito a tutti gli interlocutori l'importanza di affrontare la crisi con mezzi politici. Ho sottolineato la necessità di un credibile e concreto percorso verso la soluzione "due popoli-due Stati", con il contributo di un'autorità palestinese rafforzata e riformata. Le dimissioni del primo ministro Shtayyeh e la formazione di un futuro governo dell'Autorità nazionale palestinese sono un segnale importante in questa direzione. In parallelo, dobbiamo rilanciare i processi di normalizzazione e integrazione regionale. Un quadro regionale favorevole è essenziale per il successo di qualsiasi iniziativa politica. I Paesi arabi che più si stanno attivando per la ricerca di una soluzione possono svolgere un ruolo essenziale nella riabilitazione di Gaza e nel favorire l'integrazione economica con Israele. La condizione è che vi sia un impegno chiaro ed irreversibile per la creazione di uno Stato palestinese indipendente. In questo quadro fragile e complesso anche il Libano è in cima alle nostre attenzioni, in linea con l'impegno di lunga data dell'Italia nel Paese dei cedri. Le tensioni lungo la Linea blu restano alte; una temporanea cessazione dei combattimenti ridurrebbe i rischi dell'*escalation* e darebbe respiro agli sforzi diplomatici per consolidare le intese parziali e raggiungere un accordo sul confine terrestre con Israele, sulla falsariga di quanto fatto per la delimitazione del confine marittimo. Per questo sosteniamo le iniziative diplomatiche in atto, in particolare quelle dell'inviato speciale degli Stati Uniti Hochstein per ridurre le ostilità e stabilizzare la zona di confine. confine. Ovviamente la stabilizzazione del Libano dipende anche dall'elezione del Presidente della Repubblica. Come sapete, c'è uno stallo. Tocca ai cristiano-maroniti, ma non si trova un accordo all'interno; non si trova l'accordo con Hezbollah, che dovrebbe sostenere anch'essa il il nuovo Presidente. Se non si elegge il Presidente, non si elegge neanche il governatore della Banca centrale libanese, che deve essere sempre un maronita. qualche giorno fa il generale Aoun, capo delle forze armate libanesi, e con lui mi sono confrontato perché anche il ruolo delle forze armate libanesi è importante per la stabilità di quel Paese, anche per far sì che non siano gli Hezbollah l'unico corpo armato, l'unico Come dicevo, noi abbiamo 100 militari italiani, che non sono quelli della missione Unifil, ma sono quelli che addestrano le forze armate libanesi. Fra le manifestazioni più evidenti della crisi fra Israele e Gaza vi sono anche gli attacchi a danno di navi in transito nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Ribelli che dichiarano di agire a favore della causa palestinese. Ansar Allah, i partigiani di Allah, che abbiamo imparato a conoscere come Houthi, sono un gruppo vicino all'Iran, intendono accreditarsi come attori regionali, hanno capacità militari e una strategia politica, per quanto circoscritta. Per le modalità adottate e le capacità militari evidenziate, gli attacchi del gruppo yemenita dimostrano un concreto supporto militare proveniente da attori esterni, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione degli obiettivi e le informazioni per poterli colpire. Le conseguenze degli attacchi si riverberano solo su alcuni Paesi. Il traffico commerciale di Russia e Cina, per espressa dichiarazione degli Houthi, può transitare liberamente da Suez. Si sta quindi creando una situazione di squilibrio competitivo che avrà un forte impatto su di noi e sulle nostre economie. La verità è che siamo già alle prese con un conflitto ibrido globale e il conflitto si gioca contemporaneamente su più fronti in Europa, in Medio Oriente e nel quadrante indopacifico - e tocca più dimensioni: l'accesso alle materie prime, alle fonti di energia, alle terre rare; la capacità produttiva in settori strategici, la superiorità tecnologica; e la competitività economica. La nostra posizione sugli attacchi degli Houthi è stata subito chiara: rappresentano un attacco alla sicurezza e alla libertà della navigazione, un ostacolo al libero sviluppo dei flussi commerciali, un impedimento al regolare funzionamento delle rotte marittime. Sono attacchi inaccettabili, come sono inaccettabili le minacce delle ultime settimane attraverso i mezzi di comunicazione, dirette anche all'Italia. Il nostro Governo ha sottolineato subito, anche a questo Parlamento, la necessità di intraprendere misure urgenti per la soluzione della crisi e per contrastare l'impatto sia economico che politico. Sul piano economico è compromessa la regolarità dei rifornimenti delle merci. L'aumento dei costi ha effetti negativi sul sistema dei trasporti e sul commercio internazionale delle aziende italiane. Siamo un Paese che vive di esportazioni. L'*export* rappresenta il 40 per cento del PIL e il 40 per cento dell'*export* marittimo passa attraverso Suez ed il Mar Rosso. Il volume di interscambio commerciale da e per l'Italia che attraversa il Canale di Suez corrisponde a circa 60 milioni di tonnellate, di cui circa 18 milioni in prodotti petroliferi. Il costo del nolo marittimo è cresciuto in media dell'85 per cento fra gennaio del 2023 e gennaio 2024 e del 25 per cento nella sola settimana dal 4 all'11 gennaio di quest'anno. Siamo di fronte anche a un aumento dei tempi di navigazione, che va da otto a ventuno giorni, con conseguenze sui costi di trasporto, di assicurazione, di servizi e logistica; costi che si riflettono sul prezzo dei prodotti al consumo e che quindi incidono sul portafoglio di tutti i cittadini italiani. I giorni di ritardo pesano sull'impiego delle navi e sul ruolo dei nostri principali porti: Genova, Trieste, La Spezia, Gioia Tauro, Taranto, Brindisi e Napoli. La circumnavigazione dell'Africa rende più conveniente per le compagnie di navigazione utilizzare i porti atlantici come punti di ingresso in Europa, a scapito degli scali italiani. La riorganizzazione delle catene logistiche verso approdi diversi dai porti mediterranei potrebbe diventare duratura. Le conseguenze di questa tendenza sarebbero deleterie non solo per l'Italia, ma per i principali Paesi della regione. Vi è poi il problema legato alla trasmissione dei dati e all'infrastruttura globale di Internet. Attraverso il Mar Rosso passano 16 sistemi di cavi sottomarini che collegano l'Europa all'Asia e quattro sistemi di cavi sono stati recentemente danneggiati. Gli esperti calcolano che un quarto del traffico dati tra Asia ed Europa passa da quei cavi; ciò dimostra la necessità di agire anche per tutelare l'integrità di queste infrastrutture critiche. Noi abbiamo agito immediatamente. L'Italia è stato il Paese che per primo ha deciso di chiedere all'Unione europea di agire, attraverso una missione militare che avesse regole di ingaggio diverse da quelle di Atalanta. Quest'ultima poteva anche essere utilizzata, ma il Governo spagnolo, che ha il comando della missione, ha detto di no. Quindi la missione Atalanta rimane per per garantire la lotta contro la pirateria, mentre la missione che stava nello Stretto di Hormuz non aveva regole di ingaggio che permettessero una difesa attiva, ma serviva soltanto ad accompagnare le navi mercantili. Si è pertanto resa necessaria un'altra missione militare: Aspides. Noi abbiamo insistito perché vi fossero tempi rapidi, ma tutti voi sapete quali sono i tempi delle decisioni comunitarie. Sono servite più riunioni: il Consiglio affari esteri, poi i Ministri della difesa e poi ancora gli esteri. Alla fine siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole, con la partecipazione di più Paesi dell'Unione dell'Unione europea alla missione che oggi dovrà essere approvata da questo Parlamento. Naturalmente abbiamo anche dato il sostegno politico all'operazione difensiva Prosperity Guardian Guardian e abbiamo sostenuto alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. direi che la missione Aspides possa essere considerata un vero successo italiano, perché siamo stati veramente quelli che più di ogni altro l'hanno voluta. Potevamo contare sull'esperienza maturata con la più limitata operazione Emasoh, istituita nel febbraio 2020 al fine di sostenere l'allentamento delle tensioni nel Golfo, con compiti di sorveglianza nello stretto di Hormuz. Aspides ne integrerà le funzioni e i compiti, raccogliendone anche l'eredità in termini di credibilità guadagnata presso gli interlocutori regionali. La nuova operazione agirà nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nel Golfo Persico, con lo scopo di proteggere i nostri traffici contenendo i rischi di *escalation* regionali. Icompiti saranno di natura difensiva. La missione non potrà, cioè, intraprendere azioni di tipo preventivo.

l'ipotesi di valutare eventualmente azioni preventive. Qualora dovessero essere necessarie azioni preventive di tipo militare, nella nostra decisione, se sono azioni preventive, come credo di comprendere, tipo l'allontanamento delle navi e la separazione delle navi, quindi non operazioni belliche preventive, noi questo lo consideriamo possibile. Sono previste mansioni non esecutive, raccolte e scambio di informazioni nelle zone marittime interessate, accompagnamento dei mercantili in transito. Ma la missione avrà anche compiti esecutivi di autodifesa estesa, cioè di neutralizzare attacchi che abbiano come bersaglio diretto navi mercantili scortate e il contrasto ad eventuali tentativi di sequestro delle imbarcazioni. Mi riferisco, ad esempio, alla soppressione di missili o droni in arrivo, come dimostra il caso Caio Duilio che, al momento dell'azione, era in missione nazionale. Le attività esecutive potranno essere svolte soltanto nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, a sud della latitudine di Mascate. Dovrà in ogni caso trattarsi di risposte necessarie e proporzionate, e comunque sempre in mare o nello spazio aereo. In nessun caso, Aspides potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma. Sede del comando operativo è Larissa in Grecia. L'Italia fornirà il comando tattico imbarcato su nave Caio Duilio e il *force* *commander* imbarcato per un periodo di almeno sei mesi, già individuato nel contrammiraglio Costantino. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno, almeno inizialmente, un minimo di tre unità navali. Se il Parlamento chiede al Governo di venire a riferire, ma poi non è interessato, questo è un altro discorso.

Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno, almeno inizialmente, un minimo di tre unità navali, supporto *intelligence* e logistico, capacità di *early warning* aereo, potenziale *cyber*, supporto satellitare e comunicazione strategica. Il contributo italiano è rilevante e si sostanzia nel comando imbarcato, in un cacciatorpediniere, in un velivolo dell'Aeronautica militare, con capacità di sorveglianza, comando, controllo e comunicazioni, in grado di offrire un contributo operativo fondamentale. Aspides, tengo a ribadirlo, non è diretta contro nessuno, ma è a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione. Le risposte saranno condotte nel pieno rispetto del diritto internazionale, di quello consuetudinario e del diritto all'autodifesa in caso di attacco imminente o in corso su navi proprie o di terzi, così come previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. "Aspides" agirà inoltre in piena conformità con la Convenzione ONU sul diritto del mare. L' Unione europea assicurerà il necessario coordinamento sia con l'operazione europea antipirateria Atalanta - di cui abbiamo appena assunto il comando delle forze - sia con l'operazione Prosperity Guardian, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni. Credo in ogni caso che alle operazioni navali nell'area vada affiancata una sostenuta azione di coinvolgimento diplomatico dei Paesi della regione, per convincere anche quelli più restii a collaborare. Gli obiettivi comuni restano: stabilità, *de-escalation* e sicurezza. Assieme ai colleghi europei, abbiamo definito i possibili destinatari della nostra azione di sensibilizzazione. I primi incontri a livello tecnico si sono già svolti. Non escludiamo convergenze con altri attori non europei che possano aprire la strada a collaborazioni nelle operazioni della missione. Stiamo tutelando un bene pubblico globale. Proteggere il commercio internazionale significa fare gli interessi dell'Europa e dell'Italia. Per questo motivo è fondamentale che l'operazione abbia sufficienti contributi di personale e assetti, per poter svolgere i propri compiti con successo. L'Italia fa, come sempre, la sua parte. La crisi nel Mar Rosso e la risposta che abbiamo deciso a Bruxelles rappresentano un banco di prova importante per una difesa europea più efficace. L'esperienza del conflitto in Ucraina (dove manderemo un nuovo magistrato presso la missione europea di EUAM Ucraina), la crisi in Medio Oriente e gli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso hanno messo in evidenza questa necessità. Dobbiamo andare avanti senza esitazioni verso un'autentica difesa europea. Le sfide che abbiamo di fronte sono troppo importanti per poter rinviare ancora questo passo fondamentale. Solo uniti potremo proteggere davvero i nostri cittadini. Le crisi che stiamo attraversando dimostrano anche la crescente necessità di agire con urgenza e flessibilità. La delibera missioni internazionali è stata inviata alle Camere con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi chiediamo oggi a quest'Assemblea di approvare una risoluzione *ad hoc* per autorizzare l'avvio delle nuove missioni. Occorre però trovare una soluzione strutturale e dotarci di uno strumento che consenta una risposta adeguata, rapida ed efficace alla repentina evoluzione del quadro internazionale. La legge n. 145 del 2016 presenta evidenti criticità. Per questo abbiamo trasmesso al Senato una proposta di riforma. L'obiettivo è snellire le procedure di autorizzazione delle missioni per rispondere meglio alle rapide evoluzioni del contesto internazionale, preservando prerogative e ruolo centrale del Parlamento. di ringraziare ancora una volta le nostre Forze armate

per difendere la causa della pace, della giustizia e della libertà. *(Applausi)*.

mediante l'effettuazione di ispezioni,

è sotto gli occhi di tutti come il contesto geopolitico che è stato illustrato dal Ministro sia estremamente critico, dall'Ucraina, passando per il massacro del 7 ottobre per mano di Hamas, al contrasto tra Israele e Hamas per arrivare alle condizioni estremamente tragiche dal punto di vista umanitario della Striscia di Gaza, fino alla crisi del Mar Rosso. Il ministro Tajani ha illustrato con dovizia di particolari l'impegno dell'Italia, delle Forze armate e della Croce rossa internazionale per alleviare la sofferenza dei palestinesi e noi ci riconosciamo in questo sforzo doveroso, che rende ancora una volta le nostre Forze armate protagoniste, insieme al terzo settore, di un'azione assolutamente importante. Anche il richiamo ai "due popoli, due Stati" ci vede d'accordo, pur non potendo ignorare le difficoltà per Israele di avere un interlocutore, perché è evidente che l'interlocutore non può essere Hamas, che c'è una perdita di *leadership* da parte dell'Autorità Tutti noi auspichiamo che i Paesi arabi moderati si impegnino per restituire forza e autorevolezza all'ANP. Quindi, la situazione è più complessa di come qualche volta i *media* italiani la rappresentano. In ogni caso, veniamo alla crisi nel Mediterraneo. Chi sono gli Houthi è stato spiegato: si tratta di una milizia sciita che per un decennio ha combattuto la guerra civile dello Yemen. Si tratta di milizie finanziate, secondo alcuni anche addestrate, dall'Iran e quindi non vi è chi non veda come vi sia quantomeno se non un'alleanza palese, sicuramente una convergenza di interessi tra l'Iran e la Federazione russa, il tutto con con la finalità di destabilizzare il Medio Oriente, di indebolire l'Europa e l'Occidente. Quella nel Mar Rosso è una guerra ibrida che rischia di marginalizzare il Mediterraneo, di imporre nuove rotte commerciali e abbattere intere economie. economie. In questo intervento vorrei analizzare due dinamiche, quella economica e quella strategico-militare. Parto dalle ricadute economiche della crisi nel Mar Rosso. Intanto, oltre l'80 per cento dei beni scambiati sul pianeta si muove su nave, quindi la libertà di navigazione è sottoposta ad una minaccia globale. globale. Quello che sta accadendo rappresenta una palese violazione del diritto internazionale. La crisi di Suez significa viaggi più lunghi, spedizioni più costose, prezzi finali più alti. L'Italia rischia di subire, come l'Europa, ingenti danni. D'altronde, circumnavigare l'Africa significa anche lasciare a bocca asciutta scali importanti come Genova, Gioia Tauro e Trieste. Per un Paese come il nostro, che è un Paese trasformatore e che vive di *import*-*export*, questo ha ricadute veramente drammatiche. È stato calcolato che il valore dell'*import-export* italiano che ogni anno transita per Suez è pari a 148 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo, l'Unione europea ha deciso giustamente di intervenire, avviando l'operazione di sicurezza marittima Aspides. Il generale Camporini ha giustamente sottolineato un certo ritardo, che ha ricordato anche il Ministro nel suo intervento, tra il primo attacco degli Houthi, l'11 dicembre, e l'intervento che è datato, se non erro, 19 febbraio. Ma, certo, ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso è una priorità e noi non abbiamo tempo tempo da perdere. Vengo all'analisi delle conseguenze sul piano strategico e militare. L'Italia nell'operazione Aspides ha un ruolo importante. È quindi stato affidato e riconosciuto alle donne e agli uomini della Marina militare un ruolo molto significativo, come meritano. Le nostre Forze armate, d'altronde, sono molto apprezzate e anche le fregate italiane sono moderne e all'altezza. A differenza, però, di quanto deciso dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, abbiamo scelto un'azione difensiva in forma passiva. Noi ovviamente ci riconosciamo in questa scelta riteniamo che sia improntata alla prudenza, ad evitare in ogni modo l'*escalation*. Chiediamo tuttavia al Governo di valutare e, ovviamente, calibrare la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi. Vengo ad un ultimo aspetto. Il ministro Tajani ha dichiarato che Aspides è un primo passo verso la difesa comune europea. noi auspichiamo, signor Ministro, che ci sia da parte dell'Italia la comunicazione all'Unione europea del senso dell'urgenza e soprattutto del tempo che l'Europa ha colpevolmente perso nell'attesa di definire una una difesa comune. Questo significa qualcosa anche all'interno di questa missione, perché accanto a Paesi come l'Italia, la Francia e la Germania, che hanno aderito alla missione Aspides, ci sono Paesi come la Spagna e l'Irlanda che hanno fatto scelte diverse. Questo rimanda alla necessità e all'urgenza di una difesa comune. Noi non solo non ci scandalizziamo, ma auspichiamo che si tenda a quel 2 per cento del PIL da spendere in difesa, come chiede la NATO, perché questo è un nostro dovere. Nessuno è guerrafondaio, ma non possiamo ignorare le sfide che abbiamo di fronte e la necessità di affrontarle con i giusti mezzi. Quello che auspichiamo, e concludo, è che l'Italia sia in prima linea per giocare al meglio questa partita in Europa. Sicuramente noi, come Azione, dai banchi dell'opposizione, facciamo il tifo per l'Italia.

Signor Presidente, a seguito degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre e della conseguente operazione militare dell'esercito israeliano a Gaza, nel Mar Rosso si è registrata una situazione di crescente instabilità per mano degli Houthi, che sono un gruppo islamico di fede zaydita sciita, emerso tra gli anni Ottanta e Novanta in contrapposizione con il Governo sunnita, fortemente influenzato dall'Arabia Saudita, che nel 1962 aveva rovesciato l'imamato zaydista. Attualmente, la maggior parte della popolazione yemenita è di fede sunnita, sebbene in alcune zone del Paese prevalgano gli sciiti. Nel tentativo di individuare attori esterni che supportassero la loro causa, gli Houthi guardarono al principale Paese di fede sciita della regione, l'Iran, che era interessato a contrastare l'espansione dei musulmani sunniti e iniziò quindi ad appoggiare le rivendicazioni degli Houthi, divenendo uno stabile alleato ideologico, religioso e militare. Già dalla prima metà degli anni Duemila gli Houthi in Yemen si scontrarono più volte con le autorità nazionali, sempre fortemente influenzate dalla sunnita Arabia Saudita, rivendicando autonomia religiosa e politica, e ciò sfociò nel 2014 nell'avvio della vera e propria guerra civile. Gli Houthi hanno dato vita all'organizzazione armata Ansar Allah, che risulterebbe fatta di circa 20.000 combattenti e ad oggi controlla la maggior parte del territorio a ovest dello Yemen, circa un terzo del territorio complessivo dello Stato, inclusa la capitale Sana'a

ha infatti affermato che le sue forze erano pronte a muoversi in centinaia di migliaia per unirsi al popolo palestinese e confrontare il nemico. Dopo il 7 ottobre, per rappresaglia, dallo Yemen sono stati lanciati diversi missili verso Israele. Dal mese di novembre hanno iniziato a verificarsi degli attacchi missilistici e controlli sulle navi mercantili che attraversano il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Il 18 dicembre gli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity Guardian, dichiarando che non sarebbero restati a guardare dinanzi a ulteriori attacchi e che gli Houthi ne avrebbero subito le conseguenze. Non sono state compiute operazioni dirette fino al 31 dicembre, quando gli elicotteri della marina statunitense hanno sparato su un gruppo di piccole imbarcazioni che tentavano di avvicinarsi e imbarcarsi su una nave *container,* che ha per questo richiesto l'aiuto USA. L'attacco americano ha portato alla morte di 10 miliziani Houthi che, come rappresaglia, hanno lanciato missili e attacchi con droni verso alcune imbarcazioni americane il 9 gennaio. Stati Uniti e Regno Unito hanno abbattuto i 21 attacchi degli Gli inglesi hanno riferito che i droni usati dagli yemeniti erano di *design* iraniano, un fatto che non sorprende in virtù della già menzionata alleanza militare tra i due attori. All'operazione Prosperity Guardian hanno aderito il Canada, il Regno Unito, la Norvegia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Francia e la Grecia, le Seyschelles, Sri Lanka, Singapore, l'Australia e il Bahrain che funge da base. Anche l'Italia ha ufficializzato la partecipazione mediante l'invio della fregata multimissione Virginio Fasan, per contribuire ad aumentare la presenza nell'area, al fine di garantire il principio di libera navigazione. L'area geografica dove si stanno verificando questi episodi è fondamentale per le rotte strategiche del commercio marittimo. Il Mar Rosso è una delle principali arterie mondiali, dalla quale passa un terzo del traffico di *container* del mondo. Il fatto che gli Houthi abbiano sfruttato la vulnerabilità del collo di bottiglia naturalmente rappresentato dagli stretti, rendendo pericolosa la navigazione, ha avuto l'effetto, come anticipato, di dirottare molti traffici su rotte più lunghe e costose: passare per il Corno d'Africa comporterebbe fino a un milione di dollari di maggiori spese solo per il carburante. Basti pensare che un cargo da Singapore a Rotterdam impiegherebbe circa dieci giorni in più di navigazione per raggiungere la destinazione. I danni per l'economia mondiale potrebbero essere catastrofici. Basti pensare a quando, nel 2021, una nave incagliata nel Canale di Suez determinò, per i sei giorni in cui rese la rotta inutilizzabile, un blocco dal valore di 10 miliardi di dollari per ogni giorno. Ciò sta già avendo un impatto visibile su alcune catene di approvvigionamento colpite da ritardi nelle forniture di materie prime per i semilavorati e prodotti finiti. Come riferisce Mario Sechi dalle pagine di «Libero», Tesla e Volvo hanno sospeso la produzione di auto in Europa per l'assenza di componenti. Sechi ricorda anche che per l'Italia il Canale di Suez vale il 40 per cento dell'interscambio marittimo, pari a 82,8 miliardi di euro. Basti pensare, come riferito da Coldiretti, che le destinazioni interessate sono quelle asiatiche, verso le quali nel 2022 l'Italia ha esportato oltre 217 milioni di chili di frutta, di cui oltre 182 milioni di chili di mele, con principali destinazioni Arabia Saudita, India ed Emirati arabi. Ci sono preoccupazioni anche per il vino, con le esportazioni *made in Italy* che valgono 112 milioni di euro in Cina. Il blocco del Mar Rosso mette dunque a rischio l'esportazione del *made in Italy* in Cina, che per il solo settore agroalimentare vale oltre 570 milioni di euro l'anno, di cui oltre il 90 per cento viaggia proprio su nave. Il prezzo del petrolio è aumentato del 4 per cento, raggiungendo gli 80 dollari al barile. La crisi avrebbe fatto crollare il traffico di merci mondiale di quasi il Nell'incidere sul prezzo delle materie prime energetiche, la situazione potrebbe determinare un aumento dei costi dell'energia e quindi dell'inflazione. Anche i nuovi aumenti dei costi di spedizione globale potrebbero aumentare l'inflazione dei prezzi al consumo nei prossimi mesi. A seguito della situazione di instabilità del Mar Rosso che sta determinando forti ripercussioni sul transito di navi *container* e, di conseguenza, sulle catene di approvvigionamento, si è iniziato a discutere dell'ipotesi di istituire una missione europea finalizzata a ripristinare la stabilità e la sicurezza di un tratto di mare fondamentale per il commercio internazionale. Il 22 gennaio è stato concordato in linea di principio l'avvio della missione nel Mar Rosso denominata Eunavfor Aspides. Dopo una prima definizione di alcuni dettagli operativi alla riunione dei Ministri della difesa dell'Unione del 30-31 gennaio, il Consiglio affari esteri del 19 febbraio ha adottato la decisione formale sull'avvio della missione: l'Italia avrà il comando delle Forze della missione navale. Il Governo Meloni ha condannato le attività criminali degli Houthi sulle imbarcazioni in transito nel Mar Rosso, adoperandosi tempestivamente per individuare soluzioni atte a ripristinare la sicurezza di tale area di mare e garantire la libertà di navigazione. L'Italia è stata da subito in prima fila per dialogare con i Paesi, come Francia e Germania, intenzionati ad attivarsi per assicurare il transito sicuro dei mercantili, tanto che il documento presentato a inizio anno dal Consiglio affari esteri è proprio su iniziativa di Roma, Parigi e Berlino. Per l'Italia, la rotta navale interessata è di rilievo primario, in quanto per Suez transita circa il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo. L'iniziativa è ritenuta urgente e su di essa ci si aspetta e si auspica compattezza anche in Patria, senza sterili opposizioni che non farebbero gli interessi economici e politici del nostro Paese. Difendere i mercantili italiani, assicurare la libertà di navigazione sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - la Convenzione UNCLOS di Montego Bay dal 1982, è un impegno che questo Governo vuole portare avanti con serietà. Per questo motivo l'Esecutivo si è impegnato in prima fila con i principali *partner* europei per la celere definizione degli aspetti operativi della missione Aspides e per il suo pronto avvio. Essa avrà carattere difensivo, dimostrando l'impegno italiano per tentare di arginare una crisi che, se protratta, potrebbe comportare un'impennata nei prezzi delle energie e dei beni al consumo che ricadrebbero sulle famiglie già provate dalle ripercussioni economiche della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi. Il fatto che il comando delle forze di Aspides sia stato affidato all'Italia è un ulteriore riconoscimento dell'impegno del Governo Meloni, conferma la fiducia riposta nel nostro Paese e premia la competenza e la professionalità della Marina militare, un'eccellenza nazionale, come tutto il comparto della Difesa. *(Applausi)*. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

Ci limitiamo ad allargare la riflessione molto puntuale sui fatti esposti dal ministro Tajani a una qualche considerazione anche politica, con cinque punti molto rapidi. la Caio Duilio ha fatto l'interesse del nostro Paese *(Applausi)* e chi oggi ne mette in discussione la legittimazione non si rende conto di cosa dice. arriva un drone contro una nave militare, non si può dire: non abbiamo ancora l'autorizzazione del Parlamento, datemi il telefonino del Presidente del Senato o del Presidente della Camera. Siamo in presenza del primo atto di guerra da anni contro le nostre navi militari e di una polveriera internazionale. Il Parlamento deve solo dire grazie alle donne e agli uomini delle Forze armate *(Applausi)* che difendono la nostra Costituzione, oltre che la nostra Patria. Secondo punto: la vicenda del Mar Rosso segna, amici e colleghi sovranisti, la dimostrazione più evidente che il vostro ragionamento non sta in piedi. Il Mar Rosso è, per definizione, la dimostrazione che l'Italia ha bisogno di globalizzazione ed internazionalizzazione e il fatto che noi interveniamo e siamo e siamo favorevoli a intervenire nel Mar Rosso è il modo più efficace per difendere la nostra sovranità. Dal Mar Rosso passano le merci Dal Mar Rosso passano le merci e il futuro dei nostri porti. Nel momento infatti in cui si deve circumnavigare l'Africa, è evidente che poi si arriva a Rotterdam e non nei porti dove, in questo momento, anche amministratori di colori diversi dal nostro stanno facendo molto bene. Penso a Gioia Tauro, al presidente Occhiuto, a Taranto e a Genova. In questa cornice, difendere l'interesse nazionale significa avere una visione globalizzata del mondo. Passano i cavi, passa il futuro di riscatto del Sud e del Mezzogiorno, passa un tema di cui non parla nessuno, che è quello della maggiore esigenza di approvvigionamento energetico. si parla di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale non starà in piedi senza una quantità di energia incredibile e, se noi non approvvigioniamo l'Italia con l'energia che passa dal Mar Rosso, noi non saremo in grado di fare nessun tipo di scommessa sui rigassificatori di Porto Empedocle, di Gioia Tauro, di Piombino o persino di Ravenna. in questa cornice, il Mar Rosso è davvero casa nostra. Altro che sovranismo da tre soldi. Terza considerazione politica: le battutine che in questo Parlamento, anche da membri del Governo, ho sentito fare anche in questa legislatura, sulle *leadership* dei Paesi arabi riformisti, a cominciare da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oggi lasciano il tempo che trovano. È del tutto evidente infatti che chi, come chi vi parla, da anni sottolinea l'importanza di difendere le *leadership* moderate nei Paesi arabi contro gli estremisti islamici che vogliono la *jihad* globale, di cui gli Houti sono una parte;

si sono affrontate due diverse filiere di pensiero. C'era chi diceva che siamo in presenza di uno scontro di civiltà e voleva dire tutti contro il mondo islamico (visione stupida e sbagliata) e chi da tanti anni sta cercando di dire che, se vogliamo affrontare il rischio dell'estremismo islamico e della *jihad* globale, bisogna allearsi con i *leader* riformisti arabi. E questo è avvenuto quando nel silenzio si facevano le battutine su quello che stava succedendo in Yemen, che qualcuno portava all'attenzione, perché Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti intervenivano in quell'area, difendendo anche noi. Ma era impossibile dirlo, perché si portavano i dromedari nei gazebo, per fare ironia contro gli avversari politici. Questa è la dimostrazione, caro Presidente, della diversità che c'è tra chi fa politica parlando di politica estera e chi si limita alle battutine contro gli avversari, non capendo niente di quello che sta accadendo nel mondo oggi. Un *leader* di quel mondo mi disse una volta, quando ero al Governo: vedi, Matteo, noi stiamo vivendo tra sunniti e sciiti, quindici secoli dopo la nascita del profeta Maometto, esattamente quello che è successo nel mondo cristiano, tra Medioevo e Rinascimento, tra cattolici e protestanti. Io non so se questa lettura storicamente possa essere condivisa o meno. È interessante; ma quello che so è che la divisione non è tanto tra sunniti e sciiti, ma è tra coloro i quali credono in un mondo globale che rispetti la diversità delle visioni religiose e chi invece vuole imporre, alle Torri Gemelle come al Bataclan, come nelle città europee, la guerra santa per il tramite dei finanziamenti degli estremisti. Questo è l'argomento di cui qualcuno da mesi sta discutendo e di cui probabilmente vi sarebbe bisogno di parlare di più. cosa c'è di più sterile di chi fa le battutine sugli avversari rispetto agli *slogan*? Dividersi tra quelli che dicono *peace and love*, pace e amore, non abbiamo bisogno di armi perché la pace si fa con la diplomazia - argomento che probabilmente non troverebbe il consenso dei partigiani, che con le armi hanno liberato l'Italia dal nazifascismo

con il Risiko. Sono due opposti estremismi che vanno rigettati al mittente. È Roma la città nella quale si diceva «*si vis pacem, para bellum*». direzione - è fondamentale per il futuro delle istituzioni di Bruxelles, ma contemporaneamente serve la politica estera, perché, se nella politica estera ci limitiamo a frasi di circostanza e a discorsi retorici privi di politica, non andremo da nessuna parte. Il mondo di oggi è una polveriera, a partire dalla Corea del Nord, che questa mattina ha annunciato di replicare alle iniziative congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, fino a quello che sta accadendo nei Paesi africani, dove è giusto fare il Piano Mattei, ma diciamo anche le cose come stanno: abbiamo già perso la battaglia in Africa, se i beni materiali e le materie prime sono totalmente in mano ai cinesi e la Wagner, guidata da Putin, riesce a fare quello che crede all'interno di alcuni Stati. Questo è l'argomento su cui dovremmo discutere: tenere insieme un esercito europeo e una politica estera europea, tenere insieme una forte capacità di investire nell'armamento - perché bisogna armarsi in questo mondo - con la voglia di dire che noi facciamo politica e quindi cerchiamo di affrontare e di risolvere i problemi con la politica e con la diplomazia. La guerra non è La guerra non è una forma di prosecuzione della politica con altri mezzi, come diceva von Clausewitz; è, al contrario, la negazione della politica. Infine, caro Ministro, noi siamo con lei, siamo con il Governo, siamo dalla parte dell'Italia. Da che mondo è mondo, la politica estera deve unire, non dividere. È vero che viviamo in un tempo nel quale, paradossalmente, la politica estera divide le coalizioni, a destra come a sinistra. Ed è un paradosso, perché nella storia italiana, da sempre, la politica estera è stata l'elemento che ha unificato i Governi: Nenni, Berlinguer che fa l'intervista famosa sul Patto Atlantico, dicendo che si sente più sicuro da questa parte del mondo. Eppure, oggi noi abbiamo una situazione complessa. Signor Ministro, lei rappresenta tutti noi. Sia all'altezza di questo compito. Le battutine di oggi, rispetto al Parlamento, se è interessato o meno, se le risparmi, perché ella oggi ha una grande responsabilità. Sia all'altezza del ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. Buon lavoro a lei,

la partecipazione dell'Italia alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ucraina e di autorizzare la missione Levante nell'ambito del conflitto tra Israele ed Hamas, purché la difesa italiana non operi a favore della marina libica e purché le azioni di rafforzamento sulla presenza nel Mediterraneo orientale ricadano negli scopi umanitari. Chiediamo, invece, di non autorizzare la nuova missione Aspides all'interno della missione che proroga l'impiego di un dispositivo per la presenza, la sorveglianza e la sicurezza nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano indiano nord occidentale. Io mi concentrerò, in particolare su quest'ultima, ma voglio fare una premessa, che può sembrare, signor Ministro, solo di metodo, ma che invece è di sostanza. E lo è ancora di più in una condizione come questa, quando il mondo sembra, ogni giorno che passa, sempre più precipitare nell'incubo di una guerra globale. Noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra riteniamo del tutto insoddisfacente il coinvolgimento di questo Parlamento. Abbiamo rischiato di discutere questa missione senza nemmeno passare per le Commissioni parlamentari. Solo in virtù delle prese di posizione delle forze di opposizione abbiamo guadagnato qualche ora, perlomeno per permettere ai Gruppi di confrontarsi su una questione molto delicata che, seppure venga presentata come operazione puramente difensiva, contiene invece molti elementi di ambiguità o perlomeno di forte preoccupazione. Il Parlamento, a nostro avviso, non è stato sufficientemente e tempestivamente coinvolto. Questo ci sembra molto grave, a maggior ragione per il coinvolgimento rilevante, rilevantissimo, della Marina militare italiana e nonostante il rischio concreto che il nostro Paese possa rimanere coinvolto in una *escalation* militare decisa altrove. Peraltro, stiamo parlando, vorrei che fosse chiaro, di una missione che non può essere considerata come una semplice espansione della missione Atalanta, che si sta svolgendo nel Mar Rosso e che ha una natura diversa, innanzitutto perché, differentemente da questa, inserita all'interno di un quadro ONU, sulla base cioè di risoluzioni del Consiglio di sicurezza. missione, quella, diretta esclusivamente alla scorta dei convogli del programma alimentare mondiale e al contrasto della pirateria e del traffico di droga e di armi; quindi, rivolta alla prevenzione di fatti di criminalità di criminalità e non di un conflitto militare internazionale a rischio *escalation* come quello in corso. La missione Aspides, nonostante venga presentata fin dal nome come una missione difensiva, rischia però sul campo, in un contesto di guerra, di cambiare natura e determinare una ulteriore *escalation*. Tale rischio ci sembra colpevolmente trascurato dal Governo italiano e anche da questo dibattito parlamentare, non solo relativamente a questo contesto, ma più in generale nella fase di instabilità che il mondo vive ormai da qualche anno a questa parte. Valeva in passato, e vale ancora oggi, per il conflitto in Ucraina; vale ancor di più per il conflitto in Medio Oriente: due conflitti diversi, che sarebbe improprio assimilare, ma che hanno in comune la stessa rinuncia della comunità internazionale a cercare soluzioni diplomatiche per risolvere la crisi, nella convinzione fallace che solo il ricorso alle armi sia sufficiente per ricercare soluzioni. Eppure, la questione Ucraina avrebbe dovuto consigliare un altro approccio dopo i clamorosi errori di valutazione che continuano a segnare la strategia o meglio l'assenza di strategia dei Paesi occidentali. Si è parlato in quel caso di rapida conclusione della guerra, del sicuro successo di una controffensiva che invece non è stato tale, di un possibile collasso economico della Russia, dell'imminente caduta di Putin. Nessuno di questi scenari si è avverato, mentre continuano morte e distruzione. Noi ve l'abbiamo detto più volte in quest'Aula *(Applausi)*: non era in discussione la solidarietà all'Ucraina, ma come favorire soluzioni efficaci e non propagandistiche. La rinuncia dell'Europa a svolgere un ruolo prettamente politico ci pare ancora una volta il tema principale e vale anche oggi che discutiamo della missione Aspides. In Yemen - è stato ricordato - c'è una guerra civile in corso da dieci anni che qui è stata rappresentata in maniera totalmente sottostimata e senza nessuna evidenza mediatica. Eppure parliamo di un conflitto che ha provocato migliaia di morti, che ha costretto 4 milioni di persone a lasciare le proprie case, che ha consegnato 11 milioni di bambini all'assistenza umanitaria. Questo mentre, a proposito del commercio internazionale di armi, imprese anche italiane hanno rifornito per anni la coalizione a guida saudita che bombardava anche i civili, agendo come fornitrici dirette o appaltatrici. In questo contesto, l'operazione Aspides nel Mar Rosso avrebbe il mandato di accompagnare le navi mercantili e proteggerle dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, ma si tratta di una missione che presenta perlomeno una serie di aspetti problematici, non solo perché non si può considerare esclusivamente difensiva, tanto è vero che le regole d'ingaggio non escludono che la risposta a un attacco possa colpire le basi nelle coste yemenite, ma anche perché la missione prevede una esplicita connessione con l'operazione Prosperity Guardian, a guida americana, a tutti gli effetti un'operazione militare che comprende e contempla possibili incursioni sul territorio yemenita e attacchi preventivi contro obiettivi Houthi. Una missione peraltro priva, questa, di un mandato delle Nazioni Unite, che avviene senza che sia stata tentata una strada politica e diplomatica che protegga realmente la navigazione. Noi crediamo che il rischio *escalation* sia molto alto, a maggior ragione alla luce dei bombardamenti statunitensi che hanno recentemente colpito obiettivi in Iraq con una evidente violazione di sovranità; una *escalation* che può favorire un ulteriore allargamento globale del conflitto, senza risolvere le ragioni della destabilizzazione dell'intera regione, che evidentemente vede nella questione di Gaza l'unica possibile chiave di stabilità. Si torni a svolgere un ruolo politico; si cerchi di fermare l'orrenda strage di Gaza per aprire i valichi, per togliere l'assedio alla Striscia; si faccia cessare il fuoco: questo dovrebbe fare la politica e noi crediamo che questo dovrebbe fare il nostro Paese.

a consumare un passaggio che ci rammenta la centralità del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali, né tantomeno dobbiamo semplicemente esprimerci su nuovi e necessari impegni militari del nostro Paese. Questo voto, specie per quanto concerne la missione Aspides, segna uno spartiacque tra un prima e un dopo. È una *sliding door* tra un'Unione europea inerte che affida i suoi destini in mani altrui e un'altra Europa che, pur in formato ristretto, assume consapevolezza e prende in mano il proprio futuro; fa attrice e diventa forza anche militare e dà una risposta concreta a minacce concrete, difendendo quindi i suoi interessi e garantendo il principio della libertà di navigazione. Basterebbe questo assunto, questa prospettiva di un'Europa che con Aspides diventa protagonista e che deve necessariamente costruire una sua prospettiva di autonomia strategica militare, in sinergia e in concerto con i suoi alleati (penso alla NATO), per dare un sostegno convinto alle determinazioni dell'Esecutivo per le missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel corso di quest'anno rispettivamente in Medio Oriente, nel Mar Rosso e in Ucraina. Ma, se ciò non bastasse, se pensassimo erroneamente che questo orizzonte non ci appartiene, l'attacco terroristico degli Houthi yemeniti - che, ricordiamolo, sono di fatto una milizia filoiraniana - verso una nostra imbarcazione militare, dimostra ancora una volta la necessità di un nostro impegno diretto. È in questo scenario, in un *front test* più che mai inquieto e in un'area mediterranea attraversata da venti di instabilità e che purtroppo non sono destinati a placarsi in breve tempo, che dobbiamo sviluppare ogni nostra riflessione e progettare il nostro impegno. Lo spirito dei tempi prevede che difendersi in armi non sia più un'opzione remota; tutti siamo coinvolti in scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili, anche agli analisti più spericolati. È pertanto necessario che le nostre missioni siano in grado di rispondere ancor meglio ai nuovi contesti e alle rapide evoluzioni che non smettono di susseguirsi. Viviamo in una fase storica il cui il tempo della risposta è tanto importante quanto la risposta stessa. Non è un caso se nelle scorse settimane si è discusso sui tempi europei del varo di Aspides, su come la reazione sia maturata in ritardo rispetto agli avvenimenti che si consumavano nell'area del Mar Rosso. È vero, i tempi di reazione non sono stati ottimali, ma ciò dimostra ancor più quanto sia importante e necessaria questa scelta e quanto dobbiamo lavorare per dare vita a un esercito europeo, a un meccanismo democratico efficace e tempestivo per rispondere alle sfide che si presentano e che, in un contesto internazionale turbolento, continueranno a presentarsi sempre più frequentemente. Al pari, qualcuno in casa nostra ha criticato questo nostro impegno internazionale, richiamando le determinazioni della Spagna, la sua scelta di non inviare né uomini né mezzi. Non giudico le decisioni dei Paesi amici e sovrani che reputo legittime; ognuno si regola come meglio crede e secondo i propri interessi, ma in casa nostra, in quest'Aula, come nel Paese, non è consentito a nessuno utilizzare doppi registri, attingere a una stantia retorica pacifista e profittevoli distinguo, indugiando nell'equivoco e magari indebolendo nell'opinione pubblica questa missione, il cui fine - lo ricordo - è garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta dell'ONU. Onorevoli colleghi, membri del Governo, l'Italia non ha scelta. Non esiste un dubbio, oltre che un motivo valido, se spendersi o meno, in missioni internazionali. Siamo un Paese immerso fino al collo nel Mediterraneo, siamo parte di questo mare e in questo mare si giocano i nostri destini e i destini di un'Europa che finalmente, anche grazie all'impegno e all'azione di questa maggioranza e di questo Esecutivo, si è ridestata e ha rivolto lo sguardo a Sud, all'Africa profonda, alle realtà rivierasche di questa sponda piuttosto che all'area del Mar Rosso. Questa è l'Europa che vogliamo, che serve, per cui occorre spendersi. Tutto ciò ha un costo, è vero. Significa in primo luogo impegnarsi, anche militarmente, con i rischi e con i costi che tale impegno comporta, ma dobbiamo sapere che oggigiorno non esistono più pasti gratis. Nessuno, anche per l'effetto crescente e perverso delle proprie opinioni pubbliche, è più disposto a spendersi in cause altrui, o meglio in scenari che i propri cittadini reputano distanti e lontani dai propri interessi. Noi, con questi nuovi impegni, agiamo in scenari di nostro primario interesse, agiamo a difesa di rotte commerciali strategiche, rotte vitali per l'Italia, in un'operazione difensiva che si concentrerà sulla protezione delle navi contro gli attacchi in mare. Per questo non dovremmo stupirci se vi saranno nuove aggressioni contro le nostre unità, o nuovi scontri in un contesto come quello del Mar Rosso ad alto rischio. Questi episodi dobbiamo metterli in conto: sono la reazione a una scelta obbligata della comunità internazionale di cui facciamo convintamente parte, che ha dovuto schierare la propria forza nell'area, ancora una volta a difesa delle ragioni del diritto e in funzione della pace. Sono interessi plurimi, che rispondono a ragioni tanto geopolitiche che economico-commerciali, tanto le prime quanto le seconde sono evidenti a tutti. Desidero però richiamare i dati forniti da Confartigianato, che testimoniano l'impatto della crisi del Mar Rosso sul nostro sistema economico e produttivo, una crisi che genera danni per 95 milioni di euro al giorno, per un totale di 8,8 milioni di euro accumulati tra novembre 2023 e gennaio 2024, di cui 3,3 miliardi (35 milioni al giorno) dovuti alle mancate esportazioni e circa 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri. Mi chiedo come possa l'Italia, la cui quota di *export* manifatturiero diretto nei Paesi extraeuropei è pari al 32,7 per cento del totale dell'area (il doppio delle imprese tedesche), non spendersi in questa crisi; come può un Paese, che nel 2023 ha avuto 1,5 punti di PIL derivati dal flusso di *import*-*export* di merci nel settore del *made in Italy* transitato attraverso il Mar Rosso, non agire e rimanere a guardare. Tutto ciò, senza contare altri fattori di rischio non meno importanti. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte alla nuova frontiera della guerra ibrida, con una guerra sottomarina ai cavi, infrastrutture strategiche sensibili, prede relativamente facili nelle acque del Mar Rosso. La missione Aspides è quindi un paradigma, è una risposta rapida e multilaterale all'attacco a quello che oggi rappresenta il mare: il bene comune globale, che racchiude il maggior numero di minacce e rischi ibridi al mondo. Credo quindi che l'azione del Governo, anche sulla scorta degli impegni approvati dall'Unione europea il 19 febbraio scorso, in occasione del Consiglio degli affari esteri - e ringrazio il ministro Tajani per il grande lavoro svolto - vada nella direzione giusta. Il provvedimento dell'Esecutivo, infatti, muove da basi di realismo e di grande consapevolezza. La stessa idea di favorire una maggiore interoperabilità e una maggior flessibilità nell'utilizzo degli assetti e delle unità di personale all'interno di missioni appartenenti alla medesima area geografica ne è una prova, perché consente di rispondere con maggiore prontezza nell'eventualità di situazioni di crisi e di emergenza. Anche con la missione Levante, su cui spendo qualche parola prima di concludere, l'Italia conferma la sua proiezione internazionale come forza di pace e testimonia la nostra ferma volontà di aiutare la popolazione palestinese, prima vittima degli attacchi terroristici di Hamas, mantenendo salda una prospettiva di pace in Medio Oriente basata sui due Stati. È quindi con convinzione che, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole, esortando tutti noi parlamentari di maggioranza e di opposizione a maneggiare questi temi con grande responsabilità,

Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, stiamo per votare delle proposte di risoluzione che autorizzano tre nuove missioni internazionali che impegnano il Governo a perseguire la tutela degli interessi nazionali. Dirò subito che il Movimento 5 Stelle voterà a favore delle missioni. Entriamo nel merito della missione Aspides, quella che nel Mar Rosso è istituita per la difesa delle navi nella rotta commerciale più importante per il nostro Paese. Avevamo alcuni dubbi: il testo proposto inizialmente non chiariva a sufficienza e non ci rassicurava sul fatto che le nostre Forze armate fossero chiamate ad effettuare o meno operazioni sul suolo yemenita o che che potessimo essere parte attiva e belligerante contro gli Houthi in Yemen. Un conto è abbattere droni, come ha fatto qualche giorno fa la nave Duilio, un altro è prendere l'iniziativa e attaccare postazioni militari in un'altra Nazione. Bene abbiamo fatto ad insistere che venisse tolto quell'avverbio «eminentemente» riferito all'aggettivo «difensivo» che c'era nel testo originale. La nostra richiesta è stata accolta ed è stato chiarito che la nostra missione sarà difensiva. Nessuno avverbio. Saranno messe in campo tutte le necessarie misure per difendere le navi, proteggere i cavi di comunicazione sottomarini e il personale delle nostre Forze armate, della nostra Marina in particolare. Ci preoccupava e ci preoccupa l'interazione e la cooperazione con l'operazione *Prosperity Guardian*. Sappiamo molto bene che ci sono stati attacchi al suolo a postazioni militari Houthi da parte della coalizione angloamericana. Questo, a parer nostro, può innescare un'*escalation* militare in una parte del mondo già martoriata. Sappiamo che la motivazione che gli Houthi danno al proprio operato è la situazione a Gaza contro Israele. Vengo quindi alla seconda missione, per cui esprimiamo nuovamente il parere favorevole: la missione Levante. Va molto bene inviare assetti e aiuti umanitari e una nave ospedale e se fosse possibile aumentare questo tipo di aiuti, noi saremmo disponibili. Non possiamo, però, da una parte aiutare le popolazioni civili colpite dalla guerra e dall'altra parte non fare nulla per fermare il Governo israeliano e il suo primo ministro Netanyahu che quella guerra, invece, non intende fermarla. *(Applausi)*. Ma come si fa a chiamare diritto di difesa e a pensare che sia una cosa giusta che Israele ponga in atto una carneficina come quella di pochi giorni fa, sparando tra la folla che cercava solo di accaparrarsi il cibo? Come può essere giusto quel diritto di difesa se il risultato è la morte di migliaia di persone? Ribadisco: se il risultato è la morte di bambini, giusto o sbagliato che sia il vostro punto di vista, la guerra va fermata immediatamente. bene gli aiuti ai civili palestinesi, ma invito il Governo ad essere più concreto e meno accondiscendente con Israele. Dica forte e chiaro in tutte le sedi che Netanyahu si deve fermare. Gli sforzi umanitari vanno bene, ma fermiamo la causa e, signor Ministro, facciamo ogni sforzo possibile per riportare alle proprie famiglie gli ostaggi che Hamas ancora detiene. La terza missione, per cui esprimo il voto favorevole da parte del MoVimento 5 Stelle, è relativa alla cooperazione con l'Ucraina per il miglioramento e lo sviluppo di servizi di sicurezza, lo sviluppo dello Stato di diritto e per la lotta alla corruzione, per cui impegniamo la nostra magistratura in una collaborazione utile e lungimirante. Di questo vi diamo atto. considerazione, signor Ministro. A breve, avremo il comando tattico operativo praticamente di tutte le missioni nel Mediterraneo, quindi sarete in grado di operare direzione e controllo. Di ciò che accade o accadrà dovrete informare questo Parlamento e coinvolgerlo. Signor Presidente, abbiamo chiesto poche cose al Governo, nella nostra risoluzione, e ve le voglio ricordare: profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco; di farsi promotore di una forte azione diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti il riavvio di un processo di pace basato sul principio "due popoli, due Stati"; di adoperarsi per ampliare la portata umanitaria della suddetta operazione, considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza; di adoperarsi a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione di civili più vulnerabili, tra cui feriti gravi, bambini e anziani;

lei prima richiamava il Parlamento all'attenzione, ma lei in questo momento sta portando poco rispetto a chi parla e a tutta l'Assemblea. favore, ma il voto favorevole che il MoVimento esprime ora non è una cambiale in bianco. *(Applausi)*. Questo voto favorevole è sulla base di quanto ci è stato assicurato e messo nero su bianco nelle risoluzioni che voi avete accettato. Non esiteremo un solo istante a denunciare qualsivoglia deviazione dalla missione puramente difensiva e a chiedervene conto. link apre una nuova finestra"). Salutiamo in tribuna i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Don Paolo Galliero» da Tribano, in provincia di Padova. Benvenuti in Aula.

alcuni ergono barricate, accusandoci di essere dei guerrafondai, invocando il disimpegno e lasciando emergere un antimilitarismo militante troppo diffuso. Parlare di difesa vuol dire però parlare di migliaia di giovani italiani impegnati nei teatri più caldi per garantire difficili equilibri; vuol dire parlare di persone che con orgoglio e con il Tricolore sul petto garantiscono la nostra sicurezza in Italia e all'estero vuol dire parlare di ragazzi che nelle missioni internazionali operano a favore delle popolazioni locali, come nel caso dei nostri militari che nelle ultime settimane hanno trasportato dei bambini malati da Gaza verso gli ospedali italiani. Signor Ministro, cari colleghi, quando si parla di difesa, si parla anche di loro, dei loro atti di quotidiano e silenzioso eroismo finanche a rischio della loro vita, di una struttura che quando lo Stato lo richiede, risponde sempre presente, dei figli dell'Italia migliore, di chi sacrifica un'intera vita per la Nazione e per la Patria e di chi poi, come nel caso della missione nel Mar Rosso, difende i nostri interessi strategici, che devono essere difesi assolutamente anche lontano dalle nostre frontiere. Il momento di forte competizione globale e il mutato scenario geopolitico ci impongono un attivismo senza precedenti. Le minacce alla libertà di navigazione e al diritto internazionale sono sotto gli occhi di tutti e non volerle vedere sarebbe un errore che rischiamo di pagare a caro prezzo. Confindustria, Confartigianato, Coldiretti e altre associazioni, hanno stimato in diversi miliardi i danni alla nostra economia. I ritardi di consegna delle merci sarebbero insostenibili e qualora questo problema non venisse risolto nel breve tempo e le rotte commerciali continuassero a circumnavigare l'Africa, ecco che il rischio di marginalizzazione dei nostri porti che si affacciano sul Mediterraneo andrebbe ad avvantaggiare i porti del Nord Europa. Segnalo come i dipendenti dell'agenzia portuale che fornisce manodopera ai *terminal* del porto di Trieste, fra i più colpiti dalla crisi, stiano lavorando in media una settimana in meno al mese. Mi chiedo cosa potrebbe accadere se questa settimana diventassero due, tre o più. Anche alcune imprese della mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia, si sono già consultate con Confindustria Alto Adriatico per una possibile apertura della cassa integrazione straordinaria a causa del rallentamento della produzione dovuta evidentemente ai ritardi nell'approvvigionamento. Ecco che la missione Aspides, che ha lo scopo di riportare la sicurezza dei traffici marittimi, è strategica per il nostro Paese. Invito chi non perde l'occasione a puntare il dito contro questo Esecutivo non a criticare, ma a ringraziare questo Governo senza il quale forse nessuno in Europa si sarebbe mosso e preso la briga di prendere l'iniziativa con una sola nave. Chi si astiene, chi non vota, chi non partecipa, chi vota contro - mi auguro davvero pochi - da che parte sta? Da quella dei porti di Gioia Tauro, di Genova e di Trieste o da quella dei porti di Rotterdam e Amburgo. Chi è contro questa missione da che parte sta? Da quella delle nostre imprese e dei nostri lavoratori oppure sta con chi rema contro un'Italia forte in Europa e nel mondo? Poi, lasciatemelo dire, penso siamo l'unico Paese dove vi sia chi inneggiando al non interventismo, magari strizza l'occhio alle milizie Houti, come se fossero i paladini della libertà. Non vi è chiaro però che se loro attaccano le nostre navi che stanno scortando navi cargo, sono loro che fanno la guerra e non noi a loro. L'abbattimento del drone lanciato dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi rappresenta, ancora una volta, la conferma della preparazione e della prontezza operativa della nostra Marina militare. *(Applausi)*. Al comandante e a tutto l'equipaggio devono andare i nostri più sentiti ringraziamenti. Sottolineo alle malelingue che il cacciatorpediniere Caio Duilio si trovava sotto attacco e - come spiegato dal suo comandante - per proteggersi poteva solo intercettare ed abbattere la minaccia, per non mettere a repentaglio l'incolumità del personale di bordo. Per cui le chiacchiere evidentemente stanno a zero. Bene ha fatto il comandante e bene farà in futuro ad agire nella stessa maniera. Ma, attenzione, minacce di questo tipo possono arrivare anche dalla dimensione subacquea; l'abbiamo già sottolineato, Ministro, in altre occasioni. Alcune società di telecomunicazioni proprio in queste ore hanno lanciato delle informazioni sui danni ai cavi sottomarini per la trasmissione di dati Internet, che portano proprio alla dorsale che va dal Golfo di Aden al Mar Rosso; un'altra minaccia da non sottovalutare. Automaticamente mi viene da pensare alle infrastrutture critiche che passano proprio per il Mediterraneo, come ad esempio i gasdotti, fondamentali per l'approvvigionamento energetico di tutta Europa, le infrastrutture elettriche e, appunto, i cavi sottomarini. L'invito al Governo, anche se sono sicuro che l'attenzione e le intenzioni sono già operative in questo senso, è a non focalizzarsi esclusivamente sul Mar Rosso, ma a cercare di usare queste informazioni con un grandangolo, proprio per rafforzare quei pattugliamenti e la protezione delle infrastrutture nel

insomma, capace di dispiegare le proprie forze a difesa dei nostri interessi nazionali, ove e quando necessario, che crea una protezione in politica estera per far accrescere anche il nostro importantissimo il peso specifico nei consessi internazionali. Per tempo avevamo pensato o forse qualcuno aveva pensato che la difesa fosse uno strumento non rilevante e di secondo piano. tanto c'era dietro l'America, che c'era qualcun altro che pensava alla nostra sicurezza; sappiamo invece che oggi, a prescindere da come andranno le elezioni americane, questo probabilmente non sarà più il caso. Ecco che, con gli equilibri mutati e con un mondo sempre più conflittuale, dove le potenze autocratiche si stanno allineando per sfidare noi e l'Occidente intero, è necessario cambiare questo paradigma. Bisogna pensare a una difesa più solida, rafforzarla nei domini tradizionali, come quello terrestre, aereo e navale, ma anche nei domini *cyber* e spaziale. Dobbiamo essere realistici, signor Ministro: minacce come quelle del mar Rosso rischiano evidentemente di ripetersi, e non solo nel mar Rosso. Investire in difesa vuol dire investire in un settore cruciale per la sicurezza e la difesa dei nostri interessi nazionali. Proprio nel programma di Governo, la difesa dei nostri interessi nazionali è e non abbiamo dubbio che le missioni Aspides e, non di meno, l'importantissima missione Levante vadano inserite in questo contesto. Come Lega-Partito Sardo d'Azione, per questo motivo, voteremo convintamente in modo favorevole alla proposta

(chiederemo di votare separatamente i punti 1.3 e 1.4). Chiederemo anche di votare per parti separate la proposta di risoluzione della maggioranza, per astenerci sulle premesse e votare invece convintamente sugli impegni. impegni. Abbiamo la consapevolezza che questo sia un passaggio non facile, che non va sottovalutato. Serve il massimo del rigore e della responsabilità quando si parla di politica estera e di missioni internazionali: per la situazione di tensione nell'area; per il rischio *escalation,* cui ha fatto riferimento anche lei, signor Ministro, nel suo intervento; per l'esigenza di tutelare i nostri legittimi interessi nazionali nell'area, sulla navigazione e la sicurezza della navigazione; per la sicurezza in cui operano gli operatori umanitari e della cooperazione e i nostri militari. Noi ci uniamo a quello che ha detto lei, al plauso per i nostri militari, le donne e gli uomini impegnati nell'area, i diplomatici e a tutti coloro che garantiscono la sicurezza e la stabilità del nostro Paese. Lo facciamo esprimendo, negli impegni, tre si convinti. Sì all'operazione Eubam, perché, quando si è trattato di sostenere l'Ucraina con tutti i mezzi, il Partito Democratico ha sempre risposto sì. Noi siamo dalla parte delle democrazie liberali, quella è la frontiera su cui si misura la capacità di difendere quei valori e quei principi. Un sì convinto all'operazione Levante, un'operazione di sostegno e aiuto rispetto alla tragedia umanitaria in corso Il Governo è intervenuto prontamente con la nave Vulcano. Noi vorremmo, oltre alla nave Vulcano, che sta lì, e oltre all'azione di coordinamento con Cipro, un *hub* che permetta

Non ci sfugge che la missione Levante dispone anche dei dispositivi di Mediterraneo sicuro, che copre non solo il Mediterraneo centrale ma anche il Mediterraneo orientale, a tutela degli interessi nazionali del nostro Paese, ma anche a supporto di chi sta operando nella zona. zona. L'idea è di lavorare sul tema dell'assistenza, dal punto di vista della sanità militare, e di aiutare chi sta soffrendo, coloro che vengono portati via da Gaza e vengono curati, negli ospedali italiani ma anche sulla nave Vulcano. Approfitto per ringraziare i tantissimi volontari che stanno collaborando, insieme ai militari, ai nostri militari, perché questo possa succedere. Ciò dimostra che l'Italia c'è, in tutte le sue componenti.

sugli aiuti umanitari e su tutto quello che possiamo fare per aiutare chi sta operando: le organizzazioni non governative e tutte le organizzazioni internazionali che in un clima complicato, difficile, in un contesto davvero da tragedia umanitaria, stanno operando a Gaza. Quindi, noi siamo vicini e ringraziamo gli operatori, le organizzazioni internazionali che stanno operando. sin dall'inizio, abbiamo dato un parere positivo nel caso si svolgesse nell'ambito di una cornice europea con un mandato di tipo difensivo. Mi sembra che si stia andando in questa direzione e, per quello, il nostro sì convinto va anche ad ad Aspides. La posta in gioco è importante, notevole. Rischiamo di mandare in fumo otto miliardi di nostro saldo commerciale:

anche qui notevole sulle economie. Per non parlare del danno, nel momento in cui aumentano i costi di trasporto per le nostre aziende, per il sistema economico produttivo italiano e dei Paesi europei; così come il danno anche per i nostri porti, perché, nel momento in cui si circumnaviga l'Africa, rischiamo un effetto di spiazzamento per i nostri porti oltre al rischio di un aumento dei tempi. E l'aumento dei tempi in economia è fondamentale per un impatto negativo sulle catene del valore. Ci sono però delle criticità, signor Ministro e, per il tramite della Presidente, le indirizzo a lei. Abbiamo delle perplessità su come si siano concentrate in un'unica scheda delle operazioni di tipo diverso: due missioni di carattere europeo, una missione con dispositivi nazionale nell'ambito di una collaborazione a livello internazionale e un dispositivo nazionale - quello di fronte alle coste del Mozambico - per la tutela dei nostri interessi nazionali, in particolare di ENI. Soprattutto abbiamo delle perplessità sui ritardi: avete deciso a fine gennaio di approvare un disegno di legge di modifica della legge n. 145 del 2016. Siamo d'accordo che si intervenga per rendere più veloce la possibilità del dispiegamento di forze di pronto intervento negli scenari dove l'*escalation* arriva in maniera fulminea e dove abbiamo bisogno di intervenire anche utilizzando assetti e dispositivi già definiti.

in procedura d'urgenza. Invece voi volevate imporci un passaggio di un giorno senza approfondire. Se vogliamo approfondire è perché vogliamo che sia garantita la sicurezza di quei militari *(Applausi)*, che abbiano l'appoggio del Parlamento, che non debbano intervenire come ha fatto il comandante di vascello (che ringraziamo per il suo lavoro, così come tutte le donne e gli uomini imbarcati a bordo), senza avere il sostegno pieno del Parlamento e la piena legittimazione giuridica.

i *leader* più populisti che sostengono questo Governo, a volte evocano uno scontro di civiltà e invitano a scendere in piazza in nome dei valori occidentali.

e Houthi; si tratta anche di quella parte di Islam politico che può contare su risorse importanti di Paesi cosiddetti moderati. Noi dobbiamo impedire la saldatura dell'asse della resistenza con l'Islam politico e anche con quelle piazze dei Paesi moderati del Golfo che spesso sono con noi alleati e che hanno costruito gli Accordi di Abramo. Tali Paesi, però, nel momento in cui vedono le immagini che arrivano dalla tragedia di Gaza, rischiano di saldarsi con l'asse della resistenza. Noi lo dobbiamo impedire per questo serve un'iniziativa forte anche dell'Italia. Ricordiamoci la nostra storia, la storia di chi viene anche dall'esperienza della Prima Repubblica e sa quanto sia stato fondamentale che si sia tenuta la barra dritta in una postura - così si direbbe oggi - positiva, di dialogo con il mondo arabo moderato, che ha permesso anche la sicurezza del nostro Paese. Non dimentichiamolo. Termino con un'altra considerazione. Signor

Ebbene, lei la pensa in maniera diversa da alcuni suoi compagni di viaggio a cui bisognerebbe spiegare che, se vogliamo impedire l'*escalation* e contare di più nello scenario internazionale, non possiamo che spingere sul rafforzamento dell'Europa, della politica estera, della difesa europea. *(Applausi)*. I suoi colleghi, che siedono con lei, hanno invece dato mandato in Parlamento europeo di votare contro la riforma dei Trattati, unica possibilità per rafforzare la politica estera e di difesa comune. Cercate di ritrovare un po' di coerenza, perché la politica estera del nostro Paese e la nostra credibilità si potranno misurare e saranno più forti nel momento in cui l'Europa sarà più forte e noi saremo protagonisti dentro quelle dinamiche.

cercare di rafforzare anche alcune delle cose che lei ha detto per sostenere l'impegno del Governo e motivare la nostra posizione. Ricordo, signor Ministro, che qualche mese fa eravamo all'indomani dell'aggressione terroristica di Hamas in quest'Aula ebbi modo di ricordare un libro, quello di Francis Fukuyama, che profetizzava la fine della storia immaginando che la storia si fosse fermata e finita, all'indomani della caduta del muro di Berlino. In quell'occasione

datata due anni e aveva dato la stura a tanti conflitti: molti conflitti regionali stavano diventando globali, dissi che dovevamo prepararci a qualcos'altro e intravedevo quel che accadeva nel mar Rosso. Non è che io sia stato un profeta, bastava leggere quello che accadeva.

impegno a far partecipare personale della magistratura italiana alla missione civile dell'Unione europea in Ucraina, questo con lo scopo di sostenere l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza.

È l'operazione che noi andiamo ora a sostenere, cioè quella che vuole creare una *de-escalation* rispetto alla situazione di Gaza. È quindi una missione che impone un approccio integrato per evitare l'estensione del conflitto su scala regionale ed impone anche e soprattutto la protezione delle popolazioni civili, l'erogazione di aiuti umanitari, l'aviolancio di beni, tutte cose che sappiamo nobilmente fare. La terza, quella che politicamente è non la più importante, ma sicuramente la più controversa in questo momento e anche quella più impegnativa e pericolosa, perché le cose vanno dette,

a quattro anni prima della scoperta dell'America. Oggi, leggendo certe cronache che arrivano dagli Stati Uniti, secondo la cultura *woke* noi dovremmo chiedere scusa e abbattere le statue di Cristoforo Colombo. della scoperta dell'America, nel 1488, un esploratore portoghese, che si chiamava Bartolomeu Dias, andò a girare intorno al Capo di Buona Speranza e scoprì che si potevano così connettere via mare due Continenti che si pensava potessero connettersi invece solo via terra. Cioè navigò attorno al Capo di Buona Speranza la sua scoperta, di fatto, aprì la strada al trasporto marittimo globale, cioè permise alle navi di viaggiare tra l'Asia e l'Europa. Certo, il viaggio era lungo, ma aggirare il Capo di Buona Speranza consentiva di spostarsi via mare in due Continenti. Passarono poi quasi quattro secoli e la realizzazione del Canale di Suez, nel 1869, svuotò d'improvviso l'importanza capitale del Capo di Buona Speranza; quel canale, infatti, collegando direttamente il Mar Rosso al Mediterraneo, ha ridotto drasticamente i tempi di viaggio delle navi. Lasciatemi ora parlare da senatore di Trieste. Ricordo che il barone Revoltella, che ha lasciato una magnifica collezione d'arte, tra l'altro, vice presidente del Canale di Suez, diceva ai triestini di allora, con fascino

l'Oceano Indiano al Mediterraneo. Noi, che siamo la piattaforma avanzata sul Mediterraneo, non possiamo che temere drammaticamente quello che accade da quando gli Houthi hanno scoperto

influenza globale, attaccando le navi sul mar Rosso. Ci riguarda evidentemente in modo drammatico. Pensate che lo stretto tra Gibuti e lo Yemen si chiama Bab el-Mandeb, che vuol dire «porta del pianto funebre», quindi non potrebbe avere un nome più indicativo. Chiudendo quella porta, infatti, si interrompe una rotta critica e fondamentale per il trasporto del petrolio, delle materie prime, dei semilavorati, delle merci. L'Italia dipende dal Canale di Suez per il 40 per cento del suo *import-export;* il nostro *import-export* vale circa 150 miliardi di euro e si prospettano conseguenze disastrose sul *made in Italy*. Coldiretti, per esempio, ha calcolato che siano a rischio 6 miliardi di euro delle nostre esportazioni solo sulla filiera agroalimentare.

si sono create nuove compagnie di navigazione (non lo sa quasi nessuno): sono tutte di origine cinese e servono a passare il Canale di Suez con operazioni di trasbordo, perché, come sapete, gli Houthi fanno una pirateria selettiva,

sono un'organizzazione armata, non dei simpatici piratini come quelli che si disegnano nei cartoni animati, ma molto più pericolosi, per esempio, di Hamas. Pochi sanno quale sia la loro capacità bellica: sono muniti di missili, di razzi e missili antinave, mezzi robotizzati *underwater* (guardate la questione dei collegamenti sottomarini per la trasmissione dei dati); hanno i barchini minati l'episodio della nave Caio Duilio di qualche giorno fa lo sta a dimostrare. Di fronte a tutto ciò, è del tutto evidente che l'interesse nazionale italiano si misura e si tutela con un intervento diretto italiano ed europeo.

perché l'Italia guiderà questa missione con il ruolo di *force commander*. È un passo significativo per noi, per il ruolo dell'Italia, per la sicurezza delle rotte marittime globali e dunque per la sicurezza collettiva. Va sottolineato - lo ripeto ancora una volta - come Aspides veda l'Europa dare per la prima volta una risposta comune. Aspides sarà anche un banco di prova per il G7 a guida italiana, che già se ne è occupato nelle scorse riunioni e per il futuro certamente i *meeting* del G7 mireranno a consolidare sempre di più la sorveglianza navale per il benessere di tutti. In conclusione, quando la storia corre, gli equilibri si ridisegnano, i popoli e gli Stati possono decidere di stare in seconda fila e seguire le partite scritte da altri, oppure si assumono le responsabilità anche accettando, come è ovvio, i rischi del caso. Questo è quello che noi facciamo, con coscienza e con consapevolezza, con il voto favorevole alla risoluzione che impegna l'Italia in questa missione. nave Caio Duilio ha abbattuto un drone armato degli Houthi in rapido avvicinamento: è il primo abbattimento di una minaccia aerea su una nave della Marina militare dalla Seconda guerra mondiale. Il teatro, in tutta evidenza, è un teatro difficile. prima di tutto, agli uomini e alle donne d'Italia che oggi incrociano in quelle acque, in una missione che è difficile e pericolosa, ma vuole segnare il ruolo dell'Italia nel mondo, non in coda agli altri, ma davanti agli altri, per ristabilire le regole del diritto, della libertà, della civiltà, delle relazioni internazionali.

le care genti e quelli che per tutti noi nella cadente notte vegliano in armi sul mare.

preclusa la proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori. Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024. Per consentire i lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 15. *(La seduta, sospesa

che ha coinvolto centinaia e centinaia di esponenti, prevalentemente politici, ma anche del mondo dello sport, della musica e della cultura. Non sono ancora chiara la la motivazione di questa vicenda, che, per il luogo di provenienza assume - a mio avviso - una gravità superiore a quella di scandali che pure hanno segnato la vita ahimè - triste della Repubblica da questo punto di vista. Penso alla P2, penso alle varie P, inventate o numerate: tre o quattro. Penso alla cosiddetta loggia di piazza Ungheria: non so come l'abbiano definita.

È un'istituzione importante, per le funzioni che svolge e per come è nata, in anni drammatici della vita italiana. Fu ideata da Giovanni Falcone, che tutti spesso citiamo come atto di omaggio ad una delle icone della storia della Repubblica.

procura antimafia arriva di tutto, per accordi intervenuti negli anni - ma anche persone che non sono neanche indagate. Se si chiama procura antimafia e antiterrorismo, ci si aspetta - come avvenuto in tante occasioni, rispetto alle quali rendiamo omaggio a quella procura per le cose virtuose che ha fatto nel corso dei decenni - che si occupi di

comunque un problema che non può essere coperto dal segreto professionale. Poi ho letto il nome di tre giornalisti e non so se ce ne sono altri cinque e chi siano. La Commissione antimafia lodevolmente se ne occuperà nelle prossime ore e anche il Copasir. Credo che anche il Governo - questo è il senso del mio intervento - debba venire qui in Aula. Leggendo i giornali mi è venuto da pensare a un articolo del «Corriere della sera» che connette i nomi e le date alla cronaca politica. Se Mario Rossi - cito un nome di fantasia - veniva evocato come candidato sindaco ad esempio di Forlimpopoli, quel giorno si fa l'accesso. Potrei citare persone che sono presenti in quest'Aula e che erano alle massime cariche delle istituzioni; si parlava di elezioni alle supreme cariche e si fa l'accesso a quel nome. Ma per scoprire che cosa?

mafia e con il terrorismo, con nessuna indagine di nessun tipo, eppure vengono "visitate". Il maresciallo, poi diventato forse tenente, ha fatto tutto da solo? Che cosa hanno rilevato i magistrati preposti alla guida di quella procura? Io l'ho detto più volte e lo ribadisco anche in c'è una strana coincidenza, poiché tutti i procuratori nazionali antimafia diventano parlamentari nazionali ed europei della sinistra italiana. È un loro diritto, è una loro facoltà, ma è una strana coincidenza: tre su tre. Spero che quello attuale ci sorprenderà evitando di candidarsi in Parlamento. Questo ci fa guardare a quella istituzione con qualche dubbio, rendendo omaggio alle pagine eroiche che ha scritto, ma vedendo con più scetticismo altre pagine. Non voglio alzare i toni, anche se sarebbe facile. La mia parte politica è la più come dire - visitata nelle SOS: parlo del centrodestra e anche il mio partito è stato super visitato. È una vicenda inquietante. Credo che si dovrebbe disporre un'ispezione immediata alla procura. Non so se esista una norma per un commissariamento della procura, ma forse servirebbero misure straordinarie, perché in altri casi ci sarebbero già gli scioperi. Mi auguro che anche il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che ha giustamente vigilato sulla tranquillità del Paese in occasioni recenti, faccia sentire la sua voce su questo scandalo enorme, anche in quella sua qualità questo scandalo enorme, anche in quella sua qualità che deve dare delle garanzie, come ha fatto nei giorni scorsi, su temi dell'ordine pubblico o della legalità. Bisogna stare attenti a tutta la vita del Paese. Quindi, mi auguro che già le audizioni dei prossimi giorni ci diano degli elementi, che il Governo venga in quest'Aula e ci sia anche il rispetto di alcune incompatibilità. Nelle prossime ore solleveremo - l'abbiamo già sollevato - un problema: non è che chi ha diretto la procura antimafia, stando in Commissione antimafia, si fa le domande e si dà le risposte. È un conflitto di interesse grandioso *(Applausi)* che noi solleviamo avanti al Paese e non consentiremo la presa in giro delle istituzioni. Vorrei vedere il parlamentare che fa le domande sulla gestione che lui ha avuto, perché ci sono parlamentari in carica che hanno diretto la procura antimafia e durante la loro presidenza si sono verificati questi episodi. A loro insaputa? Certamente, è probabile, però con una loro responsabilità. Oggi, a ruoli invertiti, saremmo di fronte allo sciopero generale. Non facciamo lo sciopero generale, ma esprimiamo indignazione. Vogliamo verità e e giustizia su questo che è il più grave scandalo del tempo recente.

di ragionamento su quello che sta emergendo negli ultimi giorni. Io reputo questo sistema di spionaggio qualcosa di antitetico rispetto alla nostra democrazia ed è assolutamente evidente che dietro a questa vicenda potrebbe esserci un sistema o un disegno. Lo dico da rappresentante di una forza politica, Italia Viva, il cui *leader* è stato il primo ad essere vittima di tale sistema e anche il primo a denunciarlo. Allora, noi abbiamo il dovere di andare fino in fondo, in tutte le sedi competenti, per cercare di capire davvero che cosa c'è dietro questa incredibile vicenda e lo dobbiamo fare anche e soprattutto ascoltando delle parole I procuratori hanno già chiesto di essere auditi, per esempio dalla Commissione antimafia di cui faccio parte, e in quella Commissione è evidente che siedono

loro compatibilità rispetto a vicende che riguardano anche l'esercizio del loro mandato è serissimo. Per esempio, ieri abbiamo assistito ad un'arringa da parte dell'onorevole De Raho, che ha spiegato dal suo punto di vista che cosa è accaduto e quali sono le regole che governavano l'antimafia: perfetto. Il punto, però, siccome stiamo parlando di vicende per le quali - io credo - la Commissione antimafia ha il diritto di farsi un'opinione autonoma, bisogna capire se figure che stanno raccontando vicende delle quali sono state in qualche modo protagoniste possano essere audite all'interno di quella Commissione, in qualità di commissari commissari o di persone che hanno ricoperto delle funzioni precedentemente. Io non faccio il processo a nessuno, ma dico solo che voglio trovarmi nella condizione di autonomia nel poter esprimere il mio giudizio dentro quella Commissione antimafia e non posso assistere a veri e veri e propri comizi senza poter fare una domanda circa i fatti che si raccontano. Allora, Presidente, glielo dico qua: la richiesta arriverà anche a lei perché, se l'onorevole De Raho ha da dirci delle cose, lei è titolato a decidere se è possibile fare un'audizione dell'onorevole De Raho in quella Commissione. È lei ad avere incaricato ognuno di noi a stare dentro specifiche Commissioni, e anche in quella delicatissima dell'antimafia. Ripeto: non ho aperto io questa discussione, ma, dal momento in cui ci sono state esternazioni, a quelle esternazioni voglio porre delle domande; voglio capire qual è la verità e voglio essere nella condizione di potermi fare una specifica valutazione rispetto a fatti gravissimi che - ripeto - nulla hanno a che vedere con una realtà democratica, che aprono dei fari e degli interrogativi di una certa delicatezza e sui quali penso, in tutte le Commissioni di cui facciamo parte, dobbiamo andare fino in fondo. Nessun processo, però la ricerca della verità sì: questo è il nostro stile e su questa vicenda dello spionaggio, anche per l'entità e il numero delle persone coinvolte, per l'entità e la qualità delle persone coinvolte - imprenditori, politici e privati cittadini vogliamo vedere fino in fondo che cosa c'è dietro e capire quale possa essere il nostro ruolo a tutela della democrazia in questo Paese.

investigati, analizzati, chiariti; vanno inoltre capite e attribuite le responsabilità e capire chi eventualmente ne ha. Da questo punto di vista credo ci debba essere la massima collaborazione in Parlamento e nelle Commissioni a ciò

È del tutto evidente che anche la mia forza politica, al suo massimo livello, è stata colpita da quest'attività piuttosto irrituale, del Consiglio Conte e anche la sua compagna, che sono stati oggetto d'indagine. È pertanto evidente che anche da parte nostra ci debba essere la richiesta di chiarire i contorni di quella vicenda. Attenzione però - e lo dico con i toni più bassi possibili - a non trasformare una richiesta legittima di chiarezza del Parlamento in un chiacchiericcio politico e in un dibattito meramente politico strumentale perché su questo non siamo d'accordo. Pensare a incompatibilità di autorevoli colleghi, che a mio avviso invece si connotano per la grande esperienza che hanno nel campo della lotta alla criminalità organizzata e che possono contribuire all'interno di quella Commissione ad innalzarne il livello di capacità investigativa, credo sia un valore che questo Parlamento deve proteggere, a prescindere dal colore politico e di appartenenza politica dei parlamentari

per la giacchetta il Presidente del CSM, che - guarda caso - è anche Presidente della Repubblica e non ha certamente bisogno delle nostre sollecitazioni per decidere quando e come intervenire. *(Applausi)*.

dovrebbe interrogare tutti quanti in quest'Aula sul grado di libertà che vige nel nostro Paese da un po' di tempo a questa parte. Leggere un titolo di giornale che parla di politici, imprenditori, sportivi, VIP, uomini dello spettacolo, privati cittadini spiati o sorvegliati, con *dossier* dai quali partono delle indagini pilotate - questo è ciò che hanno titolato i giornali in questi giorni indubbiamente non può essere che giudicato - poi tutto è da verificare e chiarire - come un fatto gravissimo. Ha fatto molto bene Matteo Salvini a parlare di vergogna di stampo sovietico.

si potrebbero spiegare anche alcune inchieste che parlavano di rubli e che poi sono finite in bolle di sapone, ma che sono servite per infangare il nostro partito per anni e anni *(Applausi)*, attribuendogli responsabilità che non erano mai state messe in evidenza. Potremmo anche accennare a tante altre situazioni - adesso il tempo non c'è, perché il Presidente ha dato cinque minuti per Gruppo - però forse questi episodi e quello che sta succedendo oggi testimoniano il fatto che la libertà e la democrazia - ha ragione la senatrice Paita quando parla di tutela della democrazia - sono in pericolo, e

al quale bisogna prestare molta attenzione. I segnali sono tanti, perché li abbiamo visti negli ultimi tempi: il dossieraggio degli ultimi giorni è forse una conferma di come abbiamo già visto limitare la nostra libertà di espressione e di parola. Posso fare degli esempi vissuti in prima persona. È stato sufficiente, durante la pandemia, avanzare un dubbio sulla gestione dell'emergenza per essere subito tacciati di essere nemici della scienza. È bastato invocare una una soluzione diplomatica del conflitto per essere bollati di complicità con il nemico. È sufficiente scrivere un libro esprimendo le proprie idee, di cui magari anch'io personalmente non condivido tutto - mi riferisco al generale Vannacci - per essere indagati per reato di opinione in questo Paese.

delegittimare, discriminare e criminalizzare chi esce dal pensiero dominante, dichiarando fuorilegge tutti coloro che non si adeguano a quel pensiero. Forse di fronte a tutto questo, perché abbiamo capito che le opinioni nel nostro Paese sono libere solo se vanno in una direzione,

del fatto che esponenti delle istituzioni siano stati spiati e che tutto questo sia finito sui giornali, in quanto ciò rappresenta sicuramente un *vulnus* alle istituzioni alla democrazia. È qualcosa che non appartiene allo Stato di diritto e quindi mi auguro che si faccia piena luce su quanto è avvenuto. Al tempo stesso, riprendo una proposta del collega Costa che mi sembra molto ragionevole. Solo nel 2023 ci sono state 150.000 segnalazioni di operazioni sospette,

violare la segretezza di alcune informazioni e soprattutto svilire la dignità e la credibilità di una persona e che tutto questo avvenga in maniera ordinaria è un fatto estremamente grave, non degno di uno Stato di diritto. Quindi, penso che laddove queste operazioni vengano fatte bisogna comunque

Signor Presidente, noi siamo stati i primi a intervenire quando l'altro ieri due servitori dello Stato come il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo hanno chiesto a Copasir, Commissione antimafia e di essere auditi per le notizie che erano uscite sui giornali. Siamo stati i primi, accompagnati poi naturalmente dalla Presidente della Commissione antimafia e da tanti altri esponenti, perché siamo i primi a volere chiarezza e verità su quanto è successo.

un ufficiale della Guardia di finanza e un magistrato, temporaneamente distaccati a quell'organismo di contrasto alla criminalità organizzata - hanno tenuto e per i quali la procura di Perugia ha aperto un'indagine.

possono avere incrociato reati associativi di competenza della procura antimafia, questa allora interviene. Per la stragrande maggioranza degli accessi, però, i vertici della procura non intervengono perché non è loro competenza. Se due due persone, allocate temporaneamente, hanno fatto questi accessi abusivi all'insaputa dei vertici delle procure che si sono succedute, noi ci vogliamo chiedere perché lo hanno fatto, cosa c'è dietro, quali affari ci possono essere, leciti o illeciti; certamente non leciti perché erano accessi Ci chiediamo anche chi è questo magistrato, qual è la sua storia associativa dentro la magistratura, a quale corrente appartiene perché certamente - per usare un luogo comune che è nel dibattito politico - tutto è il dottor Laudati meno che una famigerata toga rossa,

Noi siamo orgogliosi di aver contribuito negli anni all'elezione in Parlamento di personalità come Pietro Grasso

da certe forze - nel nostro caso dal PD - perché noi volevamo e vogliamo portare la loro esperienza di lotta alla mafia in queste Aule. Noi vogliamo portare la lotta contro le mafie e la criminalità organizzata in Parlamento. Se tutti, tutte le forze politiche avessero candidato ex procuratori antimafia che hanno speso la vita contro le mafie, che vivono sotto scorta, invece di candidare condannati per associazione mafiosa, forse sarebbe stato molto meglio. *(Applausi)*. Infine, Presidente, nel chiedere davvero chiarezza,

Attenzione, però: c'è un'altra cosa che ci preoccupa. Non si può prendere il comportamento di qualche magistrato per attaccare la magistratura, così come non si può prendere il comportamento di un magistrato della procura nazionale procura nazionale antimafia. dovere e, se pubblica dei fatti, non va attaccato perché, come la magistratura, è un presidio della democrazia.

Signor Presidente, credo che siamo di fronte a un fatto molto grave e il fatto stesso che ci sia un tentativo di minimizzare o di dare la colpa a chi questo fatto denuncia, lo rende ancora più grave. Fratelli d'Italia ha chiesto subito di poter avere in Commissione antimafia questi documenti, visto che le notizie continuiamo ad averle solo dai giornali. Peraltro, non mi è chiaro come i giornali abbiano queste notizie, con tutti gli elenchi e i dati. Sta di fatto che le hanno e, a quanto pare, sono notizie reali e preoccupanti. preoccupanti. Spero che ben presto avremo, nelle apposite sedi, maggiore chiarezza e maggiori dettagli; però abbiamo appreso che queste interrogazioni, cioè gli accessi abusivi a dei dati riservati,

Abbiamo avuto un aumento straordinario di queste interrogazioni, con il picco proprio intorno alle scadenze elettorali. Ora, se questo fosse avvenuto a livello internazionale, parleremmo di tentativi di influenzare l'andamento delle elezioni. È avvenuto invece a livello nazionale e c'è sempre quantomeno il sospetto di un tentativo di influenzare l'andamento delle elezioni, andando a trovare qualche cosa di

far diventare imbarazzante per gli avversari politici. È vero che non tutti gli esponenti - a quanto se ne sa oggi, ma forse l'elenco non è completo - oggetto di questa attività di assunzione di informazioni illecite sono di centrodestra. Vero. Ce n'è solo una grandissima prevalenza e già questo dovrebbe inquietare. Aggiungiamo una cosa: abbiamo appreso che l'ex presidente del Consiglio Conte, ora *leader* di un'importante partito, il MoVimento 5 Stelle, è stato anche lui oggetto di queste cose, ma parrebbe che ciò sia avvenuto solo durante l'esperienza del Governo Conte I, mentre durante l'esperienza del Governo Conte

Credo che, se la situazione fosse opposta e se ci fossero il centrosinistra al Governo e il centrodestra all'opposizione, forse cambierebbero i criteri. Comunque ci sono dei giornalisti che dicono che va bene fare dossieraggio

un parlamentare, un esponente politico o anche non politico (ci sono diversi non politici in questi elenchi), tutto ciò dovrebbe andare bene. Allora le garanzie della riservatezza dei dati personali riguardano sempre e solo gli altri; sono gli altri che devono rispettare tali garanzie. *(Applausi)*. Quando invece fa nel nome della deontologia giornalistica. Non c'è poi solo la deontologia giornalistica. C'è anche la deontologia dei magistrati, che svolgono un ruolo fondamentale, hanno giustamente degli ampi poteri, proteggono la sicurezza di tutti; ma questo impone anche a loro una determinata accuratezza e una determinata diligenza nel condurre il loro operato. Se un magistrato, a capo di una procura, non si accorge

incompatibile con il partecipare ai lavori di una Commissione che dovrebbe fare proprio quello, e cioè andare a trovare quelli che c'erano e non dormivano. Detto questo, non entro nell'aspetto dell'incompatibilità formale, perché non è di competenza nostra. Ma ritengo quantomeno imbarazzante che una Commissione che deve svolgere delle audizioni su tale abbia, tra i suoi membri, qualcuno che era lì e che, di conseguenza, probabilmente si difenderà rispetto alle eventuali responsabilità che dovessero emergere sul suo conto. Concludo, signor Presidente, ribadendo che è necessario fare piena chiarezza e che è opportuna la collaborazione di tutti. Forse qualcuno pensa che toccherà sempre e solo agli altri, ma non si sa mai, perché le cose perché le cose potrebbero andare a danno di chiunque. Io spero di no, perché spero che queste azioni illegali non vengano fatte a danno di nessuno, tantomeno dei nostri avversari politici. Però, queste cose non vanno fatte, non vanno difese e non vanno mascherate col nobile, nobilissimo principio della libertà di stampa.

dare rilievo a un argomento che sta riempiendo le pagine dei giornali e che tocca una questione sicuramente sensibile per la democrazia e il Parlamento. **Discussione del di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico"

di essere relatore sul decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024; un decreto-legge di fondamentale importanza per la nostra nazione, che il *premier* Giorgia Meloni e il ministro Adolfo Urso hanno inteso predisporre e successivamente fare approvare con un assoluto tempismo, con l'obiettivo di determinare la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, tutelando, quindi, non soltanto la produzione, ma anche i lavoratori, l'indotto, l'ambiente e la salute dei cittadini. É un provvedimento fondamentale non soltanto per lo stabilimento pugliese, la produzione di acciaio italiana e per il sistema manifatturiero italiano, che è il secondo in Europa e si basa sulla produzione di acciaio; un provvedimento, quindi, che ha refluenze

approvare questo decreto-legge, che è stato accolto, in maniera trasversale, con grande soddisfazione dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali, dagli enti territoriali,

da undici anni a questa parte, a testimonianza dell'importanza strategica dello stabilimento di Taranto, ma a testimonianza, altresì, di alcuni gravi errori che sono stati commessi dai Governi che si sono alternati ed altresì

scese a 3 milioni nel 2023. Non sono stati mantenuti neppure gli impegni in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale. rilancio industriale. Caro presidente De Carlo, non dobbiamo dimenticare che i patti parasociali firmati con ArcelorMittal furono fortemente sbilanciati a favore del socio privato, togliendo allo Stato margine di azione e ponendolo in una condizione di subalternità rispetto al socio privato. L'anno scorso il Governo Meloni era già intervenuto con un decreto-legge, per il quale anche in quel caso ho avuto l'onore e l'onere di essere relatore, che sanciva un finanziamento di 680 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia, per garantire anche in quel caso la continuità aziendale, e stanziando altresì 1 miliardo di euro, che in realtà era stato stanziato in un precedente decreto, ma che poteva essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Grazie a quel decreto-legge è stato esteso l'orizzonte temporale per utilizzare quel miliardo di euro fino al 31 dicembre 2023 per sostenere eventuali esigenze finanziarie aggiuntive della società. il gruppo indiano ArcelorMittal si è rifiutato di ricapitalizzare la società, i cui debiti nei confronti dei fornitori sono superiori al miliardo di euro. Ecco perché, colleghi, non vi era alcuna strada alternativa al decreto-legge in discussione e non vi era alcuna strada alternativa alla nomina di un commissario straordinario che, fra le altre cose, è stato individuato nell'ingegner Giancarlo Quaranta, persona di altissimo livello qualitativo, profondo conoscitore del sistema siderurgico italiano, profondo conoscitore altresì di quell'impianto strategico tarantino. È una nomina - lo voglio sottolineare, perché credo non debba essere dimenticato - questa che è stata accolta con grande soddisfazione, in maniera assolutamente trasversale, *in primis* dalle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL, cosa che non accade con grande frequenza in situazioni similari a quella che stiamo affrontando. Prima di entrare nel merito del contenuto del decreto-legge, mi sembra doveroso evidenziare l'eccezionale lavoro sinergico che si è svolto all'interno della 9a Commissione, retta come sempre con grande competenza ed equilibrio dal presidente De Carlo, grazie al contributo importante e qualificante che tutti i Gruppi parlamentari hanno dato alla stesura degli emendamenti e al dibattito. I Gruppi d'opposizione - lo voglio dire pubblicamente - si sono caratterizzati per l'attività emendativa qualificata e qualificante che ha trovato ospitalità all'interno del testo approvato dalla Commissione. Un ringraziamento particolare voglio esternare al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto per il ruolo che ha svolto con grande costanza, con grande equilibrio, con grande competenza. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Di Cesare, al dottor Veltri, a Laura Tempestini, per il lavoro di supporto che hanno svolto a tutela del lavoro qualificante della 9a Commissione. Veniamo alla relazione. Il disegno di legge in esame interviene sulle vicende che hanno interessato gli stabilimenti dell'ex Ilva, per i quali è intervenuto dapprima il decreto-legge n. 4 del 2024, cui è seguito il decreto-legge n. 9 del 2024. Si segnala che il secondo decreto-legge in materia di tutela delle imprese e dell'indotto ha raccolto le esigenze emerse durante le oltre trenta audizioni svolte in Commissione proprio sul decreto-legge n. 4. Per dare continuità a due provvedimenti di urgenza, il Governo, con l'emendamento 2.0.1000, presentato in Commissione, ha trasfuso i contenuti del decreto-legge n. 9 nel provvedimento in esame. Durante l'*iter* in Commissione sono stati approvati emendamenti, che hanno visto - come ho detto prima - la convergenza fra le forze politiche su alcuni temi centrali riguardanti in particolare le garanzie per le imprese creditrici di Acciaierie d'Italia e per i lavoratori, un'esigenza trasversale che era stata evidenziata durante le trenta audizioni. Nel dettaglio, l'articolo 1, modificato dalla Commissione, consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. È esattamente quello che poi si è puntualmente verificato all'interno del caso dell'ex Ilva. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Proprio questa disposizione ha consentito al socio pubblico, Invitalia, di avanzare richiesta di amministrazione straordinaria dopo il fallimento delle ulteriori trattative con il socio privato, nell'ambito della quale è stato nominato il nuovo commissario straordinario. Durante l'esame in Commissione sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 1-*ter*, secondo i quali, per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, si ritiene che le prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali si verifichino non solo tramite la cessione dei complessi aziendali, come previsto a legislazione vigente, ma anche tramite la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi oggetto gli stessi complessi aziendali. Ciò consentirà maggiori prospettive di rilancio per i soci privati che subentreranno in Ilva. Entro sei mesi dal provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario deve comunicare il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 2, modificato in Commissione, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso, della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva SpA, qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Detto finanziamento è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario. Si segnala che, nelle more dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto di concessione del finanziamento, introdotto tramite un emendamento in Commissione, l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto un trasferimento di risorse, pari a 150 milioni di euro, dall'amministrazione straordinaria di Ilva SpA all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia SpA, nel frattempo disposta in virtù dell'articolo 1. L'articolo 2-*bis*, che recepisce, con modifiche, i contenuti del decreto-legge n. 9, riconosce condizioni agevolate di accesso al fondo di garanzia PMI, a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. È ammessa la procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge stesso. L'articolo 2-*quater*, modificato in Commissione, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari dei garanti tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. la non revocabilità dei pagamenti e delle cessioni dei suddetti crediti effettuati fra l'entrata in vigore del decreto-legge in conversione e l'apertura della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Durante l'esame in Commissione sono stati introdotti i commi 3 e 4, che prevedono alcuni aspetti certamente importanti. Voglio soltanto sottolineare la possibilità per le Regioni, preannunciata durante l'audizione del presidente della Regione Puglia Emiliano e confermata dal ministro Urso, di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione derivante da trasferimenti statali per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese dell'indotto, nel rispetto della normativa europea di aiuti di Stato. Poi vi sono altri articoli e altri emendamenti che ho inserito nella relazione che lascio ovviamente agli atti. L'articolo 4-*bis,* introdotto in Commissione, interviene in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, con due obiettivi principali: allargare il perimetro delle imprese che possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e anticipare la chiusura della fase concorsuale liquidatoria con la conversione in liquidazione giudiziaria quando, in sostanza, non ci sono più speranze di ripresa dell'attività produttiva, considerato che la finalità dell'amministrazione straordinaria è proprio quella di assicurare prosecuzione, riattivazione e riconversione industriale. ritengo sia stato fatto un ottimo lavoro all'interno della Commissione. Ovviamente la discussione evidenzierà eventualmente altri aspetti innovativi, con alcuni emendamenti che sono stati presentati e che mi auguro possano essere accolti anche dall'Assemblea. *(Applausi)*.

Signora Presidente, oggi parliamo dell'Ilva, una delle più importanti aziende che hanno caratterizzato la storia industriale del nostro Paese. Mi sono dedicata molte volte alle sue varie crisi che si sono susseguite in questi anni; l'unica cosa andata bene è stata l'accordo di programma di Genova, che ho firmato un po' più di vent'anni fa. In quell'accordo eravamo riusciti

non sono stati caratterizzati allo stesso modo da tutela ambientale, tutela occupazionale e produttiva. Abbiamo vissuto a più riprese quella che mi permetto di definire, signora Presidente, come una storia infinita, in cui molto spesso la politica non ha dato il meglio di sé.

a salvaguardare l'ambiente - Taranto ne è la dimostrazione davanti a tutti - ma nemmeno la qualità del lavoro, se penso, ad esempio, ai dati di infortuni e anche di morti sul lavoro che in questi anni si sono susseguiti. Tornando indietro nella mia memoria, per le cose che ho fatto per quarant'anni con tanta passione, direi che l'Ilva potrebbe diventare un caso di scuola per insegnare ai nostri giovani e alle nostre giovani cosa non si deve fare quando si ha, invece, l'opportunità di di essere tra i primi produttori, anche per qualità, dell'acciaio che abbiamo sempre prodotto come un'azienda a livello europeo.

cosa non si deve fare quando si affidano a speculatori le sorti di una grande impresa e come la politica e le istituzioni non devono diventare strumento di divisione e di conflittualità, tanto da creare danno alle

di volontà del Governo di aprire subito un confronto importante con le organizzazioni sindacali e con le con le forze di maggioranza e di opposizione in quest'Aula, hanno creato, purtroppo, un'altra condizione che ci ha portati davvero molto vicini al tracollo. Con questo decreto-legge, signora Presidente, cerchiamo di mettere un'altra pezza alla vicissitudine L'amministrazione straordinaria, uno dei punti chiave del decreto, ovviamente a questo punto non era più evitabile, e di questo siamo tutti molto consapevoli.

quelli che potremmo chiamare, stendendo un velo pietoso, i conflitti di competenza tra il ministro Fitto e il ministro Urso, probabilmente qualcosa di meglio avremmo assolutamente

che cosa ci sarà mai stato in quel rapporto che nessuno è stato in grado di discutere e approfondire? Un segreto tra un imprenditore che si è dimostrato assolutamente inefficace e inefficiente e che non ha mai rispettato i patti

signor Presidente, la produzione dell'acciaio è un *asset* strategico per questo Paese; non è qualcosa di secondario,

come il nostro (nonostante tanti nostri errori, continuiamo a essere, per adesso, la seconda potenza industriale nella nostra Europa) ha bisogno di acciaio. Ne hanno bisogno le nostre industrie manifatturiere, ne hanno bisogno, ovviamente, i nostri interventi infrastrutturali: perché si è dovuti arrivare al punto

atti di chiarezza anche sulla *governance*, altra lacuna davvero importante in questo decreto? Subentra lo Stato, finalmente. Noi tutti ci auguriamo che i commissari facciano un gran buon lavoro e abbiano finalmente competenza industriale, perché nel passato questo non sempre è avvenuto. Ma non capiamo

i gravi problemi delle tante aziende dell'indotto che in questi mesi non sono state pagate *(Applausi)* e, quando non si sono pagate le imprese, non si sono pagati gli stipendi ai lavoratori e alle lavoratrici. È da dicembre che non ricevono un euro. Ecco, forse, quei 300 milioni possono servire a questo, ma non c'è una parola, Presidente, che dia respiro

Voglio ringraziare il grande lavoro dei colleghi del Partito Democratico in 9a Commissione. A loro dobbiamo emendamenti che hanno aggiustato un po'...

È una proprietà pubblica che vuole costruire il più grande polo industriale del Sud Italia. Nel 1965 viene inaugurato lo stabilimento nella splendida Taranto e, in breve tempo, la fabbrica pugliese diventa il più grande e importante stabilimento di ferro e di acciaio d'Europa; il serbatoio che fornisce non solo il dinamico Nord Italia, ma anche mezza Europa. Tale stabilimento dà lavoro, crea ricchezza ed è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia del *boom* economico. Dagli anni Ottanta in avanti, con la grande crisi del settore, inizia il primo e significativo corto circuito. Nonostante la spinta iniziale data dal buon esito del piano Nippon Steel, il ciclo espansivo dell'Ilva si arresta in maniera irreversibile ed è in quel periodo che inizia il secondo significativo corto circuito. Lo Stato decide di privatizzare questo *asset* e lo fa svendendo - sottolineo svendendo - l'attività al gruppo Riva. A fronte di una perizia di valutazione di 4.000 miliardi, il prezzo della vendita è stabilito in 2.500 miliardi. Ve lo ricordate Dini? La storia infinita dell'Ilva potrebbe continuare ed impegnare per settimane il dibattito di quest'Assemblea. Nulla è stato risparmiato; sequestri, procedimenti penali e condanne, ma è proprio così che si divaga, perdendo di vista il punto di svolta e, ancora e, ancora una volta, di assunzione di responsabilità che fa oggi il Governo Meloni. Per quanto sarebbe comodo gettare il passato nell'oblio, rivolgere il pensiero esclusivamente al futuro, non possiamo e non dobbiamo tuttavia dimenticare gli sfregi avvenuti a partire dall'accordo con la cordata ArcelorMittal, che si aggiudicò la gara indetta dall'allora MISE. La società aveva condizionato la sottoscrizione dell'accordo al cosiddetto scudo penale alla possibilità di adottare un provvedimento *ad hoc* per garantire la protezione sia dei soci dell'azienda sia di futuri acquirenti relativamente all'attuazione del piano ambientale normato da un DPCM. Del resto, quale imprenditore sano di mente si sarebbe accollato l'industria in quello stato, senza un minimo di tutela? E qui dal corto circuito arrivano le comiche, sempre perché i comici ci piacevano. A gara conclusa, ad avvenuta aggiudicazione, l'allora ministro pentastellato dello sviluppo economico Luigi Di Maio, con la teatralità e la propaganda che accompagnavano i proclami di quell'Esecutivo, chiese di avviare una verifica per la revoca dell'assegnazione, nonostante l'Avvocatura dello Stato avesse ribadito la regolarità della procedura. Non solo. Non contento, lo stesso Di Maio, sull'onda di quello che si è detto, diffuse il messaggio sbagliato che il Governo avrebbe potuto revocare la gara, in presenza di altre aziende interessate. Quello stesso Governo da una parte interloquiva con gli amministratori per una giusta garanzia sull'esecuzione del piano ambientale correlato all'acquisizione del bene e dall'altra, a grandi colpi di *slogan* che li caratterizzavano, dichiarava che non avrebbe mai concesso lo scudo penale, per non offendere la memoria dei morti e i disastri ambientali perpetrati. Presidente, qualcuno glielo spieghi che la garanzia avrebbe operato *pro futuro* e non per il passato; quella garanzia sarebbe stata - perdonatemi la ripetizione - una garanzia per rispettare la memoria delle famiglie che piangevano i morti, per il rione Tamburi e per la città di Taranto. E siccome al peggio non c'è mai fine, il ministro del Sud della maggioranza pentastellata Barbara Lezzi, in perfetta sintonia con le dissennate azioni governative, avanzò l'idea che un colosso industriale potesse essere sacrificato sull'altare delle cozze, perché l'economia locale avrebbe potuto reggersi e riconvertirsi negli allevamenti di mitili. Per questo io non vi citerò più i banchi a rotelle, ma mi dedicherò ovviamente alle cozze. Sulle cozze, inoltre, la Ministra del Sud ha una posizione tutt'altro che isolata, che anzi viene avallata dal collega di partito e deputato tarantino Giampaolo Cassese. Questa è storia, purtroppo, e spiace constatare che oggi coloro che hanno contribuito a questi disastri preferiscono a un dignitoso silenzio la difesa delle loro scriteriate decisioni. Ma anche per chiedere scusa ci vuole serietà, quella che plasticamente è mancata in tutto questo percorso condito da scelte prive di prospettive e dal rimando ad altri, come sempre, della responsabilità di risolvere il problema. In questa confusione di ruoli e in questa assenza di una rotta è sicuramente mancata quella stabilità che rappresenta il minimo comun denominatore per attrarre gli investitori. Con ciò non si legittimano le prese di posizione dei privati, perché non è questo quello che il Governo Meloni intende fare con il provvedimento in esame. È in questo perimetro che colloco una riflessione pubblicata peraltro sulla pagina economica del «Fatto Quotidiano», poche settimane orsono. La soluzione, sostiene il giornalista, è che il Governo attivi la procedura di commissariamento, anche in ragione della pronuncia del tribunale di Milano, che ha respinto l'ipotesi di un concordato in bianco proposta dai privati. Esattamente quello che il Governo aveva già *in fieri* e che farà; volontà appunto esplicitata nel testo normativo in discussione. Il Governo Meloni decide e non palleggia le decisioni a discapito dei territori. All'articolo 1 viene prevista la possibilità, in caso di inerzia dell'organo amministrativo delle società, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico. Tale possibilità era prevista prima solo per il socio pubblico, mentre ora viene attribuita anche ai soci privati. Uno stanziamento di fondi per cinque anni, determinato dall'articolo 2, andrà a sostenerne la continuità aziendale e a contribuire ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente nei pressi degli impianti e la sicurezza dei luoghi di lavoro, che per troppi decenni sono stati un vergognoso *vulnus* non solo della città di Taranto, ma di tutta la nostra penisola. La problematica dell'Ilva ha coinvolto e coinvolge infatti anche un'innumerevole serie di medie e piccole realtà di tutta Italia, fornitrici di beni o servizi, che sono rimaste creditrici per lungo tempo e che perciò si trovano a scontare una grave crisi di liquidità. Penso ai trasportatori e agli spedizionieri goriziani o ai terzisti liguri, che in certi casi ancora stanno aspettando le liquidazioni del precedente commissario. Anch'essi in questa misura diventano destinatari di una particolare tutela all'articolo 2-*bis*; nello specifico, dietro determinate condizioni, viene garantito loro l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'ultima forma di tutela che voglio menzionare, con riguardo a questo decreto-legge in fase di conversione, spetta ai lavoratori, per i quali all'articolo 3 è prevista la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione. In questa infinita storia di passi avanti e passi indietro, i lavoratori sono sempre stati le vittime reali e i veri sconfitti. È giunto finalmente il momento di riportarli al centro e la misura indicata in questa disposizione certamente offre un contributo verso tale essenziale obiettivo. E lo fa, ancora una volta, il Governo Meloni: amministrazione straordinaria, dunque, ma con tutele importanti verso l'ambiente, la sicurezza, creditori e lavoratori, anche perché Taranto non è solo Ilva, ma è anche agricoltura, turismo, persone, esseri umani. Chiaramente, non è che mi conforti la condivisione con il principale organo della propaganda pentastellata che vi ho citato prima, perché non è su questo punto che nasce il provvedimento in esame. Certo è che talvolta, ma non sempre, la resipiscenza conduce a buon senso anche coloro i quali, sfidando il senso del ridicolo, volevano sostituire ferro e acciaio con le cozze, i tarallucci e l'alpinismo sportivo al mare.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, parto dall'intervento, concluso appena adesso, della collega di Fratelli d'Italia, che ha terminato dicendo che l'Ilva non è solo Taranto: che è l'Europa, è l'Italia. Innanzitutto, mi fa piacere venga ricordato che l'Ilva non è solo Taranto. Noi abbiamo audito il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, perché l'Ilva è dislocata in tutta

È una domanda di rito, perché la risposta è sicuramente no. Allora, quello che ci stupisce, di questo anno e mezzo,

Lo so che ArcelorMittal offriva tanti soldi - come ci ha ricordato l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia - ma nell'altra cordata, quella perdente, c'era lo Stato; Stato che poi, in qualche modo, ha dovuto rientrare, finanziando e dando una serie di risorse, che però non hanno contribuito a un rilancio industriale del Paese, per molte questioni: dalla mancanza dello scudo penale, a un certo punto, con il Governo gialloverde, all'intervento del tribunale che, tra salute pubblica e produzione industriale, ha preferito, giustamente, la salute pubblica, chiudendo la produzione di parte dei forni. Quindi, una serie di concatenazioni ed una serie di cause che sicuramente non hanno un unico responsabile o un unico colpevole, ma che hanno, in questo periodo, affaticato ancora di più un'azienda che, di fatto, passava dai Riva al miglior offerente, in una situazione di grande difficoltà; difficoltà in primo luogo ambientale, perché la salute dei cittadini di Taranto, e non soltanto dei cittadini di Taranto, deve essere la preoccupazione principale di tutti noi e non si può chiedere di sacrificarla per dei posti di lavoro. Ma la transizione della produzione dell'acciaio verde è arrivata troppo lentamente e senza una visione industriale. Vengo al decreto in esame. Anche questo decreto è interlocutorio, perché anche in questo decreto non c'è una visione una visione di cosa vogliamo fare di Ilva al posto del commissariamento. Certamente, il commissariamento è una soluzione provvisoria, che serve a rilanciare un'azione, ma non si riesce a vedere quale sia l'azione. Devo dire che, anche dalle parole

un eccesso di severità nell'accesso ai fondi da parte dei fornitori. Venivano chieste delle percentuali che avrebbero determinato di fatto il fallimento. Ricordiamo infatti che, oltre all'Ilva e ai suoi lavoratori, oltre ai lavoratori che sono in Piemonte e in Liguria, ci sono dei fornitori che per anni hanno fornito l'opera a questa azienda e che non hanno ricevuto in questi anni alcuna retribuzione del lavoro fatto. Invece di dare la possibilità a tutti

la mancanza di visione complessiva: è arrivato a fine gennaio e ogni settimana venivano presentati degli emendamenti che, di fatto, riscrivevano il decreto originario. Questo sicuramente per la complessità

Visto che si tratta di lavoratori di società che rischiavano il fallimento e che c'è un tentativo di trovare una soluzione, noi, come Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, ci asterremo e il collega spiegherà spiegherà il perché. Ci asterremo per senso di responsabilità nei confronti delle persone che oggi chiedono una risposta al Governo, e non perché profondamente convinti da quello che c'è scritto nel provvedimento in esame. Ripeto

un tentativo anche da parte dell'Europa di fare una concorrenza sleale nei confronti del nostro Paese e della nostra produzione di acciaio. Però delle Però delle due l'una: o siamo tornati protagonisti in Europa o non lo siamo. Se ogni tre per due si dice che siamo tornati protagonisti in Europa,

noi non riusciamo neanche a sederci con tanta convinzione ai tavoli europei, soprattutto quelli che riguardano l'industria, allora bisogna dirlo chiaro e tondo e bisogna trovare una soluzione anche con l'aiuto delle opposizioni. Voi sapete che non abbiamo mai fatto ostruzionismo; che non abbiamo mai posto in essere questioni solo per avvantaggiarci dello che ci interessa sicuramente il Paese. Proprio perché ci interessa il Paese e la sua serietà, non siamo disposti a considerare questo decreto come la soluzione di tutti i mali. Anzi, è ancora troppo interlocutorio per dare una risposta risolutiva all'Ilva e penso che lavoratori, sindacati, Taranto, la Liguria e il Piemonte aspettino invece soluzioni più definitive.

la conversione in legge di un decreto-legge avente lo scopo di rilanciare il complesso industriale dell'ex Ilva, continuando tuttavia ad intervenire con testardaggine in modalità senso unico, offrendo soluzioni che si collocano esattamente nel solco di tutte le azioni dei Governi precedenti, che di fatto non hanno mai funzionato e stanno condannando il complesso industriale dell'ex Ilva a un processo di eutanasia insostenibile. La logica industriale percorsa è stata sempre quella di garantire la produzione, costi quel che costi, a scapito dell'ambiente, della salute, della riconversione del polo produttivo, della riqualificazione dei lavoratori e della stessa produzione, logica fallimentare. perché la produzione non è aumentata a seguito di tutti gli interventi statali, bensì è diminuita nel tempo. Mi pare questo un chiaro e inequivocabile segnale che la strategia politica industriale non abbia funzionato, che l'ex Ilva, emblema di progresso e di riscatto per tutto il Mezzogiorno, sia oggi diventata drammaticamente un simbolo di inquinamento, malattia e morte. Poco più di un anno fa, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo dichiarato la nostra netta contrarietà ad un provvedimento salva-Ilva privo di una reale e concreta progettualità di rilancio, anche in chiave ambientalmente sostenibile, della produzione d'acciaio; un decreto tampone quello di un anno fa, un decreto tampone quello di oggi, che invece di agire un vero cambio di rotta fa di nuovo perdere tempo e allunga l'agonia ambientale, economica e sociale che si trovano a subire ingiustamente i lavoratori dell'ex Ilva, i cittadini tarantini, l'indotto e lo stabilimento stesso. Un atto inutile quello dell'anno scorso, inteso ad imbavagliare la magistratura, reintroducendo lo scudo penale che priva i giudici del potere di porre sotto sequestro gli impianti di produzione, quand'anche questi siano dichiarati pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ha funzionato il decreto? Sta salvando l'ex Ilva? Non mi pare e purtroppo, nella triste consapevolezza e rassegnazione degli stessi proponenti, avrà stessa sorte anche il provvedimento che stiamo per votare oggi. Ancora una volta, dinanzi ai sacrosanti e giustificati appelli di aiuto di coloro che vivono in una zona di sacrificio, a Taranto, città tra le più inquinate al mondo, dinanzi al rischio di perdere il lavoro e di vedere definitivamente in ginocchio tutto l'indotto, il Governo Meloni risponde in modo davvero unidirezionale e povero di slancio innovativo, cioè con la solita nuova iniezione di capitali per far fronte allo stato di insolvenza dell'azienda, ormai priva di liquidità e totalmente incapace di sostenere economicamente i costi produttivi e occupazionali dello stabilimento; tutto ciò senza contemplare una concreta misura di risanamento e riconversione ambientale dei processi di produzione dell'acciaio. La situazione che questo decreto-legge cerca maldestramente di risolvere oggi è la stessa che si era tristemente profilata nelle audizioni svolte l'anno scorso in Commissione. Era ben chiaro a tutti che le difficoltà di ieri sarebbero diventate le difficoltà del domani, o meglio dovrei dire di oggi. Dunque, in presenza di un impianto ammalorato e dei sempre più gravi impatti sanitari ambientali che i cittadini tarantini stanno subendo, questo provvedimento punta a preservare unicamente la funzionalità produttiva dello stabilimento ex Ilva, chiaramente per un breve periodo; in attesa di Godot, mi verrebbe da dire. Il Governo non specifica, infatti, come intenda sciogliere oggi alcuni dei nodi più urgenti e dolorosi di questa faccenda: la salvaguardia dell'ambiente e della salute di coloro che ci lavorano e ci vivono e la politica industriale che si intende perseguire per il reale salvataggio di questo importante polo siderurgico. Siamo in *stand-by* per il piano industriale che arriverà, speriamo prima dei sei mesi annunciati per il più grande, obsoleto e inquinante stabilimento d'Europa, di cui - come ha riferito in Commissione anche il presidente di Confindustria - non si conosce nemmeno lo Stato in cui versano gli impianti in cui i dipendenti lavorano, si ammalano e subiscono incidenti sul lavoro;

delle polveri sottili rilevate nel 2023, drasticamente aumentate rispetto all'anno precedente, nonostante la produzione si sia ridotta. La mancanza di una valutazione di impatto e di danno sanitario causato dalle emissioni inquinanti dello stabilimento ha esposto ed espone tutti i lavoratori dell'ex Ilva e i cittadini di Taranto a rischi per la salute incalcolabili e francamente inaccettabili nel 2024. La mancanza di volontà di rispondere a questa emergenza umanitaria è un fallimento della politica anche industriale di questo Governo; una sconfitta, però, che non possiamo accettare e a cui dobbiamo anzi reagire, cogliendo tutte le opportunità che l'innovazione e la tecnologia ci offrono. Personalmente sono convintissima che l'Italia abbia tutte le carte in regola per cogliere questa sfida; serve però un deciso cambio di rotta. Sappiamo che la produzione di acciaio rappresenta un comparto produttivo strategico ed essenziale per il settore manifatturiero italiano, che, per qualità e produzione, si attesta alla seconda È indubbio che l'importanza di sostenere l'attività e la produzione dello stabilimento sia vitale non solo per mantenere stabili i livelli di occupazione, ma anche per garantirci come Paese un'indipendenza dagli altri grandi *main player* del settore, come la Cina. Per fare tutto questo è necessario trasformare il paradigma industriale che ne è alla base, attraverso un piano di decarbonizzazione che consenta di impiegare metodi di produzione a minore impatto ambientale. È quindi irresponsabile che il Governo continui a esitare nel cogliere le opportunità offerte dalla *green economy*, che rappresentano un volano di sviluppo economico, mentre altri Paesi le stanno invece cogliendo al volo. Anche nel campo dell'industria, l'ambiente non è un avversario ma un alleato che scende in campo a giocare la partita in un'ottica di progresso e innovazione utile e vantaggiosa per tutti, anche a livello occupazionale: una vera marcia in più e non un ostacolo come la destra ama raccontare. C'è quindi la necessità di procedere celermente con un'efficace riconversione dell'industria, promuovendo l'innovazione tecnologica con cicli produttivi che riducano l'uso delle risorse naturali, che incentivino la decarbonizzazione dell'impianto siderurgico e riducano anche le emissioni di anidride carbonica, consentendo risparmi sui certificati di compensazione ambientale del sistema europeo di scambio di quote di emissione. Si deve infatti ricordare che tra pochi anni, in accordo con la politica europea sul clima, le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio a ciclo integrale, con conseguenze negative inevitabili anche in termini di competitività economica e di occupazione. Un concreto cambio di passo potrà esserci se si avrà il coraggio di ridisegnare una nuova politica industriale, che sia collegata ed inserita anche nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima; un piano che ponga in relazione l'economia con il criterio della sostenibilità ambientale e l'obiettivo di mitigazione climatica e di coesione sociale. Inoltre, per ridurre le esternalità negative, ossia i danni creati dalle attività economiche sugli ecosistemi naturali e sugli esseri umani, i cui costi economici per l'Italia sono stati per il 2021 pari a circa 30 miliardi di euro, vi è bisogno di un sistema di incentivi fiscali che non solo vada a premiare la produzione, ma favorisca anche chi produce inquinando di meno. È tempo di agire, è tempo che anche al Governo avvenga una transizione culturale che dia rilevanza e sostanza al binomio ambiente-economia, per deliberare con maggiore efficacia, anche perché a lungo andare l'inazione della politica sarà fatale per la nostra economia. Non si può più continuare a produrre sulla pelle di Taranto e dei suoi cittadini. Le alternative ci sono e ogni passo sbagliato rappresenta un margine di tutela in meno e un grado di sofferenza in più per Taranto e per chi la vive, un costo umano troppo alto che non possiamo più sopportare e che noi in quest'Aula abbiamo abbiamo la responsabilità civile, morale e politica di fermare. Signor Presidente, rappresentante del Governo, per ben interpretare il destino di Taranto con i numeri che circolano e che coinvolgono l'ex Ilva, ho trovato estremamente interessante una citazione del Manzoni da «Ipromessi sposi»: «Chissà che imbroglio avran fatto laggiù, che cabale». Appunto: la cabala. In effetti, l'interpretazione di questi numeri delinea uno scenario impietoso e delirante, tanto da far ritenere normale che qualche giorno fa un giovane cantautore del luogo abbia deciso di girare all'interno della struttura il suo ultimo video per un brano chiamato «Il gran ballo di Satana», per esprimere come il male influisca sugli esseri umani a livello sia del singolo che della collettività e a Taranto, Presidente, di male se ne continua a fare, eccome, così come si continua a fare del male all'industria italiana. D'altro canto, colleghi, mi dovete spiegare quale sia la politica industriale di questo Governo, una politica che possa evocare un progetto valutato e ponderato e non un progetto erratico, frutto delle paure e delle connivenze del momento o, peggio, frutto di qualche *diktat* estero. Prendiamo l'*automotive*: prima no alla via della seta, che intendeva ricondurre i rapporti Italia-Cina all'interno di un perimetro di rispetto dei diritti da parte di Pechino; poi frettolosamente sì a una sorta di via della seta automobilistica, Stellantis vi rifila un sonoro schiaffone sulla produzione di auto in Italia e voi correte in ginocchio in Cina con il piattino in mano a trattare con tre operatori cinesi. Dov'è la coerenza? Lo stesso dicasi per le auto elettriche: prima auto elettriche no, perché trasformano la transizione ecologica in ideologica, come piace tanto dire alla Presidente del Consiglio; poi auto elettriche sì, con un disperato tentativo di trattativa con la super *guest star* di Atreju, ovvero Elon Musk e la sua Tesla. E ancora, prima il taglio dei crediti di imposta per Transizione 4.0 per l'innovazione delle imprese, una delle principali leve della crescita italiana del biennio 2021-2022, crescita che voi avete azzerato tra il 2023 e il 2024; poi, il disperato recupero del piano, ora ribattezzato Transizione 5.0, quando vi siete resi conto del colossale errore rappresentato dal suo precedente affossamento. un nuovo piano Transizione 5.0, peraltro peggiorativo rispetto al nostro Transizione 4.0 in termini sia di fruibilità dei crediti di imposta da parte delle imprese, sia di non cumulabilità con altri *bonus*, per esempio quelli della ZES unica. A denunciarlo è stato quell'incredibile giornale a cinque stelle che è «Il Sole 24 Ore», pensate un po'. *(Applausi)*. Ma non stupiamoci del deterioramento economico che questo casuale, improvvisato e subalterno *modus operandi* sta provocando.

che caratterizzerà, secondo tutti gli osservatori, anche il 2024, con un dimezzamento delle velleitarie previsioni di crescita fatte dal Governo, una produzione industriale che ha fatto segnare un allarmante meno 2,5 nel 2023, dopo un incredibile *record* negativo di undici mesi consecutivi di calo della produzione industriale stessa su base tendenziale. Lo Stato italiano, Presidente, per circa dieci volte ha destinato i soldi pubblici al sito pugliese, senza garanzia alcuna, sia per i lavoratori che per l'indotto e senza avere in mano un progetto industriale valevole. Nel 2022-23 addirittura si è trattato di un prestito di 680 milioni di euro per saldare alcune importanti partite debitorie aperte tra costi delle energie e imprese dell'indotto. Dalla dichiarazione di insolvenza arrivata dal tribunale fallimentare di Milano con relativa conferma dell'amministrazione straordinaria, potrebbe aprirsi anche un'inchiesta per verificare le possibili evidenze e i possibili indizi di bancarotta presenti lungo il percorso che ha portato Acciaierie d'Italia fin qui. Proprio a tal proposito, auspichiamo fortemente che si faccia piena luce sulla gestione economica e sui conti dell'ex Ilva. Ricordiamo che la maggior parte delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia ha erogato dello stipendio dei mesi scorsi solo e soltanto acconti e che pochissime di esse hanno pagato per intero e inoltre che ci sono ancora diverse aziende che devono saldare la tredicesima. Auspichiamo fortemente di comprendere come si sia arrivati a questa catastrofe e soprattutto fortemente chiediamo che vengano accettate tutte le eventuali responsabilità del caso, senza scudo penale che tenga, perché con la vergognosa reintroduzione dello scudo penale è stato scoperto l'altarino. Lo scudo penale è sempre stato una via d'uscita per ArcelorMittal e per le forze politiche che hanno sempre sostenuto la continuità produttiva a carbone ad ogni costo, anche a discapito della salute dei tarantini e dei lavoratori. Mittal è entrata in gioco sull'ex Ilva solo per sottrarre commesse alla concorrenza, ma non di certo per il rilancio di Taranto e nemmeno per investire sulla società. Era una pagliacciata affermare che la decisione del colosso di investire o meno dipendesse dallo scudo penale. Mittal, uscendo da Acciaierie d'Italia, ha dimostrato la sua assoluta inaffidabilità. Il decreto-legge ex Ilva varato da questo Governo è ostico, mendoso e nulla risolve. Vengono riesposti i consueti problemi nel decarbonizzare una volta per tutte l'acciaieria, si persevera in logiche industriali desuete, incentrate ancora sul carbone, senza considerare che l'impianto è in parte sotto sequestro per disastro ambientale e nella totale assenza di tutele ambientali e sanitarie, oltre che in penuria di una politica mirata a favore della riconversione economica, sociale e culturale della città. In altre parole, si continua ad insistere sulla possibilità di distrarre importanti risorse a favore del ciclo produttivo, avvantaggiando diverse società controllate da privati invece che accelerare e aprire cantieri dalle tante risolutive e bonifiche su cui il Governo dimostra la totale noncuranza. Si tratta di una riconversione economica, sociale e culturale della città duramente rallentata, ma avviata con il cantiere di Taranto nel corso del Governo II, un piano strategico che offriva ristoro alla comunità e rilanciava il territorio utilizzando tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l'occupazione e avviare la riconversione. Si trattava di una complessa sfida che coinvolgeva valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l'ambiente, tutti meritevoli di tutela senza che la tutela dell'uno potesse sacrificare gli altri, convinti fortemente che i processi di ristrutturazione o riconversione del tessuto industriale e delle infrastrutture di una determinata area geografica potessero essere portati a compimento solo attraverso politiche coordinate e sinergiche, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, *in primis* il Governo, le associazioni di categoria, i comitati locali e tutte le forze produttive del Paese. Un disegno di legge è questo dell'ex Ilva fonte di enormi dubbi e di grandi nodi, come quello del futuro dei lavoratori portuali. Dal 31 marzo oltre 300 lavoratori del porto si troveranno senza tutele salariali per non essere stato prorogato il funzionamento dell'agenzia per la somministrazione del lavoro e per la riqualificazione professionale. Tali lavoratori sono nel limbo da otto anni, ai quali era stata assicurata la riassunzione di tutto il personale nel lasso di pochi anni e data la garanzia di una proroga di due anni, che poi è diventata di soli tre mesi. Parliamo di lavoratori che attendono ancora lo stipendio di novembre, essendo stata quella di ottobre l'ultima mensilità percepita. Sono tutti i lavoratori specializzati, ai quali viene negata anche la possibilità di aggiornarsi e, nel caso, di essere assorbiti da altre imprese. necessario mantenere la clausola di salvaguardia che prevede l'assunzione dei lavoratori inseriti nell'agenzia prima di procedere a nuove assunzioni sulle sei iniziative imprenditoriali. ventiquattro mesi, anzi considerati i tre in corso ne servirebbero altri ventuno, vale a dire che basterebbe prorogare oltre marzo, anche perché le iniziative imprenditoriali non partiranno prima di dodici-diciotto mesi. Si tratterebbe di una misura di buon senso, altro che assistenzialismo. Alla fine si permetterebbe a queste persone, che hanno investito tanto tempo della loro carriera professionale, di guardare al domani con più certezze. Le difficoltà per l'ex Ilva in amministrazione straordinaria iniziano ad evidenziarsi ed è di pochi giorni, se non ore, l'annuncio delle aziende dell'indotto relativo allo stop del minuto mantenimento degli impianti e degli interventi urgenti che prevede anche nuovi licenziamenti, non essendoci sufficienti garanzie per il recupero dei crediti da parte di Acciaierie d'Italia. Nel dettaglio, di tutta l'attività emendativa del MoVimento 5 Stelle, Presidente, era stata accolta solo la possibilità di estendere anche alle microimprese dell'indotto l'accesso al fondo di garanzia delle imprese più grandi, ma non erano stati sciolti i nostri dubbi sulla possibilità dell'indotto di recuperare i crediti a seguito della scellerata decisione di aderire alla procedura di amministrazione straordinaria. Proprio perché da un incontro tra le aziende dell'indotto e altri istituti finanziari non sono arrivate sufficienti garanzie, garanzie, l'Associazione italiana di giuristi di imprese, che rappresenta l'80 per cento dell'indotto di Ilva, ne ha deciso il blocco, come volevasi dimostrare. Toccherà ora al commissario Quaranta scongiurare il peggio. Continua a spaventare che quella di Taranto, Presidente, sia l'unica acciaieria a ciclo integrale attiva sul territorio nazionale, la sola che produce acciaio dalla materia prima (minerale ferroso e carbone), attraverso cockerie e altiforni, il cosiddetto processo a caldo, il procedimento più inquinante, che provoca contaminazione profonda. Non saranno mai sufficienti le nuove prescrizioni su sicurezza, emissioni e reflui e nemmeno aver coperto i parchi minerali, giganteschi depositi di ferro e di carbone situati all'interno dell'ex Ilva, quelli da cui, con il vento, si alzava la polvere che avvolgeva la città. Serve una bonifica, anche una bonifica interna, per rimuovere decenni di scarto accumulati nei terreni e nelle falde. Il Governo su Taranto sta agendo in modo sgangherato e non risolutivo, per tentativi, Presidente. Naturalmente la colpa di tutto questo non è vostra, o della nostra inadeguatezza ed estemporaneità. No, la colpa è come sempre del superbonus o al massimo dei benzinai, della brigata Wagner, della Lagarde *(Applausi)* o degli enti attuatori, tanto per citare l'ultimo scaricabarile che avete fatto per giustificare la vostra incapacità a mettere a terra le risorse del PNRR. *(Applausi)*.

solo poco più di due anni fa il Paese viveva un disagio socio-economico crescente, dovuto all'incertezza politica e all'atteggiamento troppo attendista dell'Esecutivo, che puntava sulla tecnica del rinvio lasciando che i nodi si aggrovigliassero fino a diventare inestricabili: un Esecutivo che pensava solo a trattare in modo serrato con l'Europa per ottenere aiuti a destra e a manca. Ma, si sa, le aziende che sono sull'orlo del fallimento, e che rischiano di finire nella spirale dell'usura e preda dei circuiti malavitosi, non hanno né tempo, né la voglia di attendere i soldi europei. Si aspettano invece con ansia dal Governo scelte coraggiose e immediate, cosa a cui questo Esecutivo sta finalmente pensando. D'altronde, andrebbe fatta una riflessione: a chi conviene che l'Italia viva dei momenti di ambasce? Basterebbe tirar giù un elenco di tutte le aziende italiane che negli ultimi anni hanno cambiato bandiera e proprietà e contemporaneamente osservare chi ha comprato queste aziende e da quali nazioni. A quel punto la risposta risulterebbe molto semplice. Ma oggi l'Italia, e soprattutto la sua impresa, sta dimostrando di sapere il fatto suo; la crescita registrata negli ultimi mesi ne è testimone. L'Italia ha dimostrato e sta dimostrando di saper crescere, di saper affrontare anche l'inflazione e di avere imprese e, più in generale, attività produttive capaci non solo di resistere agli urti, ma anche di fare molto meglio degli altri. La sensazione è che la forza delle imprese italiane possa creare un certo disagio a parte parte delle opposizioni, come se l'obiettivo della crescita del Paese non fosse comune, ma valido eventualmente solo se c'è una certa sinistra a governare. Con il via libera della Commissione industria del Senato, il decreto in esame oggi consentirà l'ammissione alle procedure di amministrazione straordinaria per le imprese insolventi che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, non solo, come prevede ora la norma, tramite la cessione dei complessi aziendali, ma anche dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Oggi sigliamo una tappa importante della politica industriale del nostro Paese. Dopo un lungo lavoro siamo certi di aver imboccato l'unica strada, certamente difficile, ma assolutamente necessaria, per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia e d'Europa,

di accedere al credito per i debiti accumulati e di fruire del fondo di garanzia anche in mancanza di valutazioni creditizie particolarmente favorevoli. Con ulteriori modifiche apportate in Commissione è stato abbassato al 35 per cento il limite del fatturato prodotto nei confronti del committente. Il sistema Italia è in campo per vincere questa sfida fondamentale per l'industria e la manifattura di tutto il Paese. Ma, dal momento che ci troviamo a discutere ancora di Ilva, permettetemi un necessario quanto determinante passo indietro nella storia dello stabilimento, perché quanto mai chiarificatrice della politica che è stata di questo Paese. Quando, nel 1995, la famiglia Riva fu invitata ad acquistare l'ex Ilva, lo stabilimento perdeva quattro miliardi di lire all'anno. La nuova proprietà, dal 1995 al 2012, effettuò investimenti per 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 per misure di carattere ambientale. Queste operazioni sono state confermate da una sentenza del 2019 del tribunale di Milano, in primo grado ed in appello, e nel procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei fratelli Riva, successivamente assolti. Nessuno è mai stato in grado di provare che l'ex Ilva abbia violato le leggi sulla tutela ambientale all'epoca vigenti. vigenti. Lo stabilimento ex Ilva di Taranto non sta tirando le cuoia a causa di una crisi produttiva o di mercato. Non era un'impresa avviata al fallimento. Se vogliamo dare un nome a quella vicenda, potremmo coniare una nuova fattispecie di reato: procurato disastro industriale. Quell'impianto è stato coscientemente, premeditatamente e del tutto volontariamente pugnalato da una congiura su mandato delle *lobbies* ambientaliste e di intesa con ben individuate istituzioni e forze politiche locali e nazionali. I sindacati hanno subito e in parte condiviso quel disegno criminoso, perché incapaci di sottrarsi alla gogna del politicamente corretto ecologista e di opporsi a quanti brandivano sfacciatamente quel ricatto, in spregio di tutti i provvedimenti adottati dai vari Governi che hanno cercato di evitare la catastrofe. Va ricordato che, una volta espropriati i Riva dai magistrati pugliesi, i Governi Renzi e Gentiloni avrebbero dovuto trovare un nuovo *partner* affidabile per proseguire l'attività e garantire il risanamento ambientale. Nel 2017 il ministro dello sviluppo Carlo Calenda diede il via libera all'offerta di ArcelorMittal, scartando quella della cordata Arvedi Jindal. Furono sufficienti neanche due anni per accertare l'indisponibilità indiana a farsi carico delle incombenze

Noi pensiamo l'opposto. Quando c'è una crisi, lo Stato ha il dovere di mettere in condizioni le imprese di fare economia. Il contrario non può mai valere. *(Applausi)*. Sarebbe una visione folle, che ci riporterebbe a un'ideologia del secolo scorso che è morta con la caduta del Muro di Berlino. Per anni, come se non bastasse, rispetto alla questione ex Ilva abbiamo dovuto anche subire un'ideologia perbenista e fintamente al servizio dell'uomo, che non fa nient'altro che tendere ad alimentare l'antinomia tra la protezione dell'ecosistema e lo sviluppo della produttività industriale. Gli amici del MoVimento 5 Stelle hanno sempre detto che non volevano quel mostro d'acciaio in Puglia, offrendo, come alternativa per oltre diecimila dipendenti, come ricordava anche la collega di Fratelli d'Italia, gli allevamenti di cozze pelose, come disse qualcuno di loro: e sarebbe bene non dimenticarlo. Se alle opposizioni dà fastidio la tutela dell'interesse nazionale e dell'Italia, se ne facciano una ragione, perché questo invece è il nostro solo obiettivo: evitare la paralisi delle aziende di interesse strategico nazionale. Lavoriamo su questo e per questo. A lungo abbiamo dovuto subire la mancanza di una cultura industriale nella nostra classe politica. In Italia, in qualche modo, un'ideologia antindustriale è sempre esistita e diffusa in varie aree geografiche e sociali, favorendo una stagnazione economica decennale che, a sua volta, ha rafforzato la suddetta ideologia. È ovvio che poi, *ex post*, i cultori dell'intervento di Stato, invece di criticare alla radice la propria impostazione, hanno sostenuto che erano le politiche adottate nel passato a essere sbagliate,

me. C'è un unico ponte più importante del ponte di Messina: è quello tra il dire e il fare e quest'ultimo ponte la Lega l'ha già costruito tanti anni fa. Con questo provvedimento e con tutti gli amici di tutto il centrodestra, questo ponte l'abbiamo reso più forte.

decreto-legge che stiamo discutendo è sicuramente necessario, ma non è sufficiente per affrontare la condizione drammatica in cui versa Acciaierie d'Italia. È una condizione che è precipitata fino al commissariamento deciso dal Governo nei giorni scorsi con la nomina di Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli. Rivolgiamo auguri di buon lavoro ai commissari che si affiancano agli altri commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria in atto dal 2015. Il commissariamento e l'amministrazione straordinaria derivano da una storia di errori, di ritardi, di inadempienze di errori, di ritardi, di inadempienze di Governi di ogni colore politico che si sono susseguiti in questi anni, e nessuna forza politica si può chiamare fuori, né chi sta oggi né chi sta oggi in maggioranza né le forze che stanno all'opposizione. Tutti devono assumersi la propria responsabilità. Errori, ritardi e inadempienze dei privati, ArcelorMittal, scelta nel 2017 con una gara, che si è via via disimpegnata rispetto al futuro di Acciaierie d'Italia, dello stabilimento di Taranto, degli altri impianti presenti sul territorio nazionale. Errori, ritardi e adempienze anche di questo Governo che è ormai in carica da sedici mesi e in tale lasso di tempo nel Governo Meloni hanno convissuto due linee politiche contraddittorie tra di loro, non compatibili e che di fatto hanno paralizzato un'azione coerente ed efficace del Governo per affrontare la situazione che poi è precipitata: c'era la linea del ministro Urso, da una parte, e conosciamo la sfiducia che il ministro Urso aveva ed ha verso il ruolo di ArcelorMittal, nonché le posizioni del Ministro sull'assunzione di responsabilità da parte dello Stato in questa vicenda; dall'altra parte, c'era la linea del ministro Fitto, che a un certo punto ha preso in mano il *dossier*, anche se teoricamente tale *dossier* doveva essere responsabilità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. A maggio 2023 il ministro Fitto si è imbarcato in una trattativa riservata a porte chiuse con ArcelorMittal, illudendosi di poter recuperare questo rapporto, fino alla firma di un *memorandum of understanding* a settembre, che è rimasto segreto che di fatto è finito nel nulla. Ora dobbiamo fare i conti con una condizione che - come tutti gli interventi hanno sottolineato - è estremamente difficile e drammatica, e drammatica, perché è in discussione una realtà di interesse nazionale. Quando entra in gioco l'interesse nazionale, credo che dovrebbero venire meno la demagogia, la propaganda, la propaganda, gli attacchi privi di fondamento; dovrebbe entrare in gioco l'interesse nazionale del Paese e un confronto serio e costruttivo sulle soluzioni praticabili per difendere questa realtà, per difendere i 20.000 lavoratori diretti e indiretti che vivono degli stipendi di Ilva, per difendere le imprese dell'indotto, per difendere il futuro dei territori interessati anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente, della salute e della sanità pubblica. pubblica. Oggi abbiamo una realtà la cui produzione è ai minimi termini, chiudendo il 2023 con meno di tre milioni di tonnellate, quando il punto di pareggio - lo dicono i piani industriali presentati in questi anni - dovrebbe essere a sei milioni di tonnellate, ed ha aperto un contenzioso legale che rischia di creare delle incognite nelle prossime settimane, particolarmente rischiose. Il decreto-legge che stiamo discutendo prevede una serie di misure che sono chiaramente insufficienti. Sono insufficienti i 320 milioni di prestito ponte previsti dall'articolo 2; sono insufficienti anche gli interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori e delle imprese dell'indotto; l'accesso al fondo di garanzia dell'articolo 2-*bis*, il contributo in conto interesse: misure utili, sia chiaro, signor Presidente, per dare una mano all'indotto e per cercare di risollevare una situazione drammatica, ma non sufficienti ad aggredire con efficacia i nodi che Acciaierie d'Italia ha di fronte. rispetto al testo iniziale il decreto-legge è migliorato, lo vogliamo sottolineare in questa sede. È migliorato innanzitutto grazie all'accoglimento di una serie di proposte presentate dai senatori e dalle senatrici del Partito Democratico. Voglio ringraziare il senatore Martella e gli altri membri della Commissione industria per il lavoro prezioso e costruttivo che hanno fatto *(Applausi)*. Si deve a loro e alle nostre proposte se oggi è previsto l'obbligo di presentazione di un piano industriale da parte del commissario entro sei mesi; se le misure a sostegno della liquidità verranno estese anche alle Mid Cap; se la soglia per accedere alla liquidità è stata abbassata dal 50 al 35 per cento di fatturato realizzato con Acciaierie d'Italia per le imprese dell'indotto. Si deve alle nostre proposte se è stata sbloccata e accolta nel decreto-legge l'idea avanzata dalla Regione Puglia di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati del bilancio regionale per aiutare le imprese dell'indotto e dare una mano all'economia dei territori interessati. Certo, servirà fare molto altro, servirà fare molto di più rispetto ai contenuti di questo decreto-legge se vogliamo salvare un *asset* strategico per l'Italia e fondamentale per il Mezzogiorno e per i territori interessati. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione: la posizione del Partito Democratico l'abbiamo ribadita in tutte le sedi e lo faccio anche oggi di fronte a quest'Aula. È chiaro, molto del futuro della siderurgia italiana dipenderà dalle scelte che matureranno in Europa. L'Europa con il *green deal* ha deciso un ambizioso piano di decarbonizzazione di riduzione delle emissioni e un settore *hard to abate* come la siderurgia è chiaramente impattato da queste scelte, ma deve essere accompagnato con robuste politiche industriali che oggi non sono ancora in campo. Però è chiaro che, accanto a quello che l'Europa è chiamata a decidere, serve un piano nazionale per la siderurgia e serve fare le prossime scelte con un confronto sistematico e serrato con le organizzazioni sindacali, con le forze di opposizione, con tutte le istituzioni territoriali, perché questo è il momento di fare squadra se vogliamo garantire delle prospettive a questa realtà garantire delle prospettive vuol dire lavorare per la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti, Taranto, ma anche gli altri stabilimenti, dove è urgente fare lavori di manutenzione, innanzitutto per garantire la continuità produttiva. Serve difendere l'occupazione diretta, ma anche quella indiretta, e sono migliaia e migliaia i lavoratori che dipendono dal futuro di Acciaierie d'Italia e per questo è cruciale il sostegno delle imprese dell'indotto. Signor Presidente, ci arrivano segnali allarmanti dalle imprese dell'indotto, in particolare da quelle che lavorano a Taranto e in Puglia, sull'insufficienza delle misure previste da questo decreto-legge e noi invitiamo il Governo a fare di più rispetto a quanto è stato previsto. Poi è chiaro che nel medio-lungo periodo il commissariamento dovrà cedere il passo all'individuazione di uno o più *partner* industriali; in Italia abbiamo delle eccellenze nella siderurgia che possono dare un contributo decisivo per risollevare Acciaierie d'Italia. E bisogna, *last but not least*, come direbbero gli inglesi, rilanciare il processo di decarbonizzazione, che per noi era e rimane la via maestra per garantire la produzione, ma nel rispetto dell'ambiente, dei territori interessati e della salute dei cittadini che vivono a Taranto e nelle altre realtà dove ci sono gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Su tutto questo, signor Presidente, noi collaboreremo, come abbiamo già fatto in Commissione industria al Senato, nella difesa dell'interesse nazionale.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quella dell'Ilva è una storia secolare, è la storia del sogno industriale del nostro Paese, della privatizzazione e della contrapposizione tra il lavoro e l'occupazione, da una parte, e il diritto alla salute, dall'altra. È la storia della trasformazione dei territori, che da vocazione rurale acquisiscono una vocazione industriale. È la storia di tanti contadini e piccoli artigiani che sognano il lavoro in fabbrica, ma anche di tanti che avviano, come dei satelliti intorno a un pianeta, numerose aziende sussidiarie che oggi indichiamo come aziende dell'indotto. È anche la storia di una presa di coscienza di dati epidemiologici che disegnavano un quadro insostenibile in termini di prevalenza di patologie croniche e tumorali negli adulti e nei bambini e di incidenti ed infortuni sul lavoro anche mortali. In questo scenario si sviluppano sindacalizzazione e politicizzazione, con forti contrapposizioni tra chi si schiera radicalmente a difesa dell'occupazione e del lavoro e chi sposa, altrettanto radicalmente, la causa della tutela della salute e dell'ambiente. In tale contesto, pochi cercano un equilibrio tra questi diversi valori di rango costituzionale e molte campagne elettorali si giocano su questa contrapposizione.

Il resto è storia recente, con una gara che porta all'acquisizione di un socio privato nella formazione di questa società pubblico-privata, vissuta di contrasti tra il Governo Renzi e il ministro Calenda, da una parte, e il loro presidente di Regione Emiliano, dall'altra parte. Ricordo le campagne elettorali grilline che promettevano illusori parchi acquatici o tecnologici a sfondo turistico, salvo poi vedere il Governo Conte e il ministro Di Maio arrendersi all'evidenza. altresì forti tensioni che si svilupparono dentro il Movimento, tra la parte parlamentare e governativa e il movimento territoriale guidato dalla senatrice Lezzi, che ha inciso sullo scudo penale che tanti problemi ha creato in seguito. Fa specie

una scelta, una gara che poi ha portato alla scelta di quel socio privato. Così come fa specie sentire dai pentastellati citare il Manzoni su chissà quale imbroglio avete fatto laggiù. Questa domanda andrebbe fatta a Di Maio, perché sicuramente, all'esito di una campagna elettorale vinta sull'illusione di parchi acquatici, ha poi confermato il *partner* privato ArcelorMittal, quindi questa domanda andrebbe fatta proprio a loro. Non c'è stato senso di responsabilità nella parte pubblica; non c'è stata unanimità di intenti. Il privato ha capito di avere di fronte una politica debole e divisa e di questa debolezza ha approfittato con prepotenza, al punto da farsi beffa e sfidare lo Stato. In tutto questo è inutile dire che tutte le parti politiche hanno la loro colpa. No, noi orgogliosamente diciamo che noi non c'eravamo, mentre voi c'eravate in tutto quel periodo. Noi siamo arrivati nel 2022. Ce ne siamo occupati con il Governo Meloni, per il tramite del ministro Urso, dal primo giorno dell'insediamento, cercando il dialogo, sopperendo ad impegni non mantenuti da voi, immettendo risorse, assicurando lavoratori diretti e aziende dell'indotto, in una sintonia di ambientalizzazione e miglioramento dei processi più produttivi a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro. Abbiamo dovuto scontrarci con un privato che ha fatto della prepotenza la sua arma, sfidando lo Stato fino all'inevitabile rottura, ma l'ex Ilva per noi e resta vitale per l'Italia, per il suo PIL, per la sua immagine di Paese industriale, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per proseguire nel processo di ambientalizzazione, per soddisfare scenari di mercati presenti e futuri di richiesta di acciaio *green*. Allo spettro del fallimento abbiamo contrapposto la continuità aziendale, con la gestione commissariale affidata non a scelte di appartenenza politica in quanto tale, ma a persone di alta valenza tecnico-professionale. gli ultimi due mesi sono stati molto tristi per questa vicenda. Negli ultimi due mesi la situazione dello stabilimento ex Ilva è rapidamente precipitata a causa dell'indisponibilità del socio privato scelto da voi ad investire nell'azienda, a mantenere gli impegni. Sono stati avviate interlocuzioni negoziali tra Invitalia e ArcelorMittal, sulla cui positiva conclusione il Governo ha sino all'ultimo sperato. Non si parli di *memorandum*, non si parli di interlocutori inefficaci e inefficienti. Si parli invece di un impegno continuo, permanente per poter trovare una soluzione, ma ci si è scontrati contro il muro dell'indifferenza e della prepotenza. Subito dopo, quando ancora AdI era *in* *bonis*, il Governo, in via cautelativa, ha adottato altre misure di protezione dell'indotto e dei lavoratori con il decreto-legge finalizzato a favorire l'accesso privilegiato a condizioni di favore al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, con l'istituzione di un fondo per contenere i tassi di interesse sui finanziamenti per liquidità eventualmente attivate dalle imprese dell'indotto una terza misura che ha riguardato la cedibilità dei crediti dell'indotto. Per attenuare gli effetti negativi, si è in particolare prevista la prededucibilità dei crediti vantati dall'indotto e si sono create le condizioni di sistema perché tali crediti potessero essere acquistati da istituti bancari o società di *factoring* a condizioni vantaggiose, è intervenuta la reticenza del socio privato quando non ha voluto certificare i crediti delle imprese. Questa mancata certificazione dei crediti ha nuociuto al processo che era stato messo in piedi. Alla situazione di stallo, si sta sopperendo attraverso ulteriori misure, tant'è che il dialogo tra le aziende dell'indotto e i tecnici del Ministero continua in una misura permanente e continuativa. Abbiamo quindi reagito a questa prepotenza e allo stesso tempo le aziende e le imprese dell'indotto hanno fiducia, sono consapevoli che questo Governo non le abbandona, che sono allo studio misure sussidiarie e compatibili con le norme degli aiuti di Stato. Non posso esimermi dall'esprimere sentimenti di gratitudine per il lavoro certosino, equilibrato, responsabile, improntato alla moderazione e al dialogo svolto per conto del Governo dal ministro Urso e dai suoi collaboratori. È un ringraziamento che rivolgo al Governo non solo interpretando i sentimenti del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche dando voce ai tanti interlocutori che ho incrociato in questo difficile percorso, interlocutori che erano in continuo contatto e in continuo dialogo con il Ministero. So bene che gli effetti di questo decreto-legge - come dice qualcuno - potrebbero essere inefficaci o comunque poco risolutivi, ma saranno monitorati. Certo è che la volontà di questo Governo è la continuità

pretese delle aziende dell'indotto. La volontà di questo Governo è quella di ambientalizzare i processi produttivi per determinare tutela della salute e tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro. Per tutte queste ragioni,

Presidente, come forza politica, abbiamo presentato una serie di emendamenti a tutela delle imprese e dell'indotto, in particolar modo per consentire loro di tutelare i crediti già maturati e non pagati, andando a salvaguardare a salvaguardare la natura del loro credito come credito strategico e soprattutto a sostenere la possibilità di effettuare una cessione di credito *pro soluto*, per andare poi a riscuotere legittimamente il loro credito. Sul punto chiediamo al Governo massima attenzione perché ci sono oltre 500 imprese

banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto, come ripetutamente richiesto

l'emendamento originale aveva chiesto che il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunicasse il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Quindi non era stato neanche previsto che il commissario comunicasse il piano industriale. Questo emendamento è stato riformulato. Il Governo ha messo praticamente un un freno al fatto che venga considerato il processo di decarbonizzazione e, con i nostri emendamenti 1.202 e 1.203,

originariamente formulato e di accettare i nostri due emendamenti.

davvero questa è la dimostrazione che ci troviamo di fronte a una situazione dove non solo dal punto di vista produttivo e industriale manca un imprenditore, ed è quindi giusto fare l'amministrazione straordinaria. Però il problema è che questo ordine del giorno pone una questione: il progetto con il quale bisogna intervenire a Taranto deve tener conto di

Desidero, innanzitutto, ringraziare il Governo per aver accettato questo ordine del giorno ma, allo stesso tempo, la riformulazione e il parere favorevole a questo ordine del giorno sulla possibilità di cedere *pro soluto* i crediti testimoniano, ancora una volta, che le imprese dell'indotto non sono tutelate dal provvedimento.

che oggi i crediti dell'indotto non sono tutelati con la cessione del credito *pro soluto*.

con l'impegno che si è preso in questo ordine del giorno, la massima celerità. Ciò perché il ripristino della produzione dell'impianto per la banda stagnata ha delle esigenze, anche di carattere industriale e di mercato, che richiedono la più urgente attuazione di quanto previsto nell'ordine del giorno.

una delle due necessità: se io mantengo, attraverso la continuità produttiva, l'esistenza di una serie di imprese dell'indotto che devono garantirmi, in particolare, la produzione, la manutenzione e le attività che sono indicate nell'articolo, devo permettere che quelle aziende continuino a essere vive, reali e in grado di intervenire lungo il percorso di salvaguardia della continuità produttiva. Allora, io capisco che spesso ci si distrae, ma un'azienda è effettivamente in grado di intervenire in quel percorso di salvaguardia della continuità produttiva, se mantiene i lavoratori. Se i lavoratori non hanno la possibilità di rimanere legati a quell'impresa attraverso agli strumenti di conservazione del posto di lavoro e a quelli della cassa integrazione, noi facciamo un'affermazione che neghiamo successivamente. Siccome stiamo parlando, in generale, di imprese strategiche ai fini del Paese e, in particolare, sappiamo tutti che questo non è un decreto che riguarda genericamente le imprese da salvaguardare, ma riguarda il ciclo siderurgico, dobbiamo anche sapere che salvaguardare concretamente la continuità produttiva di un impianto come quello siderurgico

gli ammortizzatori della permanenza dei lavoratori e l'intervento sulla garanzia che deve esserci. Non può essere, così come invece viene indicato nell'articolo, che quando si arriva a 10 milioni i provvedimenti non ci sono più e quindi i lavoratori non hanno la tutela. Questo è un tema molto serio perché siamo un po' troppo abituati e lo siamo stati anche nella lunga gestione della vertenza Ilva - a pensare che si mettono a posto gli aspetti societari, le relazioni tra le imprese e le forniture di imprese, e poi tutto funziona. In realtà quella macchina funziona fondamentalmente se ci sono le condizioni di manutenzione degli impianti, di efficacia degli impianti, di alimentazione

un provvedimento che poi diventa la legge che regola la possibilità di ricorrere all'amministrazione straordinaria per le aziende a valore strategico, noi non possiamo costruire delle norme delle norme esclusivamente su misura di ciò che in questo momento, cioè prima della presentazione del piano industriale e quindi in realtà in un puro periodo ipotetico, immaginiamo che sia la necessità della continuità produttiva. Potremmo fare un riferimento alle esigenze che verranno determinate dal piano, ma siccome tale piano verrà presentato tra sei mesi, dobbiamo costruire una determinazione delle affermazioni che sia coerente e garantisca, nel caso dell'Ilva e negli altri casi che potrebbero esserci, di salvaguardare effettivamente la continuità produttiva. *(M5S)*. Signor Presidente, con riferimento all'articolo 2, vorremmo segnalare al Governo due proposte emendative. La prima riguarda l'introduzione della valutazione dell'impatto sanitario e ambientale con riferimento alla decisione del Governo di concedere la continuità produttiva in assenza di Inoltre si vuole condizionare il prestito di 320 milioni contenuto nel provvedimento al pagamento sia dei crediti dell'indotto, sia soprattutto alle manutenzioni dell'impianto.

*inserire le seguenti*:

drammaticamente errata.», impegna il Governo: a proseguire nel rafforzamento del monitoraggio degli effetti sanitari derivanti dall'esercizio degli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale attraverso la valutazione del danno sanitario di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.

trovato una soluzione e i lavoratori e le lavoratrici, da una parte, e i cittadini e le cittadine, dall'altra, hanno vissuto continuamente in una situazione di una situazione di incertezza e di peggioramento delle proprie condizioni di vita e di salute. Prima ho sentito un intervento in cui si parlava contro gli ambientalisti, ma vorrei ricordare che in quella zona del Paese

statalizzazione. In qualche modo bisogna fare questa cosa; se non lo si fa, continueremo a spendere i soldi dei cittadini e delle cittadine, però non risolveremo il problema. Per questa ragione chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno G2.5.

decreti che non hanno risolto il problema Ilva, cinque società che si sono avvicendate: Italsider, Ilva, nuova Ilva, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, due amministrazioni straordinarie, con il Governo Renzi e adesso con il Governo Meloni. Il MoVimento 5 Stelle ha subito quegli errori del passato e non è riuscito a rimediarvi. Oggi siamo Oggi siamo a chiedere, con questo ordine del giorno, la soluzione che è l'accordo di programma, con la nazionalizzazione della fabbrica, perché solo lo lo Stato può garantire gli investimenti necessari per la diversificazione tecnologica e industriale dell'impianto, per le bonifiche, per le tutele dell'indotto e dei lavoratori e soprattutto per l'introduzione della valutazione dell'impatto ambientale e sanitario. Chiediamo, quindi, al Governo

per la prevenzione delle patologie oncologiche pediatriche. Taranto è infatti ai primi posti per queste malattie legate all'inquinamento. Mi rivolgo al Governo, ma soprattutto all'Assemblea, al fine di istituire questo fondo che può aiutare i bambini del quartiere Tamburi a prevenire malattie oncologiche e pediatriche.

volevo segnalare una dimenticanza del Governo con riferimento alle tutele che vengono date come garanzie alle PMI. PMI. Il Governo ha dimenticato che oltre alle piccole e medie imprese, il tessuto economico soprattutto nel Meridione e a Taranto è formato soprattutto dalle microimprese. microimprese. Chiediamo attraverso questi emendamenti che le garanzie e le tutele che sono riservate a titolo di garanzia sui crediti vengano estese anche alle microimprese.

Se volete lo accantoniamo, però ditemi voi. Senatore Scalfarotto, non lo so. Presidente, le chiedo di sottoscrivere questo ordine del giorno, a nome di tutti

confluire si intende una riformulazione del mio emendamento nel senso di quello del senatore De Carlo. È una cosa che non va esattamente incontro alle esigenze che noi avevamo posto. Il nostro emendamento era molto più estensivo e dava la cassa integrazione per tutta la durata delle

Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024. 1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Signor Presidente, vorrei ovviamente ringraziare il Presidente e il relatore. Mi sembra che quasi tutti i Gruppi abbiano apposto la firma spiegare che la proposta emendativa nasce dalla necessità di risolvere un problema storico per la parte sud orientale della Sicilia, in quanto storicamente il porto di Siracusa non ha fatto parte dell'Autorità portuale di sistema della Sicilia orientale che va da Catania a Pozzallo. Con questo emendamento -

il tema del rilancio dell'attività portuale della Sicilia e delle isole in particolare, perché adesso le Autorità possono essere fonte di attrazione, come sappiamo, di investimenti del PNRR e della nuova programmazione europea. Successivamente vorremmo intervenire con altri provvedimenti per riformulare anche le regole della *governance* di queste *authority* che sono molto antiche (risalgono al 1994). In particolare, almeno per le isole,

intervengo per tranquillizzare e confermare che, con la stessa sensibilità con la quale abbiamo lavorato agli emendamenti e agli ordini del giorno sia dell'opposizione che della maggioranza, ci siamo presi un supplemento di riflessione per vedere di riuscire ad approvare anche l'ordine del giorno G2-*quater.*200, a beneficio di tutti. Si sono spesi otto minuti del prezioso tempo del collega Patuanelli, ma sono sicuro che capirà che è avvenuto per una giusta causa.

Ilva. Ci portiamo appresso questa storia ormai da anni. È una vicenda che ha attraversato diversi Governi. Alcuni Governi hanno fatto bene, hanno provato a fare cose giuste, altri hanno fatto colossali errori. Fatto sta che l'Ilva, come ha sottolineato anche il collega e segretario di Azione Calenda, è diventato il paradigma dell'Italia, di ciò che non funziona, degli scontri ideologici, dell'incapacità a rendere sinergiche la transizione ecologica e le politiche industriali. trattava di una gara vinta con un contratto blindato, che prevedeva 4,2 miliardi tra investimenti e prezzo, cinque anni di sorveglianza, l'impossibilità di licenziare i lavoratori, con tutti i livelli retributivi riconosciuti. Una gara che non consentiva ad ArcelorMittal di disattendere gli impegni è stata travolta invece da un Governo che ha avuto la brillante idea di cambiare il perimetro legale e di far saltare l'accordo con Mittal, con la complicità di chi votò a favore dell'abolizione dello scudo penale. Cancellando lo scudo penale con un tratto di penna si è consentito ad ArcelorMittal di sottrarsi ai suoi impegni, come ha confermato anche il ministro Urso in Parlamento. Ecco quindi come trasformare una grande opportunità per Taranto, per il Mezzogiorno e per l'Italia in un enorme problema economico e ambientale.

e, laddove ci fosse l'amministrazione straordinaria precedente *(Applausi)*, noi rischieremmo di mandare sul lastrico aziende sane. Questa è l'unica ragione

andare in malora a causa dell'amministrazione straordinaria oggi purtroppo indispensabile. Sappiamo che l'amministrazione straordinaria oggi rappresenta una soluzione ponte. Sappiamo bene che i 320 milioni di euro messi a disposizione dal MEF non sono la panacea di tutti i mali, ma possono servire a garantire la continuità aziendale, tutelare l'occupazione, a garantire la sicurezza dei lavoratori e a rilanciare un'azienda che politiche dissennate hanno spesso usato solo per la campagna elettorale. Azione quindi, come ho detto, voterà a favore di questo provvedimento, che non è sufficiente, ma è sicuramente un passo nella giusta direzione. Come ho detto prima, lo voteremo per tutelare le imprese dell'indotto, che vantano circa 140 milioni di crediti nei confronti di Acciaierie d'Italia; cifre importanti, che sarebbero diventate carta straccia a causa della procedura di amministrazione straordinaria. Si tratta di aziende che finora si sono sobbarcate, in condizioni tutt'altro che facili, l'onere di assicurare il funzionamento degli impianti, l'approvvigionamento di materie prime e la consegna dei prodotti. È stato infatti chiarito il perimetro delle aziende interessate e abbiamo anche noi lavorato agli emendamenti in Commissione con questo fine. Bisogna ora ovviamente consentire al commissario di avere presto a disposizione le risorse finanziarie che servono per non far spegnere gli impianti, per la manutenzione e il rilancio produttivo del sito di Taranto e di quelli ad esso collegati. È chiaro che gli errori commessi in passato pesano, ma oggi bisogna provare a ripartire, anche se è estremamente difficile. Fatico a credere che ci siano realtà pronte ad investire in Italia, in un settore come quello dell'acciaio, che deve fare i conti con norme europee particolarmente stringenti. Ma lo stabilimento di Taranto ha e conserva una valenza strategica per l'Italia, che non può fermare la produzione dell'acciaio E soprattutto noi diciamo: basta demagogia. È tempo di disegnare un futuro industriale per questo Paese e di uscire da una logica che vede l'industria sempre e comunque come sinonimo di inquinamento; una logica secondo la quale la protezione la protezione dell'ambiente non è compatibile con le politiche industriali. Noi pensiamo esattamente il contrario. È un fatto che solo in Italia l'acciaio e l'ambiente sono ritenuti incompatibili; va abbandonata questa scellerata visione culturale e pseudo-industriale del Paese. Dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di vivere non di *bonus* e di finti profitti, ma di politiche industriali. Per fare questo, la salvaguardia dell'ex Ilva un passaggio fondamentale, come consentire la produzione dell'acciaio in questo Paese. Abbiamo ascoltato e pure condiviso le parole del ministro Urso, ma ora aspettiamo il Governo alla prova dei fatti, perché la chiusura definitiva dell'Ilva sarebbe un fallimento tragico

sia direttamente, sia indirettamente, mediante la sua filiera composta da una pluralità di settori manifatturieri per i quali l'acciaio rappresenta la materia prima fondamentale. Colleghi, quando si parla di acciaio è inevitabile che si parli anche della tenuta di larga parte del tessuto produttivo della nostra Nazione, così come di Acciaierie d'Italia, azienda strategica per il nostro Paese, che con lo stabilimento di Taranto rappresenta l'acciaieria più grande d'Europa e dell'intero bacino mediterraneo. La crisi storica che sta attraversando l'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia - inutile dirlo - affonda le sue radici nel passato e dico che ha dei precisi nomi e cognomi, e non fate finta di non saperlo. Una crisi che questo decreto-legge porta invece finalmente a soluzione, dopo un *iter* ovviamente complicato, per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia. Un provvedimento d'urgenza che, tra l'altro, si pone in continuità con i precedenti due decreti varati in questi due anni dal Governo di centrodestra, volendo perseguire il massimo bilanciamento tra le esigenze di protezione della salute e dell'ambiente e quelle di tutela dell'occupazione e della produzione. Parametri, questi, che mostrano il segno dell'azione amministrativa di un Governo attento e lungimirante, come quello appunto guidato dal nostro presidente Meloni. Anche questa volta il nostro Esecutivo e questa maggioranza hanno voluto mettere al centro della propria azione l'interesse nazionale, garantendo la tutela dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. Venendo al provvedimento in sé, che ci apprestiamo appunto a votare, al centro dell'iniziativa del Governo c'è la continuità produttiva di impianti vitali per il nostro sistema produttivo, impianti senza i quali la nostra Nazione sarebbe irrimediabilmente più povera, più debole e, soprattutto, meno sovrana. Il provvedimento, infatti, rivede la normativa inerente la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, il cosiddetto decreto Marzano, prevedendo, in estrema sintesi, che il socio con almeno il 30 per cento delle quote societarie, in caso di inerzia del legittimato per gli stabilimenti industriali di interesse strategico ad ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. Faccio una precisazione non di poco conto. Questa norma non vale solo per l'ex Ilva. Di fatto amplia i diritti dei soci pubblici e privati delle aziende industriali strategiche che così avranno avranno la facoltà di richiedere l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria in caso di pesanti conflitti tra i detentori di quote proprietarie, volendo dare ulteriore corpo alle previsioni sull'accesso alla procedura già introdotte con il decreto n. 2 del 2023, approvato lo scorso anno. Nel caso di Taranto, grazie al commissariamento, significa rispondere tempestivamente alle preoccupazioni delle imprese della filiera, che hanno in questi anni, con difficoltà e sacrifici, garantito le forniture e la manutenzione dello stabilimento, nonostante le insolvenze delle varie proprietà. A questo proposito, il mio Gruppo parlamentare ha fortemente sostenuto una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste giunte dall'indotto in queste settimane di confronto e di ascolto delle loro esigenze. Mi riferisco, in particolar modo, ai parametri di accesso al fondo di garanzia e all'accoglimento della richiesta della Regione Puglia di svincolare quote di avanzo vincolato dall'amministrazione per ulteriori finanziamenti in favore delle imprese e della filiera. È così che questo decreto-legge realizza il perfetto bilanciamento e lo fa sapendo che, quando si parla di acciaierie, i valori in gioco sono proprio questi: produttività da garantire, lavoro, ambiente e salute. Valori che noi sosteniamo nell'equilibrio con cui vengono affrontati, senza prendere lezioni da chi ha dimostrato in passato di non dare valore all'Ilva, alla sua storia e alle sue potenzialità, che invece ancora rimangono. Per dare risposte al Paese, ai lavoratori e alle famiglie

La seconda è spegnere i forni di Taranto, licenziare la gente, far chiudere le aziende dell'indotto, iniziare a comprare acciaio altrove. Certo, questa seconda opzione sarebbe sicuramente quella preferita da chi ha interesse che l'Italia sia debole, impoverita e sempre più dipendente dagli altri. Ma non è così, né per noi né per il nostro Governo di centrodestra, con buona pace di chi, anche in quest'Aula, si commuove ancora alla retorica veterocomunista. In conclusione, signor Presidente, noi non abbiamo la pretesa di essere gli unici difensori dell'ambiente, della salute e del lavoro. Noi non abbiamo la superbia dei colleghi di certa opposizione che, a quanto pare, oggi sembra avere tutte le verità in tasca. Potremmo forse chiedere dove erano, quando si appoggiavano scelte scellerate per ordini di scuderia, ma noi non lo faremo. Presidente, noi non punteremo il dito contro nessuno, come fanno loro, ma non accettiamo nemmeno che dai banchi di certa opposizione ci vengano mosse accuse senza fondamento. Noi, al contrario, continueremo a correre, perché chi c'era prima di noi ha perso troppo tempo. Noi abbiamo una visione che abbiamo delineato chiaramente nel nostro programma, quello che gli italiani hanno scelto e votato. Abbiamo una strategia che ci guida e azioni che sentiamo il dovere di compiere. Il provvedimento, piaccia o non piaccia, fa parte di quelle azioni che ci stanno aiutando a raggiungere l'obiettivo di far tornare il nostro Paese, l'Italia, forte e soprattutto credibile nel mondo. È evidente, al contempo, che, sia per le aziende di interesse strategico dell'Italia sia per tutta la vicenda legata legata all'ex Ilva, niente è destinato a concludersi con la sola approvazione di questo decreto. Ci auguriamo, tuttavia, di restituire alle aziende la solidità necessaria per raggiungere la ripresa produttiva, che è una priorità da perseguire anche a sostegno di tutto l'indotto. Nessuno deve dimenticare in quest'Aula che l'ex Ilva rappresenta un *asset* produttivo di primaria importanza per il Paese ed è semplicemente folle anche solo pensare che possa essere andato perso, insieme ad altre infrastrutture strategiche che devono, a mio parere, essere di proprietà dello Stato, che poi viceversa privatizza i servizi. Per questo motivo, augurando al contempo un buon lavoro ai neo commissari nominati dal ministro Urso, che ringraziamo per la sensibilità e la vicinanza a Taranto, annuncio che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà convintamente a favore della conversione di questo decreto. Abbiamo di fronte una sfida epocale. Rispondiamo all'appello, ancora una volta con: siamo pronti.

in testa, che farà tutto giusto. Mi auguro per il Paese che sia così, ma credo che questo modo di esporre le cose finisca per essere un danno per la democrazia e per il nostro lavoro. In realtà il Governo segue un altro Governo, si fa carico di una situazione e lascia poi al Governo successivo l'onere di farsi carico della situazione che troverà: così funziona il mondo. Oggi affrontiamo una questione controversa e delicata, su cui nessuno è esente da colpe e responsabilità, però è un'occasione per fare tesoro della lezione vissuta negli anni passati. La principale lezione, a mio modesto parere, riguarda il rapporto tra lo Stato e i grandi gruppi privati, quando a essere in gioco è l'interesse nazionale. ArcelorMittal esce di scena e oggi si dice che il suo vero obiettivo era quello di indebolire lo stabilimento di Taranto. Mi si consenta qualche considerazione. ArcelorMittal è un colosso mondiale dell'acciaio che produce nei suoi diversi stabilimenti in tutto il mondo oltre 100 milioni di tonnellate di acciaio: più di tutta l'Europa messa insieme e circa il 6-7 per cento della produzione mondiale. Quando ArcelorMittal è entrato in Ilva, questa produceva e quindi vendeva più o meno 9 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Ora la produzione è scesa a poco più di 3 milioni, ossia a un terzo di allora. Non mi permetto di mettere in discussione l'operato dei diversi soggetti coinvolti dalla politica, dalla magistratura e dal *management*, ma è evidente che un tale calo della produzione, abbinato a sequestri che hanno improvvisamente impedito di assolvere impegni di fornitura assunti e ad annunci mediatici allarmanti sul futuro dell'impianto, non hanno aiutato a conservare la clientela. Anzi, questa appena ha potuto si è rivolta ad altri produttori di acciaio nel mondo. Ciò ha comportato evidentemente come conseguenza un drastico calo della produzione e del fatturato. L'incertezza sui tempi decisionali della nostra giustizia, poi, non ha certo aiutato ed ha sicuramente inciso sul venir meno dell'interesse di ArcelorMittal per Ilva. Del resto, in particolare noi del Gruppo Autonomie, che viviamo ai confini del Paese e quindi a contatto con territori stranieri confinanti, abbiamo ben presente quanto poco riusciamo a essere concorrenziali come siti per impianti industriali finanziati da capitali esteri, perché nessun imprenditore straniero è disposto a investire somme importanti in un Paese dove c'è la totale incertezza dei tempi del diritto. È facile dire ora che si è trattato di un'acquisizione ostile gestita in gran parte con i soldi del socio pubblico, cioè di tutti noi. Ma l'ostilità ora è indiscutibile anche a causa del nostro sistema Paese; ostilità che si è manifestata, da ultimo, con la richiesta di concordato in bianco pensata per bloccare il rilancio dello stabilimento e l'ingresso di nuovi privati. Un gioco fatto sulla pelle dei lavoratori, delle aziende dell'indotto, della salute dei tarantini e dell'interesse strategico che l'acciaieria di Taranto ricopre per l'industria italiana. Nel frattempo ArcelorMittal ha stretto un accordo con la Francia per investire 1,8 miliardi sulle acciaierie di Dunkerque, con lo scopo di ridurre le emissioni di carbonio. Con le premesse di cui sopra, c'era da aspettarselo. Se è vero che dentro il Governo c'erano due scuole di pensiero opposte, quella di chi voleva costringere il gruppo franco-indiano a mandare avanti lo stabilimento e quella di chi lo voleva mettere alla porta, penso che la strada non poteva essere che quest'ultima. La condizione è che ci sia - e purtroppo ancora non lo si vede - un nuovo piano industriale che consenta la ripartenza dell'azienda. La presidente Meloni si è detta contraria alla nazionalizzazione e in linea di principio siamo d'accordo, anche perché di tutto abbiamo bisogno fuorché che si torni ai tempi dello Stato imprenditore. Del resto, al giorno d'oggi è difficile pensare che lo Stato possa essere un imprenditore più abile di un privato. Ma è anche vero che, al netto di qualche indiscrezione giornalistica che parla di questo o di quel gruppo imprenditoriale interessato a entrare nella partita, ad oggi non se ne vedono all'orizzonte. L'invito che noi vogliamo e possiamo fare è che un'eventuale nuova gestione mista non ricada nell'errore del passato, quando il controllo era in mano al socio privato e le spese a carico del socio pubblico. Per arrivare a ciò serve che questa ennesima fase di transizione sia costruita con maniacale attenzione rispetto al mantenimento dei livelli produttivi, alla manutenzione degli impianti, alla sicurezza dei lavoratori, alla salvaguardia della capacità occupazionale, alla tutela dell'indotto al percorso di ambientalizzazione; il tutto dando modo al socio privato di guadagnare, perché un imprenditore fa impresa per guadagnare e non per perdere denaro. Purtroppo, il decreto che oggi discutiamo appare, con beneficio di inventario, appena sufficiente rispetto alla tenuta in campo di tutti questi obiettivi. Lo è per l'importo del prestito ponte, che garantisce la produzione solo fino a fine marzo, e lo è rispetto all'onorare le pendenze con le imprese dell'indotto, a cui non si può chiedere di andare oltre le loro possibilità, avendo anch'esse pendenze da onorare e lavoratori da pagare. Gli emendamenti *bipartisan* approvati in Commissione sono riusciti a migliorare alcuni aspetti: penso ai criteri per l'accesso al fondo di garanzia e all'estensione dello stesso alle piccole e medie imprese grazie al lavoro della Commissione. Ma quello che noi temiamo, Presidente, è che in attesa di un privato che tarda ad arrivare lo stabilimento perda ulteriormente capacità produttiva e veda assottigliarsi la sua forza lavoro. Questo magari perché qualcuno pensa che un'Ilva più piccola sia più gestibile, anche rispetto alle prospettive di ingresso di un socio privato. Ma se qualcuno lo pensa non sta solo prendendo in giro i lavoratori, ma sta anche facendo un drammatico errore: un'Ilva ridotta con alcuni altiforni spenti e produzioni abbandonate significherebbe aumentare la dipendenza nostra ed europea dall'acciaio straniero. La storia di questi anni, da quando cioè la Russia ha invaso l'Ucraina, ci ha sbattuto in faccia l'importanza di un'autonomia energetica e in tutti quegli ambiti legati allo sviluppo industriale. È chiaro che nessuno pensa a un modello autarchico, ma la sovranità di un Paese, concetto al quale l'attuale maggioranza è molto affezionata, passa da un certo grado di autosufficienza, quantomeno negli ambiti fondamentali, tutte cose che questo Governo sa benissimo. Mi riferisco alle costanti dichiarazioni del ministro Urso sulle materie prime critiche, dove addirittura preconizza una riapertura delle miniere dismesse; per non dire del braccio di ferro con Stellantis, a conferma che quella dell'Ilva si iscrive pienamente nella pagina difficile e importantissima del futuro industriale del Paese. Per tutte queste ragioni, Presidente, il nostro Gruppo oggi voterà a favore del provvedimento, pur conservando una serie di perplessità nel merito e sulla strategia che il Governo sta seguendo per sbrogliare questa difficile matassa. Votiamo a favore e lo facciamo con un augurio: su Ilva nessuna contorsione machiavellica. Parlate un linguaggio di verità coi lavoratori, con la città di Taranto, col sistema industriale del nostro Paese. Tutti devono prendersi il loro pezzo di responsabilità

Signor Presidente, sottosegretaria Bergamotto, colleghe e colleghi, parto dalla fine di questo mio intervento in dichiarazione di voto per dichiarare che, come Gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe, ci asterremo. Ci asteniamo perché riteniamo che il discorso di cui ci stiamo occupando, cioè la conversione in legge di questo decreto, tra l'altro prossimo alla scadenza, sia soltanto un elemento estremamente marginale di tutta la vicenda, ben più sostanziosa, di Ilva e dell'Acciaieria di Taranto e anche del ruolo dell'acciaio e della siderurgia nell'economia nazionale. La ragione per la quale il Governo ha dovuto deliberare e approvare questo decreto-legge è che, in questo anno e mezzo di vita, il Governo ha preso una decisione che è stata quella di andare all'amministrazione straordinaria. Ovviamente, avendo preso quella decisione, era necessario assumere una serie di decisioni a cascata per proteggere l'acciaieria e tutto l'indotto da quella decisione.

soprattutto se lo si fa quando si è azionisti di minoranza. Di conseguenza si introduce un elemento di instabilità, di inaffidabilità della Repubblica italiana come soggetto economico nel grande mercato degli investitori globali:

può abdicare alla sua responsabilità di socio, per rilanciare, per far partire, per far prosperare quell'impresa e può dire qualcosa del tipo: cari signori, no, io chiamo i commissari. Questa è una sconfitta, sottosegretaria Bergamotto, perché, comunque vogliamo etichettarla, l'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale, è un fallimento. La situazione diventa ancora più grave grave sapendo che Acciaierie d'Italia vanno in amministrazione straordinaria essendo soltanto le locatarie di impianti di un'altra azienda in amministrazione straordinaria. *(Applausi)*. Io non credo che esista al mondo una situazione nella quale il titolare degli impianti è in amministrazione straordinaria

Le aziende che hanno subito l'amministrazione straordinaria della prima azienda se lo ricordano benissimo, perché nelle procedure concorsuali - in tutte le procedure concorsuali - il meccanismo è quello del monte attivo patrimoniale, che poi si distribuisce come e quando nelle quantità in cui si potrà. Quando c'è il commissario si va dall'impresa che ha fornito i beni e i servizi e le si dice che

prendersi in carico la più grande acciaieria d'Europa non è una cosa che trova 100 concorrenti e dunque poteva esse l'una o l'altra cordata. Il problema era quello di gestire quell'investimento, quell'investitore internazionale (e che fior di investitore internazionale, perché ArcelorMittal non è l'ultimo arrivato) e farlo in modo adeguato. Purtroppo, però, il nostro Paese non lo ha fatto. Mi interessa poco attribuire delle responsabilità, però mi chiedo cosa avrebbe dovuto fare il Governo attualmente in carica, quello che si è candidato a risolvere i problemi degli italiani e sulla base di quello è stato votato e ha ottenuto la fiducia del Paese. Ora il Governo deve rispondere e non può dire: abbiamo ereditato, le cose

vi è da chiedersi - scrive l'autore - come mai, se a Taranto l'acciaio uccide, come molti integralisti sostengono, nel resto del mondo si producono miliardi di tonnellate di acciaio da impianti molto efficienti, senza fare stragi. Chi si pone questo interessante interrogativo è Davide Tabarelli, uno dei commissari che avete scelto per l'amministrazione straordinaria. Io sono d'accordo con lui, a parte il fatto che purtroppo a Taranto

sia possibile che per esempio a Linz, in Austria, ci sia una acciaieria più piccola che però produce acciaio quasi in centro città senza procurare quei danni. Si può fare l'acciaio in maniera pulita e compatibile? La risposta è sì, ci vogliono gli investimenti, ci vogliono i soldi e ci vogliono, per questo, gli investitori. *(Applausi)*. Signora Sottosegretaria, se il nostro Governo attuale è il Governo del ministro Urso, quello che dice di essere contrario alle multinazionali, capisce che trovare i fondi per mettere in sicurezza quell'impianto diventa molto difficile e ancor di più se poi si ricorre all'amministrazione straordinaria. La domanda è

se ci vorranno altri soldi, perché questa azienda ha tre miliardi di debiti e quindi con 350 milioni esattamente cosa ci facciamo? Mi viene da chiederle se sia normale che la fiscalità generale ripaghi i debiti di un'azienda privata, anche in presenza di un socio pubblico come il nostro. È normale che si prendano i soldi della Regione Puglia, per cui i pugliesi devono pagare di tasca loro le obbligazioni dell'Ilva? Le pare normale? Le chiedo che cosa si intende fare con i lavoratori: pensate di avere un piano per rilanciare le imprese e dar loro lavoro o avete eliminato il reddito di cittadinanza per dare poi la cassa integrazione a vita a queste persone? persone? Ci sono ancora 1.600 lavoratori della vecchia amministrazione straordinaria infatti che ancora aspettano di avere il lavoro indietro. Ci sottoponete un decreto di questo tipo che - ripeto - serve soltanto a gestire una decisione che avete preso voi, quella dell'amministrazione straordinaria, che non è un dato di realtà, cioè non ce l'aveva ordinato il medico, si poteva anche gestire la controparte, perché voi vi siete fatti prendere in castagna al punto tale che

uno dei più grandi esportatori del mondo, seconda manifattura del mondo, qual è il futuro di quello stabilimento e di quella acciaieria nelle mani del Governo Meloni, perché questo non l'abbiamo capito noi e non l'ha capito neanche il potenziale investitore che avete annunciato e che è ancora di là da venire.

Signor Presidente, premetto che non credo di avere nessuna verità in tasca, ma credo di conoscere un po'

delle acciaierie, considerato che il processo di ristrutturazione dopo la chiusura dell'azienda FAAC a Sesto San Giovanni mi ha visto purtroppo tra i protagonisti. quando ho sentito, nei giorni scorsi, il ministro Urso dire che l'Ilva deve diventare lo stabilimento più sostenibile d'Europa, oggettivamente ero molto contento, pensando che significasse affrontare seriamente una situazione che ha

In sostanza, quindi, la ragione per la quale votiamo contro questo provvedimento non è l'intervento di amministrazione straordinaria, scelta obbligata in questo momento. Di fronte al fatto che non c'è un accordo tra

Noi pensiamo che lo Stato debba giocare un ruolo fondamentale. Non deve escludere il privato, ma noi stiamo parlando in sostanza di una situazione che rischia di essere

devono vivere in tranquillità, poter andare a lavorare per vivere e non per ammalarsi. In sostanza noi stiamo affrontando un problema tra i più importanti.

da sedici mesi continuate a far ballare e a far capire e non capire, perché non si capisce assolutamente nulla di dove si vuole andare; il problema è questo. Qual è la prospettiva

senza far sì che il privato rischiasse; si è portato via il mercato, ma non ha investito. In sostanza la politica deve affrontare questo dato. Chi governa ha la responsabilità dato. Chi governa ha la responsabilità nei confronti dei cittadini di far capire dove vuole andare, in quale direzione intende marciare, quali soldi mette a disposizione e con quali tempi. Questo è l'altro dato fondamentale. Non possiamo continuare in questa

manteniamo a galla. Ma, se galleggiamo, rischiamo di continuare a depauperare la potenzialità dell'impresa, perché, se l'impresa non produce se l'impresa non è in grado di trasformarsi per rispondere alla questione sanitaria e alla questione ambientale, cioè ai problemi che ci sono nella città, fa dei passi indietro. Se non si investe sulla sicurezza, non si può continuare a produrre.

E voi venite a spiegarci che, in sostanza, ci sono quelli che pensano al sol dell'avvenire e via dicendo. Io no, io sono molto pragmatico e molto concreto: trovatemi un'impresa italiana, o anche straniera, che sia disponibile a venire qui, a fare una *partnership* con Ilva e a fare le cose che bisogna fare, cioè dare una risposta ai problemi che ho detto prima. Questa cosa non c'è, non esiste, e per questa ragione noi votiamo contro. Sottolineiamo il fatto che questa proposta sostanzialmente ci fa galleggiare

che ha detto che questi sono interventi che portano a galleggiare. Vorrei però ribadire, con certezza e con fermezza, che oggi finalmente, dodici anni e dopo tanti Governi che si sono alternati in questo periodo, c'è un Governo che interviene di petto sulla vicenda Ilva e che cerca di rianimare un paziente che, come viene detto, è quasi morto. Cerchiamo di farlo portandolo fuori dalla rianimazione e cercando di salvare 10.000 posti di lavoro. E la sinistra che fa? La sinistra sindacalista vota persino contro questo provvedimento, che cerca oggi di salvare i posti di lavoro. Ecco perché dico che posso capire tutti i giochi di parte della maggioranza e dell'opposizione in quest'Aula, però ci sono dei fatti concreti che vanno visti con grande attenzione. Voglio ribadire come solo due mesi fa ci siamo ritrovati in quest'Aula, perché due mesi fa, dopo numerose trattative, tavoli ed impegni tra il Governo e ArcelorMittal, finalmente abbiamo saputo (e certamente non abbiamo scoperto l'acqua calda) che ArcelorMittal non ha nessuna intenzione di investire un centesimo di euro sulla transizione dell'azienda verso la produzione di quello che noi crediamo invece si possa fare, cioè l'acciaio *green*. Due mesi fa, con il ministro Urso, siamo stati in quest'Aula ad analizzare la questione a chiedere appunto degli interventi. Oggi, a distanza di due mesi, siamo intervenuti subito e con tempestività sulla questione, con interventi concreti. È chiaro che c'è da fare tanto altro, ma lo vedremo successivamente. Però oggi noi interveniamo e lo facciamo - come dicevo - con determinazione. Auspicavamo già due mesi fa che lo Stato riprendesse in mano la situazione, vista l'indisponibilità

stesso. La dichiarazione di insolvenza ha dato il via libera al commissariamento e alla possibilità di concedere un prestito. Oggi abbiamo 320 milioni che servono,

che sono stati recepiti oggi in questi due decreti e che riguardano, in particolar modo, l'indotto, la possibilità di intervenire con il fondo di garanzia, come anche l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per sostenere l'impresa e la filiera. In questi due mesi di tempo abbiamo fatto due decreti, trovando e mettendo sul tavolo 320 milioni di euro, appunto all'Ilva. Abbiamo previsto misure a tutela della continuità produttiva e occupazionale anche per le aziende dell'indotto. Ci sono diecimila posti di lavoro da salvaguardare e noi non lo dimentichiamo, perché a Taranto sono legati anche i destini di altre due aziende e di altri due territori. Abbiamo fatto tutto questo in due mesi e dico a tutti i colleghi senatori che sono intervenuti, di tutti i Gruppi, che quindi qualcosa sicuramente l'abbiamo fatta. Ed ecco perché guardiamo in prospettiva alla futura possibilità di salvare ancora meglio l'azienda. Sono decreti, questi, che intervengono sui lavoratori

strategico aziendale importante per il Paese Italia. Come dicevo, bisogna certamente guardare anche al futuro, al fatto che oggi si può produrre acciaio *green*, perché è chiaro che nel 2024 non possiamo più tenere in conflitto diritto al lavoro e diritto alla salute. Quindi, questa è la possibilità oggi, di di produrre acciaio e di avere sul territorio un'azienda che guardi anche agli aspetti importanti della tutela ambientale. Abbiamo ricordato tutti le ferite e i sacrifici che il territorio, la città e la popolazione, hanno sopportato in tutti questi anni. La città di Taranto porta ancora

Ad oggi, il Governo mette sul tavolo, come dicevamo, due decreti-legge, la continuità dell'attività, 320 milioni di euro, ed è già attivo anche sul tavolo europeo per non permettere che la stessa azienda che oggi va via da Taranto,

già facendo sui tavoli europei che competono. Questo è un passaggio importante. Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni. Vorrei ribadire come in questi mesi - e lo ha fatto anche in questi anni - sulla vicenda dell'Ilva, dell'Ilva, il mio Gruppo parlamentare, Forza Italia, è stato sempre attivo. Personalmente vengo da quel territorio, sono pugliese, quindi a livello locale ho partecipato a numerose attività. l'indotto, così come ho incontrato l'azienda tante volte in passato; l'ho fatto e continuerò a farlo. Ho partecipato a tutti i tavoli ed è per questo che Forza Italia ha dato il suo contributo. Si chiude in questo momento un capitolo vecchio, ma si apre una nuova pagina che dà speranza e fiducia ai lavoratori e alle comunità, mettendo al centro, come dicevo, un piano industriale che preveda la tutela ambientale, la piena salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo. È per questo, con il nostro contributo,

che solo recentemente ha fatto una passerella a Taranto; a questo punto la sua assenza è una mancanza di rispetto nei confronti della città. *(Applausi)*. La complessità delle tematiche La complessità delle tematiche comportava anche la presenza del Ministro della salute e del Ministro dell'ambiente, dato che la tematica Ilva è complessa e si estende a diversi temi. temi. Con questo provvedimento il Governo attesta il fallimento della sua politica industriale. Il Governo ripropone, come il gioco dell'oca, un vecchio paradigma che abbiamo già sperimentato, quello del 2015 con il Governo Renzi, ovvero l'amministrazione straordinaria, che significa il fallimento dell'azienda. Questa volta però l'amministrazione straordinaria è è peraltro anche senza soldi. Inoltre il Governo con questo provvedimento va a proporre per l'ennesima volta il bidone di Stato, perché questo sarà poi il destino di tutti i crediti, di tutte le imprese e anche dei lavoratori, perché ci sarà l'ammissione di un fallimento e quindi l'incertezza di poter riscuotere i crediti. La gestione dello stabilimento Ilva di Taranto è stata sempre deficitaria e lo dimostrano le società che si sono avvicendate, le gestioni private e pubbliche che si sono susseguite: Italsider, Ilva, nuova Ilva, Ilva in amministrazione straordinaria, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Mantenere la fabbrica aperta e funzionante in questi dodici anni è costato agli italiani oltre 20 miliardi. Vorrei i crediti stralciati ammessi al passivo dell'ex Ilva dei Riva (oltre 6,5 miliardi di crediti ammessi al momento), le sofferenze oggi lasciate in eredità da acciaierie Italia, stimabili in base al decreto ultimo dell'ammissione alla all'amministrazione straordinaria (4,5 miliardi, come ha detto il Governo).

ci sono degli studi, da ultimo uno studio dell'università di Firenze, che li stima in 280 milioni annui. Vi sono poi i fondi sequestrati ai Riva, dirottati per garantire la funzionalità dell'impianto: ricordo i 150 milioni, che nel corso del Governo Draghi e con il nostro voto contrario tutte le forze politiche hanno destinato alla funzionalità. A queste spese sociali aggiungiamo i prestiti pubblici: solo quelli concessi dal Governo Meloni sono circa 900 milioni, che non recupereremo mai; le garanzie statali sui prestiti bancari, quelli sì che li avete protetti e garantiti, perché sapete che l'azienda non è bancabile e gli investimenti errati nella cosiddetta ambientalizzazione, che non esiste, perché questo è dimostrato dai dati ultimi sull'inquinamento. in tutti questi anni, soprattutto in questi ultimi dodici anni disastrosi, si sono susseguiti i sequestri giudiziari. Gli impianti Ilva sono tuttora sotto sequestro.

la sentenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. Vi sono inoltre gli interventi dell'Unione europea in termini di infrazione; l'ONU che definisce Taranto «zona di sacrificio»; l'OMS che ha ritenuto insostenibili quei livelli di inquinamento per l'essere umano. Tutto questo non è servito a nulla, non è bastato a porre fine all'accanimento terapeutico, perché questo è quello che la politica oggi fa con questo provvedimento. Noi, quando siamo andati al Governo, abbiamo subìto gli errori di quelle scelte del 2015, quando si è decisa l'amministrazione straordinaria e la continuità produttiva. È vero, non siamo riusciti a chiudere quell'impresa per gli errori commessi nel passato, però oggi è diabolico riproporre quel paradigma del passato, ovvero la continuità produttiva a carbone. Si invoca la strategicità dello stabilimento, ma - attenzione - nella letteratura scientifica economico-aziendale non esiste un'azienda strategica che realizza perdite che vengono trasferite ai cittadini italiani, perdite anche umane. Questo è soprattutto quello che accade a Taranto, che noi non possiamo accettare: malattie e decessi. Il Governo Meloni si sta assumendo delle responsabilità. Il gioco dell'oca adesso non produce più la responsabilità degli altri, ma è il Governo Meloni che si assume la responsabilità della continuità produttiva. Cosa ha fatto in questi diciotto mesi? Ha reintrodotto lo scudo penale, che era stato cancellato dal MoVimento 5 Stelle; ha annullato il progetto di nazionalizzazione, quello che noi stavamo cercando di fare nel corso del Governo Conte II, a salvaguardia degli investimenti e della chiusura delle fonti inquinanti, a salvaguardia e a tutela delle imprese e dell'indotto, dei lavoratori e dell'ambiente. Ha annunciato un *memorandum* con ArcelorMittal, che nessuno ha visto (e mi riferisco al ministro Fitto); ha cancellato il finanziamento di 1,2 miliardi di euro dal PNRR proprio sulla diversificazione industriale. poi bloccato i fondi della transizione equa, i 900 milioni; infine, ha regalato i 680 milioni di soldi pubblici, perché quello è un regalo che è stato fatto ad ArcelorMittal prima di dichiarare lo stato di insolvenza. a proposito di bidone di Stato, con questo provvedimento voi state trasferendo sul territorio una serie di perdite: oltre 200 milioni di euro per le sofferenze dell'indotto, che voi non garantite, perché non riconoscete la cessione la cessione *pro soluto* dei crediti; 500 imprese dell'indotto che oggi sono a rischio di chiusura; 5.000 lavoratori indiretti a rischio di licenziamento e per i fortunati anni di cassa integrazione, nella speranza, vana, di tornare un giorno a lavorare. Presidente, con riferimento ai lavoratori dell'indotto, le tutele per sole dieci settimane ci sembrano ridicole.

e il fatto che a breve la Commissione europea aprirà un fascicolo di infrazione, perché i due finanziamenti (di 680 milioni e 320 milioni) che state dando all'azienda sono illegittimi, il primo per la mancanza del piano industriale, il secondo sia per la mancanza del piano industriale, sia perché si sta finanziando un'azienda deficitaria, un'azienda in crisi, e abbiamo la certezza che i due finanziamenti non rientreranno. Dovete dire agli italiani il costo della vostra operazione. intervento con quello che ha dichiarato il ministro Urso nel corso della sua passerella a Taranto. Vuole realizzare acciaio pulito, ma lo vuole fare confermando la produzione a carbone. Vorremmo ricordare al ministro Urso che dalle ciminiere a carbone non usciranno mai fiori. Inoltre, il Ministro ha detto che la produzione di Taranto è fondamentale per la produzione delle auto in Italia, ma forse non sa che oggi per tutta la produzione di auto in Italia i laminati vengono dall'Asia, perché sono più convenienti e hanno la stessa qualità dell'acciaio di Taranto.

che produrre acciaio sarà sempre più difficile e oneroso. Concludo, signor Presidente, con la linea politica del MoVimento 5 Stelle, che giustifica la nostra contrarietà al provvedimento

come è dimostrato dal vostro disinteresse a proseguire quell'attività di riconversione che noi avevamo iniziato nel corso del Governo Conte II. Inoltre,

straordinaria, lavoratori di Acciaierie d'Italia, lavoratori portuali, lavoratori dell'arsenale, lavoratori della Cementir. Diciamo basta a questo suicidio di Stato. Liberiamo Taranto, perché Taranto ha la necessità

noi conosciamo le vicende che hanno attraversato e stanno attraversando gli stabilimenti di questa azienda, per i quali è intervenuto dapprima il decreto n. 4 del 2024, poi il Governo il Governo ha emanato il decreto-legge n. 9 del 2024 a tutela delle imprese dell'indotto, che ha raccolto le esigenze emerse durante oltre trenta audizioni svolte nella nostra Commissione. Per dare continuità poi ai due provvedimenti di urgenza, il Governo, con l'emendamento 2.0.1000 presentato in Commissione, ha trasfuso tutti i contenuti nel decreto-legge n. 9. Questo Governo e questo Parlamento, soprattutto la sua maggioranza, intendono assicurare una continuità produttiva ad Acciaierie d'Italia, nonché quella delle aziende dell'indotto e hanno seguito, fin dall'insediamento la vicenda, che sta duramente colpendo i lavoratori, la città di Taranto, il territorio, ma anche - non dimentichiamocelo mai - gli altri stabilimenti del gruppo: Cornigliano, Genova, Novi Ligure, Racconigi, Gattinara, Salerno, Paderno Dugnano, Legnaro. Credo non serva ricordare che l'acciaio è un *asset* strategico perché interessa tutta l'industria. Il settore siderurgico italiano è al secondo posto in Europa dopo la Germania, all'undicesimo posto nel mondo per tonnellate prodotte e Acciaierie d'Italia è il più grande impianto siderurgico italiano ed attualmente dà lavoro, come abbiamo detto più volte, a oltre 10.500 dipendenti, di cui 3.000 in cassa integrazione, 2.500 di questi solo nella città di Taranto. L'impatto dell'ex Ilva sul prodotto interno lordo del nostro Paese è di oltre lo 0,2 per cento, ma su quello del Mezzogiorno è dello 0,7 È quindi fondamentale continuare a sostenere con convinzione le sorti del gruppo, impostando un piano di recupero e progetti di rilancio affinché *player* privati possano essere interessati a investire sull'impianto. È inutile ogni volta guardare indietro, cercando le colpe di tutti quelli che ci hanno preceduti: dobbiamo guardare avanti con convinzione e con forza, se crediamo in questo settore. Il decreto va in questa direzione, include varie misure di sostegno, toccando aspetti fondamentali, in particolare - non dimentichiamolo - l'indotto. A tutela delle imprese dell'indotto, il decreto riconosce condizioni agevolate di accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ammesse, queste, alla procedura di amministrazione straordinaria. In Commissione sono stati modificati i requisiti di accesso al fondo indicando quali beneficiari le imprese che hanno prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente. In origine, la norma era rivolta a imprese che producevano oltre il 50 per cento del fatturato medio complessivo degli ultimi due esercizi ed escludeva troppe imprese. La modifica è frutto dell'approvazione di un emendamento presentato anche dal Gruppo Lega, con il quale si salvaguardano gli interessi di tutte le imprese di piccole e medie dimensioni fornitrici dell'ex Ilva. dell'approvazione di tale modifica, la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente fino alla misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90 per cento in caso di riassicurazione. Questa mi sembra una cosa molto buona. Inoltre, è previsto che per l'anno 2024 sulle operazioni finanziarie possa essere anche richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. L'effetto del contributo è dunque quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale e grazie, anche qui, all'approvazione di un emendamento presentato anche dal Gruppo Lega, sono stati raggiunti due importanti obiettivi. garantita anzitutto a tutte le imprese fornitrici la prededucibilità dei crediti, anche nel caso di soluzioni non continuative del rapporto tra la prestazione resa e l'avvio della procedura. Sono state esplicitate le prestazioni per le quali si riconosce la prededucibilità dei crediti. È un punto fondamentale. Inoltre, sempre sulla tutela occupazionale negli stabilimenti, si è intervenuti anche nei confronti dei lavoratori dell'indotto, prevedendo un'integrazione al reddito che, attualmente pari a sei settimane, potrà essere prolungata, grazie all'emendamento approvato, fino a dieci settimane. Altrettanto importante per salvaguardare produzione, messa in sicurezza e occupazione è la norma che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze possa concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo dei 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici Ilva, al fine di supportare le esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Il prestito ponte consentirà anche la gestione ordinaria dello stabilimento, gli investimenti necessari, la messa in sicurezza degli impianti, per rilanciare la produzione e attrarre investitori. È anche previsto il riconoscimento fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali, del trattamento straordinario di integrazione salariare per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000.

Il nostro lavoro va nella giusta direzione per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia. Occorre lavorare per garantire il diritto alla salute, procedendo alla riconversione ecologica del sito produttivo, ma al contempo dobbiamo tutelare lavoratori e filiere produttive di un *asset* strategico del nostro sistema produttivo. È tuttavia notizia di questi giorni - e questo è molto importante, Presidente che le banche non avrebbero intenzione di comprare i crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti di Acciaierie italiane per mancanza di garanzie. Una situazione che avrà come effetto quello di paralizzare centinaia di piccole aziende, già duramente provate dall'impossibilità di riscuotere il dovuto in termini utili alla prosecuzione dell'attività. Faccio appello allora agli istituti di credito affinché non rimangano sordi alle istanze delle piccole imprese altresì, Sottosegretario, signor Ministro, che il Governo si faccia promotore con le banche di un tavolo volto alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa *(Applausi)* che definisca le modalità di di cessione dei crediti deteriorati. Tutto questo anche alla luce dell'impegno del Governo per evitare in parte il pagamento alle banche sugli extra profitti. Il sistema bancario ce lo deve. Il Governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze degli istituti; oggi il nostro Paese si aspetta che questi ultimi facciano altrettanto nei confronti di coloro che hanno effettivamente bisogno dell'aiuto di tutti.

nota a tutti, di Taranto. Ricordo infine che l'attuale Governo ha chiesto all'Unione europea di cambiare obiettivi e modalità della politica industriale siderurgica per evitare che le imprese europee subiscano ingiustamente la concorrenza sleale di chi produce al di fuori dell'Unione senza rispettare le adeguate condizioni ambientali, sociali e di salute. abbiamo cercato di lavorare su un testo per dare continuità. Il Parlamento ha affiancato il Governo, come credo dimostrerà il il voto dei vari Gruppi parlamentari, per cercare di dare delle risposte concrete. Non dimentichiamoci dell'aspetto fondamentale: una produzione fondamentale per il nostro Paese, l'occupazione, le imprese piccole e medie, ma anche quelle un po' più grandi dell'indotto vanno tutte tutelate e salvaguardate, per una garanzia di fornitura di beni e servizi. Il voto della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è favorevole a questo provvedimento. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la lunga, lunghissima vicenda dell'ex Ilva vede chiudersi un capitolo disastroso, quello della gestione fallimentare di ArcelorMittal, e aprirsene un altro, l'amministrazione straordinaria con la nomina del commissario Giancarlo Quaranta, un uomo di industria, un professionista che ha esperienza nel settore siderurgico e al quale è d'obbligo fare gli auguri di buon lavoro. Un lavoro - voglio sottolinearlo fin da subito - che non sarà facile, perché la situazione di Acciaierie d'Italia è oggettivamente drammatica e la scelta appena compiuta con l'amministrazione straordinaria è una scelta drastica, delicatissima e densa di incognite. Basti ricordare che la produzione è precipitata ai minimi termini: meno di 3 milioni di tonnellate di acciaio, a fronte dei 5-6 milioni previsti dai piani industriali. Basti ricordare che migliaia di dipendenti sono in cassa integrazione. Basti ricordare l'assoluta assenza di liquidità e lo stato di insolvenza dichiarato pochi giorni fa dalla sezione fallimentare del tribunale di Milano. E questo - è bene ricordarlo, perché in quest'Aula ne abbiamo parlato e abbiamo approvato delle somme in precedenti decreti - nonostante le ingenti risorse pubbliche che sono state stanziate solo nell'ultimo anno. Accanto a tutto questo c'è il rischio che gli impianti, senza l'acquisto di materie prime, possano fermarsi e possano fermare la loro capacità produttiva. produttiva. Ho fatto questa premessa dicendo che non c'è dubbio che si debba voltare pagina e non c'è dubbio nemmeno sul fatto che o si riuscirà a farlo ora o non si riuscirà a farlo più. più. Va aperta una nuova fase, nella quale non si ripetano gli errori compiuti nel passato e in particolare non si ripetano gli errori compiuti nell'ultimo anno e mezzo, nel quale abbiamo assistito agli effetti di un pessimo combinato disposto, quello formato dal progressivo disimpegno di ArcelorMittal, che a Taranto ha quasi del tutto rallentato, fino a fermarsi, mentre in altre realtà all'estero invece ha corso, e dalla linea ondivaga di questo Governo. Anzi vorrei dire - come è stato ricordato anche da altri colleghi - da due diverse linee: da una parte la linea del ministro Urso, che è qui presente e che saluto, di sostanziale incapacità di incidere rispetto all'effettivo impegno di ArcelorMittal per il rilancio dello stabilimento di Taranto; dall'altra quella del ministro Fitto, che lo scorso maggio ha avviato con il socio privato una trattativa che non ha portato a nulla, se non a un *memorandum*, sottoscritto a settembre, di cui non abbiamo mai saputo termini e condizioni, nonostante le nostre ripetute richieste con interrogazioni e interpellanze in sede parlamentare. Ad accomunare queste due linee, cioè la linea disastrosa di ArcelorMittal e quella ondivaga del Governo, c'è il fatto di aver prodotto, in questo periodo, solo ritardi, incertezze *(Applausi)*, decreti di corto respiro, miopi e incapaci di affrontare le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria e occupazionale che riguardano le Acciaierie d'Italia. vale anche per il decreto di cui stiamo discutendo, che poi non è solo un decreto, ma ha visto confluire nello stesso testo due decreti. Dal 18 gennaio si sono susseguiti, non solo questi due decreti, ma un terzo quello che fa riferimento al PNRR, che è stato approvato sabato 2 marzo, relativo al fatto che vengano previsti ulteriori finanziamenti. Ciò a dimostrazione del fatto che tutto questo è avvenuto con una linea con una linea ondivaga, con una certa improvvisazione, con aggiustamenti di volta in volta. Anche i 320 milioni di prestito ponte stanziati dal decreto sono assolutamente insufficienti, come abbiamo detto nel corso dell'esame in Commissione. Così come non è abbastanza forte l'azione sul versante degli ammortizzatori sociali e su quello delle misure a sostegno delle imprese dell'indotto. Positivo, invece, voglio ricordarlo, è il via libera dato in Commissione al nostro emendamento, che consente di utilizzare parte degli avanzi vincolati di amministrazione della Regione Puglia per sostenere le imprese dell'indotto. È un fatto importante che consentirà di sbloccare quelle risorse, di soddisfare i crediti e significa assicurare la continuità produttiva, in alcuni casi la stessa sopravvivenza delle aziende, oltre che permettere, finalmente, ai lavoratori che sono in attesa da tanti mesi di ricevere le loro retribuzioni. *(Applausi)*. Altro emendamento su cui abbiamo insistito e che è stato approvato in Commissione è quello che ha introdotto l'obbligo per il commissario di redigere e comunicare al Ministero, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione dell'amministrazione straordinaria, un apposito vero e proprio piano industriale. Colleghi, questo è un punto fondamentale. Dopo, non solo le incertezze, ma anche la scarsa trasparenza di questi lunghi mesi, finalmente potremo avere a disposizione i numeri reali sullo stato economico finanziario e patrimoniale, sulla consistenza del debito, sulla platea effettiva dei creditori e sullo stato degli impianti, anche per verificare l'attuale livello di sicurezza degli impianti, la loro manutenzione, anche per la sicurezza dei lavoratori. Il piano industriale sarà indispensabile per comprendere e valutare aspetti decisivi. Il primo è capire se il settore della produzione dell'acciaio avrà ancora prospettive di ripresa e di sviluppo nel nostro Paese. Parliamo di un settore produttivo fondamentale per la nostra economia, indispensabile per il funzionamento di altri settori manifatturieri e cruciale per l'occupazione. Oggi, purtroppo, ancora ad oggi, nonostante le molte dichiarazioni, il Governo non riesce a mettere a punto un piano nazionale della siderurgia. D'altro canto, per farlo servirebbe avere una strategia, una previsione compiuta di politica industriale, cosa di cui da un anno e mezzo sinceramente non si riesce a vedere l'ombra. Il secondo aspetto è che il piano del commissario dovrà chiarire se gli stabilimenti appartenenti ad Acciaierie d'Italia saranno soggetti a spezzatino e venduti separatamente a più acquirenti. capire se verrà intrapresa la strada della *bad company* sul modello Alitalia, in particolare per lo stabilimento di Taranto, e, ancora, quale sarà il livello di occupazione e di capacità produttiva per tutti gli stabilimenti e, conseguentemente, di approvvigionamento di acciaio per il nostro sistema produttivo. Quali saranno i livelli di produzione? Questo sarà fondamentale per capire quale sarà il livello di occupazione e quello della cassa integrazione per tutti gli stabilimenti: Genova Corigliano, Novi Ligure, Porto Marghera. E rispetto all'ex Ilva di Taranto, come verrà portato a compimento il processo di decarbonizzazione? È vero, ha detto la collega Aurora Floridia, dal mio emendamento sul piano industriale è stata tolta la parte relativa l'ambientalizzazione, ma noi su questo continuiamo a insistere perché il processo di decarbonizzazione è fondamentale per garantire un'innovazione e a tutela della salute e dell'ambiente dei territori interessati. Sono tutte informazioni, quelle che ho appena sintetizzato, che, allo stato attuale, non sono disponibili, ma che nei prossimi sei mesi dovranno consentire di procedere in modo ordinato e consapevole verso un possibile rilancio degli stabilimenti industriali in amministrazione straordinaria. Di numeri e scelte trasparenti c'è bisogno. È questa la prima cosa di cui c'è davvero bisogno. È così che si possono aiutare le imprese dell'indotto; è così che si possono aiutare i lavoratori: con il procedere dell'amministrazione straordinaria e la vendita degli *asset* ai nuovi investitori. Difficoltà che di certo non mancheranno e che noi dovremo affrontare con serietà, responsabilità, lungimiranza. Un segnale importante è rappresentato dal fatto che che il commissario già nei primi giorni del suo incarico abbia voluto incontrare le rappresentanze sindacali. È bene ricordare anche in questa sede che, grazie a un nostro emendamento, è stata ripristinata la ripristinata la consultazione sindacale per la cassa integrazione: è un fatto anche questo significativo. Sarà necessario anche un confronto costante con le istituzioni locali, come nei mesi e nei giorni scorsi abbiamo chiesto proponendo la creazione di un tavolo istituzionale permanente di confronto. Signor Presidente, le questioni aperte sono grandi e decisive, come garantire innanzitutto la continuità produttiva e l'occupazione e come creare le condizioni perché nuovi soci privati possono entrare in questa realtà. Le possibilità di ripartenza passano da qui: confronto, visione, assunzione comune di responsabilità. Noi, da parte nostra, ci mettiamo il nostro contributo, lo abbiamo messo nel lavoro in Commissione e siamo disponibili a dare una mano. Anche il nostro voto di astensione su un decreto-legge di cui pure vediamo tutti i limiti, che abbiamo messo in evidenza nei mesi precedenti, vuole essere un segnale in questo senso. Certo è, però, che nel merito delle scelte che farete, come anche rispetto a tutte quelle che non avete ancora compiuto, continueremo a non farvi sconti proprio in nome dell'interesse nazionale, per il bene del nostro Paese che merita molto di più...

oggi in Aula stiamo discutendo uno dei *dossier* più complessi che come Nazione siamo chiamati ad affrontare. Ereditiamo purtroppo uno scenario desolante che richiama per più aspetti quello del 2015. L'impegno che il Governo Meloni, del ministro Adolfo Urso e di tutta la maggioranza è quello di non ripetere gli errori del passato *(Applausi)* e di vagliare tutte le possibili opzioni per il risanamento e il rilancio di uno stabilimento ritenuto strategico non solo per il territorio pugliese, in sofferenza ormai da tempo, ma per l'intero sistema Paese. Per la seconda industria manifatturiera d'Europa, la siderurgia non può che essere ritenuta strategica. Parliamo di 20.000 lavoratori e di tantissime imprese dell'indotto sul cui futuro si è stagliata un'ombra a causa di una politica industriale spesso anche scellerata, che ha ridotto in condizioni deprecabili lo stabilimento a ciclo integrale più grande di Europa. Che ciò sia frutto di una precisa volontà di avvantaggiarsi sullo scenario internazionale grazie ad investimenti maggiormente remunerativi e più d'avanguardia, magari in Francia, non è nostro compito definirlo. A questa Assemblea e alla parte coscienziosa del Paese spetta invece il compito di trovare soluzioni concrete ed efficaci per rilanciare le produzioni, per garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie del sito produttivo a beneficio dei cittadini del territorio tarantino, della loro salute e dell'ambiente in cui vivono *(Applausi)*, nonché per tutelare i tantissimi lavoratori frenando il processo distruttivo in atto e per salvaguardare la continuità produttiva. Riteniamo ancora possibile, infatti, produrre acciaio in modo responsabile ed efficiente, seppure in una situazione a dir poco complessa e ingarbugliata, in cui tante decisioni ereditate dal passato rappresentano oggi dei macigni di difficile trattazione, ma su cui invece il Governo Meloni sta imponendo la propria impostazione risolutiva. Soluzioni che in parte ritroviamo nel testo che ci accingiamo ad approvare. Infatti, come è noto, la scelta certamente difficile, ma assolutamente necessaria per il lancio dello stabilimento è stata quella dell'amministrazione straordinaria di un'impresa che questo Governo ritiene assolutamente strategica non solo per il territorio pugliese, ma anche per l'intero sistema Paese. Con questa decisione riusciamo ad evitare pertanto che gli ordinari strumenti del codice della crisi siano utilizzati a fini dilatori. Avevamo dinanzi un bivio: o rischiare un ulteriore procrastinarsi di una fase di stallo a danno della produzione industriale, delle tante imprese dell'indotto e dei numerosi lavoratori dello stabilimento, oppure agire per ripartire. All'inerzia abbiamo preferito l'azione, come nostra caratteristica *(Applausi)* e come dimostriamo ogni giorno su tanti *dossier* differenti, dai più semplici ai più complessi, come quello che stiamo affrontando anche oggi. Una scelta che ha trovato conferma ulteriore nelle decisioni del tribunale di Milano, che si è espresso nelle scorse settimane. E dopo aver definito le modalità con cui procedere alle operazioni di rilancio del sito produttivo tarantino, il ministro Urso ha provveduto a finalizzare la nomina dei commissari: Giancarlo Quaranta, già nominato commissario straordinario di Acciaierie d'Italia lo scorso 20 febbraio, è stato dunque affiancato dal professor Giovanni Fiori, esperto di *corporate governance* e *internal auditing*, e dal professore Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia ed esperto di tematiche ambientali. Come si può osservare, profili autorevoli in grado di guidare i prossimi passi, ad iniziare da ciò che ci hanno ribadito tutte le associazioni delle imprese audite negli approfonditi lavori della Commissione industria, voluti dal presidente Luca De Carlo, che ringrazio. Evitare il 2015 è stato praticamente il *mantra* che ci è stato ripetuto in queste settimane: il riferimento è ovviamente ai 150 milioni di euro andati in fumo, un'ipotesi per noi inconcepibile, che ha trovato risposta nella possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze conceda uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici tarantini. Ciò al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A questi fondi si aggiungono altri 150 milioni di euro che lo Stato concede per il tramite dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Anche qui il ministro Urso ha provveduto al rinnovo dei commissari, nominando il professor Francesco Di Ciommo, esperto di diritto bancario e finanziario, delle crisi di impresa e di diritto amministrativo e societario, e la dottoressa Daniela Savi, esperta in gestione della crisi di impresa in materia fiscale, nonché ha confermato il professor Alessandro Danovi, già commissario della procedura ed esperto di risanamento di impresa, gestione dell'insolvenza e operazioni straordinarie. L'approccio teso alla migliore risoluzione possibile della faccenda lo si denota dalla novità normativa introdotta in Commissione, con cui si permette alla Regione Puglia di utilizzare avanzi finanziari per sostenere le imprese dell'indotto, nel rispetto della direttiva europea in materia di aiuti di Stato, oggetto di attente valutazioni da parte dei Ministeri competenti. Siamo intervenuti poi nella cassa integrazione straordinaria, estendendo ulteriormente il periodo, sino a dieci mesi, con un emendamento d'Aula del presidente De Carlo, sui parametri di accesso al fondo di garanzia, nonché sul perimetro delle imprese interessate dai sostegni economico-finanziari, proprio perché consci di quanto sia determinante l'impatto dello stabilimento su tutto il territorio tarantino e non solo. La salvaguardia di ciò che oggi continuiamo a poter avere, la preservazione della speranza che si possa ancora fare acciaio e lo si possa fare in maniera sempre più attenta ai risvolti ambientali, a beneficio della popolazione che con il sito produttivo vive e convive lo dobbiamo alle tante micro e piccole imprese e ai lavoratori che non hanno mai smesso di pensare al futuro. A loro sono stati demandati non solo i trasporti e le pulizie, ma anche gran parte delle attività manutentive ordinarie e straordinarie, tutta la messa in sicurezza e gli interventi di bonifica e di materia ambientale. A questa gente vanno il nostro pensiero e tutte le nostre attenzioni. A chi ha perpetrato politiche industriali intrise di abbandono, silenzi e inazione, auguriamo comunque il meglio, ma assolutamente lontano dalla nostra gente e dalla nostra terra. Il Governo e il Parlamento continueranno a fornire tutto il supporto normativo e di risorse necessarie a questo stabilimento strategico per l'intera Nazione e che da pugliese mi sta particolarmente a cuore. Saremo vicini ai commissari neonominati, a cui non faremo mai mancare il nostro supporto. Li attendono mesi cruciali, in cui dovranno elaborare soluzioni non semplici, come dimostra il confronto in corso con Sace e gli istituti bancari, nonché un piano industriale triennale con cui si possa finalmente risanare e rilanciare lo stabilimento tarantino, proiettandolo nel futuro con scelte strategiche, efficaci e intelligenti, per garantire innovazione e produttività. Riteniamo che la strada tracciata sia la migliore per giungere a soluzioni concrete per i lavoratori, i cittadini e l'intero territorio tarantino: chiarezza di analisi, determinazione e lucidità d'azione.

Credo che il Senato voglia esprimere congiuntamente un grande augurio a tutte le nostre senatrici e a tutte le donne del mondo